Comunico che in data 7 maggio 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR* «Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materie di politica di coesione» "Il link apre una nuova finestra") ***Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente

onorevoli colleghi, si sottopone all'esame dell'Assemblea il disegno di legge costituzionale n. 935 di iniziativa del Governo, come è risultato dalle modifiche accolte dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente. A seguito degli emendamenti approvati, il disegno di legge si compone di otto disposizioni e interviene sugli articoli 57, 59, 83, 88, 89, 92 e 94 della Costituzione. In particolare l'articolo 1, al quale la Commissione ha apportato una mera specificazione nella rubrica, abroga il secondo comma dell'articolo 59, ossia la previsione in base alla quale il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, in un numero complessivo non superiore a cinque, cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti. L'articolo 2, introdotto dalla Commissione, modifica l'articolo 83, terzo comma, della Costituzione prevedendo che l'abbassamento del *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, ossia da due terzi alla maggioranza assoluta, operi non più dopo il terzo scrutinio, bensì dopo il sesto scrutinio. L'articolo 3, comma 1, interviene sul primo comma dell'articolo 88, sopprimendo la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle Camere. Per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione, è stato aggiunto un ulteriore comma che modifica il secondo comma del medesimo articolo 88 della Costituzione, Costituzione, laddove si deroga al divieto di scioglimento delle Camere nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica (il cosiddetto semestre bianco). Il testo vigente dell'articolo 88, secondo comma, prevede infatti che il Presidente della Repubblica non possa sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. La modifica proposta dalla Commissione stabilisce invece che il divieto di procedere allo scioglimento delle Camere nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica non trovi applicazione nei casi in cui lo scioglimento costituisca un atto dovuto. L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce interamente il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione, in materia di controfirma degli atti del Capo dello Stato, stabilendo che, in linea generale, gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Si prevede altresì che non necessitino di controfirma una serie di atti, ossia la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia, la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei *referendum*, i messaggi alle Camere, il rinvio delle leggi alle Camere. L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce l'articolo 92 della Costituzione, mantenendo inalterato il primo comma, ai sensi del quale il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Si introduce poi la previsione dell'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri a suffragio universale e diretto per cinque anni, fissando un limite al numero dei mandati. Infatti si stabilisce che il Presidente del Consiglio possa essere eletto per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Si dispone altresì che le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio abbiano luogo contestualmente. Si rinvia invece alla legge la disciplina del sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo l'assegnazione di un premio su base nazionale che garantisca, in ciascuna delle Camere, una maggioranza dei seggi alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio eletto, fermo restando il rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche. Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera nella quale abbia presentato la sua candidatura. In base all'ultimo comma del nuovo articolo 92, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio eletto e, su proposta di quest'ultimo, nomina e revoca i Ministri. La revoca è stata aggiunta con un emendamento approvato in Commissione, per specificare che al Presidente della Repubblica compete anche questo potere. L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame in Commissione, integra il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, prevedendo che il principio dell'elezione a base regionale del Senato debba comunque far salvo, oltre ai seggi assegnati alla circoscrizione estero (come previsto dal testo vigente), anche il premio su base nazionale di cui all'articolo 92 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 5 del disegno di legge costituzionale. L'articolo 7, nel testo risultante dall'esame in Commissione, modifica l'articolo 94 della Costituzione. In particolare, la lettera *a)* sostituisce il terzo comma. Mentre rimane invariata la previsione secondo cui, entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia, si introduce una nuova disposizione in base alla quale, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in questo caso il Governo non ottenga la fiducia, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere. La lettera *b)* aggiunge infine tre ulteriori commi, ai sensi dei quali, in caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio dei ministri eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. In caso invece di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora il Presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. Tale ultima possibilità è prevista anche nel caso di morte, impedimento permanente o decadenza del Presidente del Consiglio eletto. L'articolo 8 reca due norme transitorie. Al comma 1 si prevede che restino in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione nel testo previgente, alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Il comma 2, al quale la Commissione ha apportato una modifica meramente formale, stabilisce infine che la legge costituzionale si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle

finestra"). Saluto studenti e docenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari. Benvenuti in Senato.

Signor Presidente, quest'Assemblea ha già visto la discussione di questioni pregiudiziali sia in questa legislatura che in quelle passate. Qui ci troviamo di fronte però ad una questione pregiudiziale peculiare particolarmente grave. Si tratta dell'incostituzionalità di una legge costituzionale; sembra un paradosso, quasi una cosa impossibile, eppure è esattamente ciò di cui quest'Aula sta per discutere e il provvedimento che nelle prossime ore, molto probabilmente, ci troveremo ad affrontare. L'incostituzionalità delle leggi di eventuali modifiche incostituzionali

italiana ha affermato che «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i princìpi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede, come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i princìpi che, pur pur non essendo espressamente menzionati tra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana». Questa è la Corte costituzionale, nei cui confronti mi auguro che anche l'attuale maggioranza e il presente Governo ancora nutrano una qualche forma di fiducia. Perché affermiamo a gran voce che questa modifica della nostra Costituzione repubblicana è incostituzionale? Il Governo si è vantato di agire su pochissimi articoli e, attraverso questo messaggio, vuole far credere all'opinione pubblica che si tratta quindi di modifiche minimali. No, si tratta di cariche esplosive piazzate sotto gli architravi portanti dell'intera struttura della nostra Costituzione. In che modo? La separazione dei poteri; capisco che lì fuori questi discorsi possono risultare forse poco comprensibili, ma io qui mi rivolgo invece ad onorevoli senatori e senatrici e al Governo che dovrebbero sapere esattamente il significato delle parole parole e dei poteri. La separazione dei poteri viene assolutamente a mancare, anzi, viene sovvertita perché la nostra Costituzione, per quanto possa sembrare strano nei tempi che corrono, ha posto il Parlamento - espressione diretta del popolo sovrano - al di sopra del Governo. Con questa mini riforma letale della nostra Costituzione voi sovvertite questo rapporto e mettete il Governo al di sopra del Parlamento e il Parlamento al guinzaglio del Governo, anzi al guinzaglio di una sola persona, quella eletta direttamente dal popolo non si sa ancora bene come. Questo perché di incostituzionale, o quantomeno di inusuale, c'è anche la scarsa chiarezza di questo testo, che pure viene presentato in quest'Aula. Come avverrebbe l'elezione diretta del *Premier*? «Contestualmente», qualunque cosa questo avverbio, poi, nella pratica, nelle urne e in sede elettorale, significhi. È un salto nel buio, quindi, a cui costringete questa Assemblea e l'intera Nazione, che evidentemente non vi sta così a cuore come Giorgia invece afferma. Come dicevo, il Parlamento sarà messo al guinzaglio del potere di una sola persona, quindi con una sovrapposizione dei poteri assolutamente incostituzionale. Ma vediamo cos'altro c'è di incostituzionale in questa riforma. Voi affermate che in questo modo date maggiore potere al corpo elettorale, che finalmente potrà scegliere chi è a capo del Governo.

del Presidente del Consiglio. Ebbene, anche qui la risposta ci viene proprio dai costituzionalisti: perché il potere del corpo elettorale si riduce all'esercizio di una sola volta ogni cinque anni, senza possibilità di avere alcun tipo di rappresentanza, che dovrebbe invece essere espressa nel Parlamento, perché questo è il luogo della rappresentanza popolare. Vi è poi l'accentramento dei poteri

un premio di maggioranza non meglio definito e questo è un altro *vulnus* di questa modifica costituzionale, è un'ipoteca sul futuro politico del Paese, in quanto costringerete in via costituzionale il Paese ad avere un sistema forzatamente maggioritario e questa è assolutamente una una forzatura. Il corpo elettorale si potrà esprimere, quindi, una volta ogni cinque anni, indicando il capo che accentra potere di vita o di morte sul Parlamento. Lo scioglimento delle Camere,

crisi istituzionali che si possono aprire, passa completamente in capo al Presidente del Consiglio, esautorando quindi il Presidente della Repubblica e voi sapete bene che affermate il falso quando dite che non ne toccate i poteri perché andate a colpire al cuore i poteri rappresentativi principali della funzione e del ruolo del Presidente della Repubblica, che da arbitro diventa esclusivamente spettatore, e non potrà più intervenire in alcun modo. C'è di più, perché dobbiamo denunciare anche il fatto che voi

e si elegge il *premier* contestualmente alle Camere parlamentari? Non funziona così da nessuna parte, noi dobbiamo smentire anche questa falsità per cui si ripete che succede altrove. Non è così, perché altrove c'è il presidenzialismo o il semi-presidenzialismo e le elezioni avvengono

tutte le materie che vogliono. Noi potremmo avere ipoteticamente 20 Regioni con 20 tipi di competenze diverse: non è uno Stato arlecchino, è anarchia assoluta. In quest'Aula è stato lo stesso presidente della Commissione affari costituzionali Balboni, un noto esponente della maggioranza e di Fratelli d'Italia, a denunciare in più occasioni lo strapotere del Governo e di come del Governo e di come l'abuso della decretazione d'urgenza umili il Parlamento. Con questa riforma istituzionalizzate l'umiliazione del Parlamento, che non avrà più alcun tipo di potere, perché lo depauperate dall'alto, attraverso l'accentramento dei poteri nel Governo e in una persona sola, e dal basso, con l'autonomia differenziata e quindi il deferimento delle competenze ai governatori. Fermatevi, perché questa riforma è incostituzionale.

dei tanti rilievi di incostituzionalità che arrivarono inizialmente dalla stragrande maggioranza dei costituzionalisti intervenuti in audizione e che hanno analizzato il testo proposto dal Governo, l'Esecutivo, come ben sappiamo, l'Esecutivo, come ben sappiamo, ha deciso di presentare quattro emendamenti che hanno sostanzialmente riscritto il contenuto di questa riforma, senza però riuscire a risolvere i gravi problemi di illegittimità costituzionale che erano stati evidenziati fin dall'inizio. una prima questione che attiene addirittura alla formulazione tecnica e formale del disegno di legge. Questa riforma fa nascere - ma lo vedremo certamente nel corso dei mesi che verranno, se malauguratamente dovesse essere approvata - una serie di equivoci, di difficoltà interpretative e io credo, noi crediamo, che ciò costituisca, quando si parla di un testo di revisione costituzionale, un difetto davvero insuperabile. Eppure i costituenti ci hanno consegnato un testo scritto con parole molto accurate, che è stato oggetto di studio da parte dei migliori giuristi dell'epoca, analizzato addirittura dai letterati del tempo, proprio a dimostrazione che quando si mette mano alla Costituzione, bisogna farlo nella maniera migliore possibile. Oltre a questo, il testo disegnato con sapienza dai Padri costituenti è davvero - e credo che questo sia uno dei punti decisivi anche della discussione di stamattina - un esempio mirabile di equilibri, di pesi e di contrappesi sui quali, con ogni evidenza, voi invece pensate di poter intervenire a colpi di accetta, tagliando qua e là in maniera molto maldestra, con l'unico obiettivo di accentrare più potere possibile nella figura del Presidente del Consiglio, incuranti quindi di preservare quegli equilibri costituzionali, quei contrappesi che hanno consentito in tutti questi anni al nostro Paese e alla nostra democrazia di diventare effettivamente una democrazia parlamentare. L'obiettivo di questa riforma è soprattutto quello di depotenziare il Parlamento, che viene completamente svuotato della sua centralità e che, da organo di massima rappresentanza del popolo che lo elegge, diviene in questo disegno di revisione costituzionale del tutto ancillare rispetto al Presidente del Consiglio, titolare invece, quello sì, di un potere davvero smisurato che gli deriva direttamente dall'investitura popolare. Io insisto molto su questo punto, perché il provvedimento in discussione, come sappiamo e come abbiamo detto tante volte in quest'Aula, viene portato avanti contestualmente al provvedimento sull'autonomia differenziata, che abbiamo esaminato in questo Senato nei mesi scorsi e che oggi è alla Camera. due provvedimenti che sembrano ispirati da logiche addirittura opposte (il massimo accentramento di potere da una parte, il massimo decentramento invece dall'altra), ma che hanno in comune esattamente questo punto, cioè la totale marginalizzazione del Parlamento e questo mi pare evidentemente un problema di prima grandezza. L'altro obiettivo, poi, è il Presidente della Repubblica. Anche qui, senza girarci intorno, privato di ogni discrezionalità, ridotto a mero organo ratificante delle decisioni del Governo. Voi cancellate i pesi, i contrappesi, gli equilibri stabiliti dal costituente per difendere questo Paese, questa Repubblica, questa democrazia da tutti i rischi, anche quelli di possibili torsioni non democratiche. Rischio reale, purtroppo, anche e soprattutto adesso, a causa della fragilità delle democrazie contemporanee, che sono oggi prive della solidità di quei corpi intermedi attorno ai quali si è determinata per decenni la partecipazione democratica e sono quindi esposte molto più di prima a lacerazioni potenzialmente molto pericolose. Questa riforma non ha davvero nulla di chirurgico. Essa interviene sull'attuale impianto generale della stessa forma della democrazia parlamentare posta a fondamento della nostra Costituzione, tanto da indurre tutti gli auditi che sono stati ascoltati dalla 1ª Commissione, anche quelli ascoltati per ultimi, dopo le modifiche che sono intervenute, a definire del tutto inaccettabile e inemendabile questo disegno di legge costituzionale: non solo per la sua inadeguatezza tecnica, ma anche per il suo contrasto con i principi che reggono le basi della nostra democrazia rappresentativa. La premessa a tutte le critiche è sempre la stessa. Contrariamente, infatti, a quanto viene affermato, questa riforma non interviene chirurgicamente soltanto su alcuni articoli della Carta costituzionale. investe il nucleo centrale della nostra forma di governo e finisce per colpire l'intero impianto repubblicano nel suo insieme, cioè il quadro esatto dei poteri e delle libertà tracciato dal costituente, imprimendo a questo impianto una curvatura totalmente diversa da quella attuale. Tale curvatura, dal nostro punto di vista, è inaccettabile, perché ribalta il principio che regge le fondamenta del nostro vivere comune. Con la Carta del 1948 i nostri costituenti intesero, dopo l'esperienza autoritaria, costruire una democrazia fondata sul pluralismo, assegnando in questo modo la sovranità popolare al Parlamento. Si ritenne allora, dopo un'analisi molto approfondita del sistema politico, che questa forma di governo, quella parlamentare, fosse la più adatta a favorire la convivenza pacifica e lo scambio tra le diverse forze in campo che si contrapponevano e che erano, per l'appunto, espressione di un sistema politico caratterizzato da un livello molto elevato di frammentazione e di conflittualità. Forma di Governo parlamentare, la nostra, fondata sull'equilibrio tra una funzione di indirizzo politico, affidata alla maggioranza ed esercitata attraverso il raccordo con il corpo elettorale, con il Parlamento e il Governo, ed una funzione di controllo costituzionale, affidata, invece, a organi imparziali, espressione dell'unità nazionale, quali il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Questo equilibrio, attorno al quale si è determinato e si è costruito il principio decisivo della separazione dei poteri, oggi viene messo totalmente in discussione. Ad essere violati sono i princìpi stessi della rappresentanza politica, stritolati tra la pretesa della legge maggioritaria come panacea capace di curare l'instabilità del sistema politico e la necessità di vincolare il *Premier* e la sua maggioranza in un legame davvero indissolubile. Legame che ci fa parlare di un Parlamento che sarà eletto per trascinamento, che contrasta, secondo noi, esso stesso con la funzione del mandato parlamentare, anche in questo caso in palese ed evidente contrasto con la Costituzione repubblicana. Altro tema è quello del sistema di fiducia, della sfiducia, delle dimissioni, degli impedimenti di varia natura del futuro Presidente del Consiglio. Avete creato un sistema così complicato che darne una interpretazione certa diventa molto difficile. Poi c'è la questione della legge elettorale, il totale pasticcio degli italiani all'estero, che è stato giustamente sottolineato in tante audizioni. Soprattutto, ciò che è del tutto illegittimo è proprio la compressione dei poteri e del ruolo del Presidente della Repubblica - da una parte - e il contestuale accentramento dei poteri nella figura del Presidente del Consiglio, accompagnato dall'assenza totale di contrappesi - dall'altra - in questo caso in maniera molto diversa anche dai Paesi

che adesso ho espresso e che naturalmente esprimeremo anche nel corso delle prossime settimane nella discussione generale e poi quando illustreremo gli emendamenti, vi diciamo di fermarvi e di non procedere oltre con questa riforma illegittima, totalmente sbagliata e segno di una totale regressione politica, ma anche culturale, che riteniamo produrrebbe la distruzione di quel sistema delle garanzie e dei contrappesi che sono stati ritenuti indispensabili dai Costituenti e che rischiano oggi di essere profondamente alterati. Cambiare così la nostra Costituzione in una logica che rifiutiamo, contraria ai princìpi ispiratori della nostra Repubblica, a noi sembra un atto davvero scellerato. Cominciamo oggi con questa questione pregiudiziale un percorso lungo, che ci vedrà contrapporci

ne violi di fatto i princìpi fondanti, chiaramente espressi e richiamati soprattutto nella Parte I della nostra Costituzione. Vi è poi una ragione politica accorata, che sentiamo di dover sottolineare in queste ore e settimane, dopo peraltro la quasi approvazione alla Camera del disegno di legge sull'autonomia differenziata, che ci spinge a chiedervi di fermarvi: state smantellando l'impalcatura istituzionale e costituzionale del nostro Paese, minandone le fondamenta e soprattutto le ragioni che ci hanno visto insieme e ci hanno visto forti in una Repubblica parlamentare per tanti anni. Direi di partire da un'operazione verità: avete chiamato con un titolo roboante, fatto di tante parole, una cosa che poteva essere chiamata in maniera molto più semplice, ossia abolizione del sistema della Repubblica parlamentare, istituzione della Repubblica del *Premier*. stato più onesto, più diretto e più trasparente. Prima però di parlare delle ragioni per cui - a nostro avviso - in questa questione pregiudiziale proviamo chiaramente a dirvi perché violate i princìpi fondanti della Parte I della Costituzione, voglio fare due premesse, che sono state esplicitate dai miei colleghi quando luogo, questo disegno di legge definisce un *unicum* nel quadro e nel sistema mondiale dei sistemi costituzionali dei Paesi, nessun Paese al mondo escluso. Ci verrebbe da chiederci una cosa e facciamoci una domanda: facciamoci una domanda: certo, si può essere sempre i primi, ma forse qualche ragione ci sarà se anche chi l'ha approvata è stato costretto a tornare indietro. di un disegno di legge di natura governativa per mandare a casa in soffitta il parlamentarismo, quindi una Repubblica costruita sul protagonismo del Parlamento, e affermare il protagonismo del *Premier*: una ragione in più per riflettere, forse, e fermarsi. È questo il nostro appello a voi e al senso di responsabilità: capiamo la bramosia di dire «abbiamo vinto e comandiamo noi», perché di questo si tratta, si tratta, ma rivolgiamo alle istituzioni che rappresentate un appello al vostro senso di responsabilità. E qui vengo al primo degli articoli che ho richiamato e nel solco del quale avete varato sicuramente questo disegno di legge di modifica della Carta costituzionale, ma che violate nel fondo e alla radice nei suoi principi, ossia l'articolo 138.

così chiaramente nella nostra Carta costituzionale? Perché è la radice stessa della nostra Costituzione, scritta all'indomani di pagine tristi della nostra storia, che si è provato a chiudere, suggellare e mettersi alle spalle, spalle, chiedendo a tutti di contribuire a scrivere una Carta, chiedendo e credendo nel pluralismo e nelle differenze come una grande ricchezza. questo spirito: lo avete tradito in Commissione in questi mesi e lo state tradendo in quest'Aula. Non siete stati attenti ai nostri emendamenti e nemmeno alle ragioni, non alle nostre, ma a quelle che coloro che vi dicevano chiaramente che il vostro è un disegno di legge il vostro è un disegno di legge sbagliato, che prevede un sistema che non esiste; proviamo a costruirne uno alternativo e ci mettiamo a disposizione. Non solo, lo avete fatto anche quando abbiamo provato a emendare nel merito e a mettervi di fronte a contraddizioni di un sistema. Penso, in modo particolare, ai temi del voto degli italiani all'estero e di una maggioranza messa in Costituzione senza una soglia. Anche di fronte a palesi contraddizioni, difficoltà e incoerenze, non avete dato alcuna risposta e vi siete mostrati allergici al confronto, tradendo lo spirito dei nostri Padri e delle nostre Madri costituenti. In nome della

che apportare modifiche alla Carta costituzionale a maggioranza non premia ed è sbagliato, ma forse è coerente con l'allergia che dimostrate al confronto democratico, ai sistemi democratici e alle differenze. Del resto, il dibattito sul sistema pubblico di informazione di queste ore forse ci ricorda il modo che avete di stare - o che scegliete di praticare - nel confronto con le altre forze e con le differenze di pensiero e cultura politica.

nelle contraddizioni, nei veti e nei contro veti della vostra maggioranza. E così avete costruito un disegno di legge pasticciato, incoerente e non omogeneo, fatto e riscritto più volte per tentare in qualche modo di accontentare parti della maggioranza, probabilmente senza riuscirci. Vengo ora alla seconda parte

Inoltre, l'articolo 139 si lega evidentemente all'articolo 1, ai sensi del quale la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione. La vostra risposta sarà: ma noi stiamo cambiando la Costituzione e prevediamo un'altra forma di esercizio della sovranità. Mi voglio allora soffermare su questa sovranità che voi pensate o dite, con un grande *bluff*, di dare al popolo. Vediamo come date questa sovranità al popolo. Anzitutto, chiedete una delega in bianco, perché dite: cittadini, venite a votare che poi ce la vediamo noi; voi state tranquilli che per tutto il tempo della legislatura ce la vediamo noi. Minate alla radice

e sconquassare il sistema costituzionale e istituzionale dell'architettura del nostro Paese. Eppure la Costituzione - ci è stato sempre detto - andrebbe maneggiata con cautela, mentre voi vi siete approcciati a tutto questo con nessun tipo di cautela, ma con arroganza, prepotenza e prevaricazione non solo del rispetto delle minoranze, ma anche di quel sano pluralismo di cui è espressione madre il Parlamento italiano. Allora calpestate equilibri, pesi e contrappesi, minate il sistema delle garanzie

Governo e Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica vedrà ridotti i propri poteri. Anche qui nessuna operazione verità: ci siamo sentiti dire per settimane che non vengono toccati i poteri del Presidente della Repubblica. Non si capisce come si fa a fare un'affermazione di questo tipo, se di fronte alle crisi parlamentari, di fronte alle crisi di Governo, di fronte alla nomina di un *Premier*, di fronte allo scioglimento delle Camere, questi poteri saranno naturalmente inevitabilmente ridimensionati, se non addirittura resi automatici e, quindi, privi di qualsiasi margine di discrezionalità e di possibilità di intervento. Vi chiediamo: se siete così convinti della vostra riforma, almeno perché non dite parole di verità?

il Parlamento a traino del Presidente del Consiglio è una scelta scellerata e irresponsabile. Lo è nella misura in cui il Parlamento del vostro disegno di legge nascerà, vivrà e morirà a seguito e per mano del Presidente del Consiglio. Allora, se il tema era risolvere la crisi del parlamentarismo, perché non mettere mano a quella che è la vera ragione della crisi? crisi? Pensiamo a come viene trattato oggi il Parlamento: diamo più dignità al Parlamento e soprattutto diteci come eleggete il Parlamento. *(Applausi)*. Lo dovevate dire adesso, ve lo abbiamo chiesto, ma avete ignorato questa richiesta a più riprese. È una legge elettorale che non dice come come vengono eletti i parlamentari, come scatta un premio di maggioranza, addirittura senza soglia, in barba ai princìpi dettati dalla Corte costituzionale: soprattutto non dice come si costruiscono quel pluralismo e quelle libertà che sono garanzia e sale della democrazia. Si poteva fare qualcosa in più, mettendo mano sicuramente a una legge elettorale, ma soprattutto affrontando di petto la crisi della partecipazione democratica, di cui all'articolo 49 della nostra Costituzione; una riforma dei partiti, che sono il sale della democrazia, perché corpi intermedi che aiutano a costruire un processo democratico. Ci avete per settimane detto che il principio di riferimento erano le Regioni: io vi dico che il 50 per cento degli aventi diritto oggi vota nelle nostre elezioni regionali. Se di fronte a un astensionismo così alto prendete quello a modello

cosa ne sarà della nostra democrazia? Allora, chiudo chiedendovi: per favore, fermatevi ed esercitate con dignità e onore, ma soprattutto con senso di responsabilità, la funzione che gli elettori vi hanno concesso.

grazie ai colleghi che hanno illustrato le pregiudiziali e grazie al Governo che è presente, con la ministra Casellati, in questa discussione.

le forze democratiche che si esprimono in questo Parlamento hanno ritenuto che fosse arrivato il momento di riflettere sulla nostra forma di governo e come si arriva alla sua formazione. Non

su questo tema essenziale, inteso proprio come forma di elezione diretta, ovviamente Italia Viva è favorevole alla riforma. Ne condividiamo la *ratio*, ne condividiamo l'essenza e ne condividiamo anche la funzione, che è quella di superare l'attuale forma con la quale si arriva alla formazione del Governo, attribuendo ai cittadini un potere diretto di elezione del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò perché è evidente perché è evidente che c'è una necessità - e anche da parte dell'elettorato c'è una richiesta in tal senso - di aumentare la capacità rappresentativa, di aumentare la possibilità per i cittadini di scegliere il proprio rappresentante, di scegliere colui al quale affidare le sorti del Governo e consegnare la responsabilità di realizzare il programma per il quale si presenta alle elezioni e chiede di essere votato. È ovvio che in quest'Aula nessuno può negare o può fingere di non sapere che la prassi parlamentare italiana ha portato a numerosi Governi tecnici, Governi tecnici, che sono nati sulla scorta di crisi di fiducia che si sono poi ricomposte attraverso l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione del Presidente della Repubblica, e di formazioni di alleanze all'interno del Parlamento che lo hanno sostenuto. Molto spesso, però, le alleanze che si formavano in Parlamento dopo le crisi e dopo l'intervento del Presidente della Repubblica erano del tutto diverse rispetto a quelle che avevano portato alla formazione del Governo originario; c'erano degli stravolgimenti, delle modifiche che gli elettori non sopportano, che gli elettori scoraggiano e che ritengono essere un tradimento dell'espressione del loro voto. Non è vero che gli elettori non sono in grado di capire la portata di questa riforma. Al contrario, gli elettori ritengono - e condannano la politica, anche noi - che, quando si va al voto e si esprime con chiarezza una preferenza, com'è l'espressione del voto, del voto, tale preferenza poi debba trovare la sua esplicazione nel Governo e nell'attività parlamentare che si svolge successivamente. Tutti gli stravolgimenti, i Governi tecnici, le nomine del Presidente del Consiglio dei ministri ad opera del Presidente della Repubblica, le consultazioni e le formazioni di nuove maggioranze allontanano l'elettorato dalla politica. In queste forme l'elettorato non si riconosce più, perché dice di aver votato qualcuno e poi governa qualcun altro, e ciò non gli sta bene. Questa è una prassi che la nostra Repubblica conosce in maniera direi invalsa; come si suole dire, è una prassi che ormai è invalsa nell'uso. nell'uso. Sull'essenza di questa riforma, Italia Viva è d'accordo e ritiene che sia il momento di farla, di portarla avanti. Non siamo d'accordo invece sulle modalità con le quali tale riforma vuole essere portata avanti e attuata dal Governo. È un disegno di legge che non ci convince per tanti aspetti, per tante lacune che lascia aperte e perché introduce una riforma senza avere riguardo all'organo sistematico con cui si deve poi attuare una riforma costituzionale. Non si possono introdurre - come ha detto il relatore, il senatore Balboni - poche modifiche concentrate in pochi articoli e pensare che questo valga la bontà della riforma. Al contrario, dato il testo sul quale stiamo intervenendo e dato che incidiamo direttamente sulla nostra forma di governo, abbiamo ritenuto - e lo abbiamo rappresentato più volte in Commissione - che una riforma del genere debba far parte di una più organica, a partire

che fa operare una Camera mentre l'altra si deve limitare a ratificare i provvedimenti. È ciò che ci è successo fino alla settimana scorsa sul decreto-legge sul PNRR.

il diniego del Governo e della maggioranza, con una risposta che ci ha anche un po' mortificato nel nostro lavoro. Ci è stato detto: «Sì, l'emendamento è buono, ci piace, sarebbe anche il caso di discuterne, ma non è questa la sede».

È davvero un approccio inaccettabile. Altra espressione di un approccio che non si può condividere e che certamente ci rende contrari al disegno di legge in esame, nella formulazione con cui sta arrivando in Aula, è il fatto che venga inserito nella riforma un richiamo espresso alla legge elettorale, che addirittura nel testo originario prevedeva anche l'indicazione della percentuale da raggiungere per il premio di maggioranza, originariamente fissata al 55

prevedendo che sulla base di tale legge avverrà l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e delle due Camere - quindi si sta introducendo un principio per il quale evidentemente ci saranno tre elezioni, quella del Presidente del Consiglio dei ministri, quella della Camera e quella del Senato - non si può pensare di portarle avanti senza portare avanti anche la legge elettorale. È impossibile ed è soprattutto illogico e incoerente *(Applausi)*, perché si pretende di far votare una legge alla cieca. Sono tanti i punti rimasti irrisolti nell'ambito dell'esame che è stato condotto in Commissione e del dibattito che abbiamo svolto. Quanto sarà questo premio di maggioranza? Nessuno lo sa. Sarà previsto un eventuale ballottaggio fra i migliori due candidati? Non si sa, sono voci: forse sì, forse no. Come saranno poi distribuiti i seggi? Ci sarà un effetto trascinamento? Cosa ne sarà del voto degli italiani residenti all'estero? Sono tutti quesiti che sono rimasti irrisolti. La legge elettorale nel dibattito che abbiamo svolto in Commissione su questa riforma ha fatto la parte del convitato di pietra, come la sta facendo e la farà anche in questo dibattito, perché è il riferimento

Sentivo come al solito un brusio di sottofondo, ma ormai abbiamo capito che è la colonna sonora della legislatura.

la forma repubblicana viene preservata, nessuno altera la forma repubblicana, nessuno sottrae poteri al Parlamento e nessuno sottrae poteri agli elettori; anzi, semmai c'è una responsabilizzazione degli elettori. Non viene alterata la forma parlamentare nella misura in cui non posso condividere l'argomentazione per la quale il Parlamento sarebbe sotto lo scacco e sotto la minaccia del Presidente eletto, che potrebbe minacciare di mandare a casa i parlamentari. Non sono questi gli argomenti per sostenere un'eventuale incostituzionalità, per la semplice ragione che esiste un principio di responsabilità degli eletti, nel momento in cui ci si siede in Parlamento. E questa responsabilità significa che tutte quelle prassi parlamentari che hanno portato nel tempo a mozioni di sfiducia per far cadere il Governo eletto sulla base dei voti degli elettori, per poi ricomporre nuove maggioranze, con questo sistema verranno meno o comunque saranno sicuramente ridotte e saranno molto più evidenti nella percezione degli elettori. Questo disegno di legge, a seguito degli emendamenti presentati dallo stesso Governo, che ha tenuto conto dei rilievi fatti dagli autorevoli costituzionalisti che sono stati auditi in Commissione, ha previsto espressamente che, a seguito della mozione di sfiducia, il Governo si scioglie e le Camere si sciolgono. Questa è la più evidente evidente garanzia che il potere appartiene al popolo. Non c'è quindi una violazione del principio di sovranità, una violazione della forma repubblicana perché, al contrario, proprio questa

che ho esposto Italia Viva-il Centro-Renew Europe si esprime in senso contrario alle pregiudiziali

Dobbiamo dirci chiaramente le cose. È da tempi antichi che la storia ci insegna che, per garantire la non degenerazione del potere,

un solo potere, quello esecutivo, mentre gli altri erano cancellati, hanno costruito una Costituzione sostanzialmente basata sulla centralità del Parlamento. Questa è la vera forza della Costituzione nata - come si usa dire - dall'antifascismo contro l'autoritarismo fascista. Questo è il dato fondamentale. Noi siamo di fronte al fatto che quei poteri vengono messi in discussione, con il con il rischio fondamentale di poter scivolare sul terreno di una concentrazione tutta architettata nelle mani di una sola persona, mettendo così in discussione i i reali poteri del Parlamento. Come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, in Paesi diversi dal nostro ci sono modalità ovviamente di elezione del Presidente della Repubblica

in sostanza i parlamentari sono eletti grazie al trascinamento dell'elezione del *Premier*, che saranno meno liberi di esprimere la propria opinione perché più ricattabili. È normale, è quello che succede. In ogni situazione, se un diritto viene dato da un altro, sei succube dell'altro. Il diritto deve essere un fatto indipendente ed è per questo che viene messo in discussione questo punto. Vogliamo sottolineare con forza l'eleggibilità e la libertà dei parlamentari. È questo che prevede la Costituzione. Noi dovremmo essere eletti in modo proporzionale. Tutte le posizioni dovrebbero essere rappresentate in questo Parlamento, ed è il dato che hanno fissato i Padri costituenti non a caso era fondato. La democrazia è un fatto di partecipazione: ci sono i partiti, ci sono delle associazioni e poi il popolo elegge i propri rappresentanti che esprimono il Governo. In questo caso si rovescia questo dato democratico ed è il *Premier* che elegge e trascina il Parlamento. Voglio sottolineare con forza questo dato. Il rischio della degenerazione, della concentrazione di un potere assoluto nelle mani di una sola persona è

Qual è il problema? Se non siete in grado di governare, è un problema vostro, ma non potete dire che c'è un problema di instabilità politica. Giustamente rivendicate il fatto che il vostro è un Governo politico e io sono d'accordo sui Governi politici, ma a quel punto assumetevi la responsabilità.

Bene, allora perché bisogna mettere in discussione il Parlamento? Qui ci va di mezzo prima di tutto il ruolo del Parlamento. Il rischio è sostanzialmente che i parlamentari stiano qui a dire sì o no alle decisioni che si prendono da un'altra parte.

voteremo contro questa proposta, proprio perché mette in discussione i princìpi fondamentali che stanno alla base della nostra Costituzione vorrei sottolineare - nata dalla lotta partigiana, dalla lotta antifascista, dalla battaglia per la libertà di questo Paese. E, quindi, cercheremo di impedire tutto quello che cerca di concentrare in una sola persona tutti i poteri dello Stato. *(Applausi)*.

fa parte del programma politico di Forza Italia, ma devo dire del centrodestra in tutte le sue accezioni. E credo che anche il presidente Berlusconi, a suo tempo, era partito con una proposta presidenzialista che caratterizzò fin dall'inizio il suo impegno politico. Nel tempo questo tema è emerso, è scomparso e oggi torna in una versione che è già una volontà di accordo più ampio con il Parlamento e con tutte le forze politiche. Le procedure di modifica della Costituzione impongono dei *quorum* e delle procedure qualificate; c'è comunque sempre la possibilità di un *referendum* confermativo, perché sappiamo che, quando si mette mano alla Costituzione, bisogna farlo con cautela, con senso di responsabilità, con spirito costruttivo. Ed è quello che noi stiamo facendo. Ieri, nell'intervento sul calendario dei lavori, ho fatto delle considerazioni che mi permetto di ribadire di fronte alle eccezioni di costituzionalità che sono venute. Non fa parte dell'aspetto delle eccezioni di costituzionalità, ma noi respingiamo la questione della tempistica, che molto anima le opposizioni. anima le opposizioni. Arriviamo a discutere questo disegno di legge nella prima delle quattro letture che la Costituzione prevede dopo un anno e mezzo di legislatura; faceva parte del programma della nostra coalizione, se ne discute da decenni - come ho avuto modo di ricordare più volte - e quindi nessuno può dire che c'è un colpo di mano, una accelerazione, una improvvisazione da parte nostra. Si è discusso a lungo in Commissione e voglio ringraziare il ministro Alberti Casellati. Quando si dice che non c'è stato ascolto, non si dice il vero: il testo è stato modificato; i nostri colleghi in Commissione, Ternullo e Occhiuto, hanno partecipato sempre con spirito costruttivo al dibattito e continueremo a farlo anche in Aula. Ieri ho citato delle osservazioni dell'onorevole Ceccanti, che poi le ha ascoltate, abbiamo avuto un rapido scambio e oggi ho visto i suoi ulteriori articoli di riflessione. Sulle proposte serie noi siamo aperti alla discussione. Il pregiudizio noi possiamo rispettarlo, ma non subirlo. Se uno è contro un meccanismo di democrazia diretta, ha diritto di esserlo, ma non ha il diritto di impedire agli altri di volere una democrazia più forte e più aperta al parere dei cittadini. Questa è la realtà dei fatti. Ci sono idee diverse, non è che noi non vogliamo rispettare il ruolo del Parlamento. Ora siamo in fase di esame delle questioni pregiudiziali Qualche settimana fa su «Il Foglio», che è un giornale a volte molto critico nei confronti della maggioranza, un giornale libero per definizione, il suo direttore con un articolo. A volte il giornalista riesce a sintetizzare meglio dell'accademico alcune questioni, perché deve svolgere un'azione divulgativa rivolta a chiunque, mentre l'accademico, il professore, ovviamente, a volte si rivolge a un circuito più esperto.

valutazioni che permettono di capire perché il premierato, pur non essendo la riforma più bella del mondo, può aiutare la Costituzione più bella del mondo a essere ancora più bella, più moderna, più efficiente,

di avere un Governo più stabile; una legge che consente a un Parlamento di avere coalizioni meno ballerine; una legge che sana un *virus* del sistema, ovvero la possibilità che vi siano Parlamenti governabili solo attraverso maggioranze artificiose ideate dal Capo dello Stato; una legge che preserva gran parte delle funzioni del Presidente della Repubblica: presiedere il Consiglio supremo di difesa, detenere il comando delle Forze Armate, presiedere il CSM, nominare un terzo dei componenti della Consulta, concedere la grazia, commutare le pene, eccezion fatta per la possibilità di sciogliere a propria discrezione le Camere. Cito Cerasa, perché tanto di professori e di accademici se ne citano tanti. A me sembra che questo sia un riassunto molto chiaro delle cose che si aggiungeranno. È ovvio la riforma sposta un po' il baricentro dalla parte del Governo, ma di un Governo eletto dai cittadini. La riforma non ha messo in Costituzione i numeri della legge elettorale, ma chiaramente prevede che ci possa essere un premio di maggioranza

primo in un Paese frammentato può avere il 51 per cento dei seggi. È evidente che numeri di congrua rappresentatività sono già scritti in sentenze della Corte e nella nostra piena consapevolezza

della scelta di sistema, con un premio di maggioranza che deve partire da una rappresentatività adeguata. Non si trasforma il 10 per Questo è molto chiaro nel testo che noi proponiamo. Leggo nelle questioni pregiudiziali alcune affermazioni apodittiche. Si parla di derivazione plebiscitaria del solo Presidente del Consiglio dei ministri.

non sono certo Paesi che possiamo accusare di mancanza di un impianto democratico solido e accettabile. Quindi, parlare di derive plebiscitarie,

ma noi, come abbiamo avuto già modo di dire, non stiamo ragionando con la fretta dei giorni. Signor Presidente, io non so nemmeno quale sarà la data di conclusione di questo dibattito. Superate le questioni pregiudiziali si aprirà un dibattito generale. Molti colleghi interverranno, anche il nostro Gruppo interverrà. Non abbiamo ragione di fare una serie di interventi ostruzionistici. Ci saranno interventi di merito di qualità che arricchiranno il dibattito, e concluderemo quando sarà il momento. Non vi è il problema di concludere prima o dopo le elezioni europee. Come abbiamo già avuto modo di dire, abbiamo trent'anni di ritardo perché, accanto alla Costituzione formale, che dobbiamo modificare con tutte le cautele e le attenzioni del caso, esiste una Costituzione materiale, termine che esiste anche in dottrina. Molte volte, le interpretazioni della Costituzione ne hanno modificato la portata in questo o in quel punto e spesso anche la Corte costituzionale interviene, non solo cassando leggi, ma con sentenze interpretative

L'esigenza di una *leadership*, di un mandato democratico e popolare, è avvertita da tempo. Dal 1994 ad oggi, le elezioni questo hanno rappresentato nella dialettica e nella sfida democratica di questo o di quel *leader*. Quindi siamo noi, come Parlamento, in ritardo su un tema,

gli argomenti della pregiudiziale. I tempi non erano maturi. L'Italia usciva da vent'anni di dittatura e capisco benissimo che, in quel momento, le decisioni non portavano verso questa realtà. Oggi, dopo decenni di democrazia consolidata, l'azione che il Governo e la maggioranza stanno svolgendo è legittima. Tutto quello che noi proponiamo è compatibile con i princìpi della prima parte della Costituzione. l'organizzazione della Repubblica potrà essere definita dal Parlamento e dal popolo. Se ci sarà un *referendum*, per noi sarà molto facile dire che, da un lato, c'è un sistema che dà più potere ai cittadini e, dall'altro, c'è chi vuole tenere nel palazzo

Cercherò di non entrare nel merito della riforma, perché avremo tempo durante l'ampia discussione generale di spiegare le motivazioni per cui riteniamo

È stato detto in modo molto chiaro che fa parte del programma di maggioranza e di Governo la riforma della Costituzione con l'elezione diretta di un Presidente

a quel mandato, quindi di conseguenza la riforma della Costituzione va nella direzione del mandato ricevuto. Non ho trovato in nessun passaggio, né dei singoli programmi elettorali delle forze di maggioranza di oggi, né nel programma di coalizione, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio che è fattispecie totalmente diversa dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Credo allora che forse questa maggioranza e questo Governo avrebbero dovuto avere più coraggio e proporre alle Assemblee parlamentari una una Repubblica presidenziale con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, perché, quello sì, sarebbe stato coerente con il mandato ricevuto dai loro elettori. Questo ragionamento introduce la prima eccezione di costituzionalità: dire che è indifferente eleggere in modo diretto il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio, perché è l'effetto rispetto al mandato elettorale quello di dare pieni poteri a un soggetto eletto dal Parlamento o eletto direttamente dai cittadini, mostra come i pesi e i contrappesi della Costituzione, che oggi sono garantiti attraverso le funzioni del Presidente della Repubblica, del potere esecutivo e del potere legislativo, con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio vengano totalmente stravolti, proprio in funzione del fatto che è la maggioranza a dire di voler dare poteri al Presidente eletto direttamente dal popolo, individuando i poteri del Presidente della Repubblica come naturali rispetto a quelli del Presidente del Consiglio. Quindi proprio nella manifesta volontà della maggioranza sta l'incostituzionalità della riforma. Entrando poi nel merito di altre questioni, può essere una riforma costituzionale oggetto di riflessione di costituzionalità? Ovviamente sì e cito la Corte costituzionale e la sentenza n. 1146 del 1988: «La Costituzione italiana contiene alcuni princìpi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali». Perché riteniamo che siano i princìpi contenuti nella Costituzione ad essere lesi e toccati da questa riforma? Perché è proprio il sistema di Stato repubblicano che si basa sui pesi e i contrappesi previsti nella Costituzione che viene intaccato da questa riforma costituzionale: non è vero che vengono fatti salvi o addirittura rafforzati i poteri del Presidente della Repubblica, perché il combinato disposto dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, del premio di maggioranza e del potere che si sposta quindi sulla parte dell'Esecutivo mette a repentaglio l'indipendenza del potere legislativo, ma soprattutto con una legge elettorale... Grazie, presidente Gian Marco. Dicevo che proprio il cuore di questa riforma, nel combinato disposto con la previsione del premio di maggioranza (che potrà determinare la vittoria elettorale di forze politiche che non saranno maggioranza nel Paese, se non maggioranza relativa molto limitata, ma che avranno un controllo totale dei numeri di Camera e Senato che saranno poi chiamati a eleggere il Presidente della Repubblica, i membri del Consiglio superiore della magistratura e i giudici della Corte costituzionale),

per cui la sfiducia al Presidente del Consiglio eletto porterà sostanzialmente, come conseguenza immediata, allo scioglimento delle Camere metterà il Presidente del Consiglio nelle condizioni di poter dire: io faccio quello che voglio, perché se non mi si dice fai quello che vuoi, faccio mandare a casa tutti. Questa è una stortura enorme rispetto ai pesi e contrappesi costituzionali. Ci sarà una sovrarappresentanza. La nostra Repubblica è fondata sulla sovranità che appartiene al popolo, che la esercita attraverso i dispositivi normativi. Il modo in cui i rappresentanti del popolo portano la sovranità popolare in queste Aule non è indifferente. È evidente che prevedere un premio di maggioranza in Costituzione e non nella legge elettorale porterà a una sovrarappresentazione di parti politiche che, peraltro, con l'astensionismo con cui siamo ormai abituati a confrontarci, farà sì che ci siano maggioranze che rappresentano una parte veramente minoritaria del Paese. poi la questione dell'elezione del Senato, prevista ovviamente su base regionale, che sarà soggetta a un premio nazionale di maggioranza. Voglio capire come si risolverà questa stortura costituzionale in un Senato che, in qualche modo, garantisce

una stortura sulla questione del voto degli italiani all'estero, che ha un elemento costituzionale forte e che non viene assolutamente risolta da nessun tipo di previsione all'interno della riforma. Ci sono milioni di cittadini italiani residenti all'estero, che hanno diritto di tribuna con elezione limitata di senatori e deputati, ma il cui voto avrà lo stesso peso di ciascun italiano residente in Italia. Su questo non vi è alcun tipo di risposta alle eccezioni che sono state fatte non soltanto delle forze politiche, ma anche da tutti i costituzionalisti che sono stati coinvolti nelle numerose audizioni

che oggi paghiamo rispetto ad altri Paesi, ma che domani pagheremo all'interno del nostro stesso Paese, con intere parti produttive che si sposteranno da una parte all'altra, a seconda di dove avranno maggior convenienza fiscale e di incentivo) e la riforma

Presidente, colleghi, saluto i rappresentanti del Governo, anche se sono in piedi e non al banco del Governo, sperando che possano lo stesso ascoltare quello che abbiamo da dire; anzi, chiederei al Presidente se può garantire che il Governo ascolti gli argomenti dell'opposizione, Per il Gruppo Partito Democratico questo disegno di legge a firma della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della ministra delle riforme Casellati, che saluto, è un provvedimento fortemente dannoso e negativo. Noi abbiamo presentato la questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del

sul metodo che la maggioranza e il Governo hanno seguito per portare avanti questo provvedimento e a considerazioni di merito. Cercherò di trattarle entrambe in questo intervento. Quelle di metodo, colleghi e rappresentanti del Governo, sono per noi questioni molto importanti. Noi svolgiamo questo dibattito sulle pregiudiziali in un giorno nel quale la Presidente del Consiglio parteciperà alla Camera dei deputati ad un convegno intitolato «La Costituzione di tutti». Io trovo che ci sia dell'ipocrisia dell'ipocrisia e anche della mendacità - lo dico alla ministra Casellati in modo che possa riferirlo alla Presidente del Consiglio - nel partecipare a un convegno che si intitola «La Costituzione di tutti», quando ogni giorno abbiamo la prova che, per la Presidente del Consiglio e per questo Governo, la riforma costituzionale è un affare di parte e la Costituzione non è di tutti, ma è una cosa che si intende cambiare e cambiare male da soli. che sia imbarazzante partecipare a convegni con questo titolo; o non vi si partecipa o si chiede che abbiano un altro titolo. Non c'è stata alcuna apertura reale al dialogo in questa operazione di riforma della Costituzione che il centrodestra sta portando avanti. Voglio dirlo al senatore Gasparri, che in una parte importante del suo intervento ha detto che abbiamo ascoltato. Forse, senatore Gasparri, avete ascoltato, ma di sicuro vi siete comportati come se, anche ascoltando, non aveste sentito nulla. Questo è quello che è avvenuto nel dibattito che abbiamo svolto fin qui, perché ai nostri argomenti, alle nostre proposte avete opposto una chiusura ermetica, pregiudiziale, che credo sia stata una scelta molto sbagliata. Qualcuno dirà che l'opposizione ha sbagliato e ha dimostrato un atteggiamento pregiudiziale perché ha presentato, sia in Commissione, sia in Aula, tantissimi emendamenti. Attenzione, anche qui - lo voglio dire all'opinione pubblica - c'è una fregatura: noi non abbiamo presentato tanti emendamenti perché non vogliamo il dialogo; noi abbiamo presentato tanti emendamenti esattamente perché ci è stato impedito di dialogare ed è una forma di difesa, non di attacco. Non accetteremo rovesciamenti della realtà rispetto a questa nostra decisione. Altre cose che nel metodo ci lasciano estremamente perplessi hanno a che vedere con la logica del baratto che ispira questa riforma. che c'è nella maggioranza uno scambio, un baratto appunto, tra il premierato, l'autonomia differenziata e la separazione delle carriere, come se la Costituzione si potesse fare a pezzettini e si potesse regalare un pezzettino di Costituzione a ciascuna delle anime di questa maggioranza. Sì, lo si può fare, ma è un tentativo molto pericoloso che denunciamo come tale e che è del tutto incompatibile con lo spirito della Costituzione di tutti. Questa è la Costituzione dei bassi scambi, non la Costituzione di tutti. che c'è, da parte soprattutto di una componente della maggioranza che rappresenta una cultura politica che fu esclusa dal patto costituzionale del 1946-1947, il tentativo di mettere le mani pesantemente sulla Costituzione per cercare una nuova legittimazione, per lasciare la propria firma su un cambiamento radicale e stravolgente della forma di governo. Ma lo spirito di rivincita e di rivalsa non va bene quando si parla di Costituzione, e anche questo tentativo credo che debba essere criticato. Passiamo alle fortissime perplessità di merito che abbiamo; nell'esaminarle mi aiuta molto l'intervento organico, benché da me non condiviso, che ha fatto il senatore Gasparri. Il senatore Gasparri, discutendo della pregiudiziale, ha messo in fila tutti gli slogan che sentiremo per un anno e mezzo a difesa di questa riforma. L'ha fatto in maniera ordinata propinandoci tutti i cavalli di battaglia che saranno oggetto di una martellante campagna di comunicazione. Ci ha detto che con questa riforma la nostra democrazia sarà più forte: questa è una bugia, la forza di una democrazia dipende dall'equilibrio che c'è tra i poteri che della democrazia sono il pilastro, dipende da quanto è forte il pluralismo, da quanto sono forti le garanzie e gli organismi di garanzia. democrazia con questa riforma diventa più debole e più povera, altro che una democrazia più forte; avviene esattamente il contrario. Il senatore Gasparri ci ha detto, sempre con tono molto solenne:

è estremamente sgradevole ed è spia di un atteggiamento antiparlamentare *(Applausi)* che trovo da condannare e che tutti dovremmo condannare. Non c'è niente di rispettabile nel dipingere queste Aule come palazzo, in maniera spregiativa. Noi, anche alle scuole che salutiamo sempre alzandoci in piedi nell'Aula del Senato quando vengono a visitarci, diamo un segnale pessimo se per primi definiamo

dare più potere ai cittadini, avreste preso un impegno solenne e presentato un disegno di legge per restituire ai cittadini il potere di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento *(Applausi)*, che è un Noi sappiamo che per voi le liste bloccate e l'esclusione dei cittadini dalla selezione dei parlamentari sono un dogma e non ci rinuncerete mai, perché le liste bloccate sono funzionali alla vostra concezione del Parlamento, che non vedete come un potere che equilibra quello esecutivo, ma come un ammasso di soldatini che deve dire signorsì al Presidente del Consiglio: questa è la concezione del Parlamento che voi portate avanti *(Applausi)* e che è evidente nella vostra riforma. Se non si dà ai cittadini il potere di eleggere i parlamentari in maniera che il loro voto sia incisivo, se si cancella l'autonomia del Parlamento con l'elezione a strascico di una carica monocratica, non si dà più potere ai cittadini:

altro argomento - che non si toccano i poteri del Presidente della Repubblica. A me questa idea che ripetere una menzogna

non viene indebolito da questa riforma, ma l'effetto di questa riforma è esattamente quello di indebolire e svuotare le prerogative del Presidente della Repubblica, che non ha più una legittimazione pari a quella del Presidente del Consiglio, che ha poteri di nomina del Presidente del Consiglio e di scioglimento fortemente lesionati dalle disposizioni che del provvedimento fanno parte, che viene sostanzialmente messo alle corde e che non ha più la possibilità, per questo motivo, di svolgere quella funzione di motore di riserva e di coordinamento dei poteri costituzionali che si è rivelata preziosissima in questi decenni. E poi pensate quanto è davvero buffo

Infine, ci ha detto sempre il senatore Gasparri - mi scuserà se lo cito in continuazione, ma il suo intervento ha fornito la traccia per il mio - «noi vogliamo Governi più stabili». Ma, insomma, non prendiamoci in giro. L'Europa è piena di Governi stabili: la Germania, la Spagna, la Svezia. E l'Europa dimostra che si possono avere Governi più stabili e più efficienti rimanendo nella forma di governo parlamentare, senza liquidare la centralità e l'autonomia del Parlamento e soprattutto senza fare l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che - voglio ricordarvelo - non è presente in nessun Paese del mondo. In tanti Paesi del mondo ci sono Governi stabili, ma in nessun Paese del mondo c'è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Questo vostro argomento vi si sgonfia in mano, non ha alcuna validità. Avreste dovuto prestare più attenzione alle nostre proposte, ispirate al modello tedesco, perché noi crediamo che delle riforme servano, ma che si debba rafforzare e razionalizzare la forma di governo parlamentare, non pensiamo che la forma di governo parlamentare vada buttata via e liquidata. questa è una forma di governo parlamentare, come ci è stato ripetuto più volte, e che anzi è una forma di governo neoparlamentare, ci è stato spiegato, perché il Parlamento conserva il potere di sfiduciare il Governo. Sì, è vero, conserva il potere di sfiduciare il Governo, ma nella riforma sta scritto che, se approva una mozione di sfiducia, il Parlamento si estingue. Ora, che potere è un potere che, se lo eserciti, determina la tua morte? È un potere...

ci è stato detto che questo disegno di legge è un passo verso le opposizioni, perché voi volevate il presidenzialismo, le opposizioni non lo volevano e quindi ci siete venuti incontro facendo il premierato. No, è falso. Lo squilibrio tra i poteri che c'è in questa proposta di legge e soprattutto l'umiliazione del Parlamento e del Presidente della Repubblica disegnano uno squilibrio complessivo dei poteri che è molto peggio di quello che c'è nei sistemi presidenziali. *(Applausi)*. Non ci siete venuti incontro; vi siete ulteriormente allontanati dalla strada della ragionevolezza e dalla strada che ha indicato l'opposizione. Chiudo dicendo questo: ieri il senatore Malan ci ha accusato di svolgere un'opposizione cieca e inefficace. Lo voglio rassicurare: ci vediamo bene e abbiamo elencato bene tutti i limiti di questo provvedimento. Siamo determinati a svolgere un'opposizione molto efficace e il senatore Malan potrà rendersi conto della determinazione con cui contro questo provvedimento. Infine, non so se c'è la senatrice Musolino, ma lo dico al Gruppo che la senatrice Musolino rappresenta. L'articolo 93 del Regolamento del Senato non dice che le questioni pregiudiziali vanno approvate solo se si ritiene che un provvedimento sia incostituzionale. Invito a leggere l'articolo 93 del Regolamento, il quale dice che la questione pregiudiziale è la proposta di non passare alla discussione di un provvedimento, per ragioni che possono essere costituzionali o meno. Ho letto che il *leader* del Gruppo Italia Viva ha definito questa riforma con un giudizio preciso una tale schifezza da...

Signor Presidente, discutiamo di una questione pregiudiziale che è stata motivata.

vuole fare una riforma costituzionale e che tale riforma potrebbe essere incostituzionale è già complesso di per sé. Questo esercizio diventa ancora più complesso e difficile leggendo quello che è stato scritto nelle questioni pregiudiziali.

quali sarebbero i principi fondamentali e supremi che questa riforma costituzionale lede. Anche perché, l'articolo 1 della Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo. Ritenere incostituzionale concedere ai cittadini la possibilità di scegliere il proprio Presidente del Consiglio è un esercizio abbastanza ardimentoso. abbastanza ardimentoso quanto quello che è stato fatto da qualche collega che mi ha preceduto che ha addirittura parlato e ci ha accusato di voler mantenere le liste bloccate. La stessa sinistra che ha votato

volete che i parlamentari siano eletti a preferenza, ma che il Presidente del Consiglio non sia scelto dagli italiani. *(Applausi)*. Nelle argomentazioni ci deve essere quantomeno una coerenza di base. Una coerenza che non c'è stata nel corso di tutta la discussione perché si è oscillato in maniera caotica e in maniera del tutto irrazionale tra una legge costituzionale che, ad avviso di alcune delle opposizioni, non risolve alcun problema, e una legge costituzionale che prevede ed è premonitrice di un sistema non più parlamentare, non più repubblicano, ma di un autoritarismo che potrebbe dilagare nel Paese.

La verità - ed è questo uno dei motivi per i quali non c'è alcun vizio di costituzionalità in questa legge costituzionale - è che questa legge non altera in alcuna misura gli equilibri dello Stato. Non altera e non modifica in alcuna misura i poteri del Presidente della Repubblica. Non altera e non inficia in alcuna misura i poteri che avrà il Parlamento, che manterrà la possibilità di sfiduciare, come è avvenuto sino a oggi, il Presidente del Consiglio e avrà la possibilità di sfiduciare anche, eventualmente, il Governo, qualora alcuni provvedimenti non gli piacciano. Lo dico perché si continua volutamente a intorbidire e a confondere le acque sul tema del Presidente della Repubblica, pensando che probabilmente i cittadini non lo capiscano, avendo sempre il retropensiero che i cittadini non abbiano abbastanza strumenti per capire tali questioni,

l'instabilità, dal 1946, ha prodotto 67 Governi che hanno avuto la durata media di 414 giorni. A fronte del problema dell'instabilità, del problema della difficoltà del Parlamento di esprimere dei Governi stabili, delle vicissitudini parlamentari, si è avuta, soprattutto negli ultimi decenni, un'espansione

Aula, i Presidenti della Repubblica hanno molti meno poteri del Presidente della Repubblica italiano *(Applausi)*, poteri che noi vogliamo mantenere, poteri che sono giusti, che sono indispensabili all'esercizio della democrazia e che nessuno si sogna minimamente di togliere. Certo è che di fronte a meccanismi e a difficoltà parlamentari, se possiamo togliere qualche problema al Presidente della Repubblica, che appunto nel corso degli ultimi decenni ha dovuto espandere le proprie attività per risolvere i problemi che il Parlamento non è riuscito ad affrontare, lo facciamo. È per questo che il tema principale è l'instabilità il tema principale è l'instabilità dei Governi ed è l'obiettivo fondamentale di questa riforma, comunque nel contesto e nel mantenimento dei princìpi repubblicani, che restano completamente inalterati, tanto che stiamo parlando di una riforma neo-parlamentarista, non neo-autoritaria. Stiamo parlando di una riforma che è esattamente nel solco dei principi fondamentali della Costituzione.

di una riforma che invece vuole restituire o dare maggiore pienezza a quella sovranità che appartiene al popolo, che l'articolo 1 della Costituzione richiama. tanti, i pregiudizi: il pregiudizio che i parlamentari non siano abbastanza liberi da poter scegliere se votare o non votare la fiducia, rappresentati come incollati alle poltrone, col terrore di rimanere senza stipendio, e che quindi non sarebbero liberi, nel caso in cui il *Premier* poi esercitasse il potere di scioglimento, di decidere autonomamente se dare o non dare la fiducia. È questo il rispetto del Parlamento e del ruolo che tanto viene decantato dalle opposizioni? Oppure il pregiudizio che la stabilità debba trasformarsi automaticamente in autoritarismo; oppure il pregiudizio che soltanto voi possiate toccare la Costituzione e anche qui, forse è meglio avere un po' di memoria storica, perché non ricordo che le precedenti riforme costituzionali, che dall'altra parte avete votato, le abbiate fatte in condivisione con l'opposizione. *(Applausi)*. Non ricordo che quella riforma, l'ultima riforma costituzionale del Governo Renzi, sia stata votata da un solo partito dell'opposizione.

una propria legge elettorale e una propria riforma costituzionale, ma sia costretto, come hanno chiesto alcune delle opposizioni in Commissione, ad andare a scopiazzare le le riforme costituzionali della Francia, della Germania o di altri Paesi. Uno dei principali pregiudizi che avete avuto è quello di dire che noi siamo gli unici che avremo questa

noi viviamo e vivremo sempre di fede e di fiducia nei confronti dei cittadini italiani; la stessa fede e la stessa fiducia che ci hanno portato a restituire loro la volontà popolare e la possibilità di scegliere il proprio Presidente del Consiglio.

della manifestazione per la festa della mamma, che è oggi e che desidero celebrare augurando una felice giornata a tutte le mamme del mondo.

l'idea dalla quale parte questa riforma è che la democrazia rappresentativa, che ha svolto una funzione decisiva nei primi decenni del Dopoguerra, debba essere oramai sostituita dalla democrazia decidente: il passaggio quindi da democrazia pluralista a una democrazia identitaria, il tutto senza preoccuparsi dei necessari contrappesi. La giustificazione fornita dalla stessa relazione al disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa n. è definita dall'esigenza di operare un intervento minimale: si rafforza il Governo, così viene scritto, al fine di risolvere il grave problema dell'instabilità politica. Questo assunto è del tutto scorretto, signor Presidente, almeno a nostro modo di vedere, per tutta una serie di ragioni. La prima è tecnica ed è stata sollevata dalla grandissima parte degli auditi: questa riforma era scritta male nel testo iniziale, anche per questo è stata ampiamente modificata dagli emendamenti governativi, ma ancora adesso, nel testo approvato dalla Commissione affari costituzionali, problemi interpretativi complessi e irrisolti, alcuni del tutto nuovi, sui quali non si è fatta la dovuta riflessione. Come possiamo oggi approvare un testo, sapendo già che è ambiguo e darà luogo a difficoltà interpretative? Il secondo rilievo è di merito e riguarda proprio la scelta di fondo del cosiddetto premierato. La riforma interviene sottraendo potere al Parlamento e al Capo dello Stato per assegnarlo al Presidente del Consiglio. L'accentramento dei poteri in una sola persona, il Primo Ministro, senza prevedere adeguati nuovi e importanti contrappesi, è un errore che rischia di dimostrarsi irreparabile, che pone in pericolo la tenuta democratica del Paese e che noi non possiamo permetterci. C'è dell'altro, però, signor Presidente. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio costituirebbe un caso unico nel moderno costituzionalismo democratico, che certo prevede regimi presidenziali e semipresidenziali, ma disciplinati in modo diverso, con l'istituzione di robusti contrappesi, che invece in questo caso vengono completamente depotenziati, dove addirittura non eliminati del tutto. Il rischio è chiaro, o almeno lo è per noi: il grande pericolo che la storia di questo Paese dovrebbe averci insegnato è quello di accentrare in un solo esponente politico, in una sola persona, per un lungo periodo, un'enorme concentrazione di poteri come quella tipica del vertice del Governo nei settori delle relazioni internazionali, della sicurezza e della difesa, dell'economia e della moneta, dell'ordinamento delle istituzioni amministrative e giudiziarie e del sistema delle autonomie territoriali, per di più contemporaneamente riducendo - dove non annullando del tutto, addirittura - i normali poteri del Presidente della Repubblica e del Parlamento. Ed è pacifico che questo avvenga, che i poteri del Presidente della Repubblica con questa riforma vengano fortemente ridotti. Egli infatti non perderebbe solo il potere di nomina dei senatori a vita e di scelta di un Presidente del Consiglio estraneo ai parlamentari, ma non potrebbe più sciogliere, in modo anticipato, una Camera. Soprattutto, vedrebbe disciplinato in termini molto restrittivi il potere di nomina del Presidente del Consiglio e quello di scioglimento delle Camere, ormai del tutto vincolato. Potrei continuare, signora Presidente, con i numerosissimi dubbi sollevati dai costituzionalisti intervenuti in Commissione, dubbi su nomina e poteri dei Ministri, fiducia, sfiducia, legge elettorale e, Presidente, chi più ne ha più ne metta. Vorrei chiudere con una considerazione: con grande enfasi si è sostenuto che sarà il popolo a scegliere il *premier* e che con la riforma verrà restituito il potere di scelta al corpo elettorale, ma non è vero. Quello che vorrei sottolineare è che, invece, ad essere spogliato del potere sarà proprio l'elettore: ad essere ridotti in modo radicale sono infatti i poteri del corpo elettorale, chiamato a fare una sola scelta tramite un'unica votazione di tipo maggioritario, ogni cinque anni, sulle proposte comunque avanzate dai vertici del sistema politico. L'elettore, dunque, indicherà un nome e poi per cinque anni più nulla. In conclusione, Presidente, vorrei unirmi a chi prima di me questa mattina ha evidenziato che con questa riforma si stravolge il centro del nostro sistema di governo e lo si fa in modo maldestro e approssimativo, senza tenere nella dovuta considerazione i rischi connessi alla concentrazione di tutto il potere nelle mani di una sola persona. Ad essere del tutto assenti - lo abbiamo già detto - sono i contrappesi indispensabili per bilanciare lo strapotere assegnato al Presidente del Consiglio e ad essere depotenziati in modo insostenibile Parlamento e Presidente della Repubblica. Siamo contrari a questa riforma perché è scritta male, ma anche e soprattutto perché non condividiamo l'idea di fondo che la sostiene. Per questo motivo, Presidente, la contrasteremo

onorevoli colleghi, ministro Casellati, credo che la forte opposizione a questa riforma che ci accingiamo a fare e che la ministra Alberti Casellati ha giustamente definito la madre di tutte le riforme, derivi dal fatto che la stessa sarà un successo storico, direi epocale per il Governo, se riuscirà a portarlo a compimento. Io interpreto l'atteggiamento dell'opposizione come una forma di rivalità politica, non voglio dire di invidia politica, più una competizione naturale tra partiti che aspirano a lasciare un'impronta duratura nella storia del Paese attraverso riforme significative. Rispondendo a chi sostiene che la Costituzione non debba essere modificata, credo sia essenziale riconoscere che le Costituzioni debbano evolvere per rimanere al passo con i cambiamenti sociali, tecnologici ed economici. Una Costituzione statica potrebbe non riuscire a proteggere, infatti, efficacemente i diritti e a soddisfare le esigenze di una società in rapida evoluzione. Aggiornare la Costituzione può essere necessario per affrontare nuove sfide, come la digitalizzazione, le diversità crescenti e le crisi globali, come i cambiamenti climatici e le pandemie. Modificare la Costituzione non significa stravolgerne i princìpi, però, ma piuttosto aggiornarla per rispecchiare e gestire la realtà del mondo contemporaneo, assicurando che rimanga uno strumento vivente al servizio della giustizia e della democrazia. Non è certo un capriccio del momento, come ha sostenuto qualcuno, ma un necessario adattamento di fronte ai cambiamenti in atto nella società e ad una cronica instabilità governativa che ha visto in Italia alternarsi Governi cosiddetti tecnici e giochi di Palazzo troppo frequentemente. È una riforma coraggiosa, dal punto di vista della maggioranza, che non ha paura di mettersi in discussione anche ricorrendo, se è il caso, a una consultazione popolare; un passo avanti verso un sistema più stabile e rappresentativo, un sistema in cui ogni voto possa contare realmente verso la formazione di un Governo solido e duraturo. Desidero chiarire alcuni punti fondamentali, contrastando talune affermazioni emerse recentemente in quest'Aula. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni (il presidente Boccia, per esempio), il nostro impegno in Commissione non è stato silente. Io, la collega Ternullo e gli altri colleghi della maggioranza, diciamo la verità, abbiamo fatto il contrario. Abbiamo affrontato con serietà e dedizione, grazie anche al presidente Balboni che ha diretto molto bene la Commissione, l'esame di migliaia di emendamenti, molti dei quali tendenti all'ostruzionismo, ripetitivi e non costruttivi. Abbiamo ascoltato un po' di tutto: teorie interessanti, ma poco attinenti al tema in discussione; richiami frequenti all'idea di voler creare l'uomo forte al potere, con l'accostamento a personaggi come Hitler e ad altri dittatori. È essenziale a questo riguardo ricordare che i regimi autoritari sorti in Europa nel ventesimo secolo non sono emersi a causa di riforme democratiche come quella proposta oggi, ma attraverso l'abolizione di strutture democratiche esistenti e approfittando di crisi profonde e di disperazione sociale. Nonostante questa opposizione strumentale, a volte però sono state accolte e integrate nel testo quelle proposte costruttive che hanno arricchito la riforma, con la dimostrazione concreta che da parte del Governo e della maggioranza c'è stata e c'è ancora una reale apertura al dialogo costruttivo. Mettendo da parte le divergenze è stato possibile lavorare su aspetti cruciali come il limite dei mandati o la struttura del voto di fiducia. Il Governo ha risposto con attenzione alle proposte di modifica quando si è trattato di questioni tecniche complesse, come il premio di maggioranza, ha mostrato anche grande disponibilità. Questo atteggiamento costruttivo, grazie alla costante presenza della ministra Alberti Casellati, al suo incessante lavoro - per questo la ringrazio

e che è disposta a perfezionare la sua azione legislativa in risposta alle esigenze che emergono anche dall'opposizione. Semmai, l'atteggiamento di chiusura è stato quello dell'opposizione. Sul principio dell'elezione diretta si è scelto devo dire in questo caso legittimamente, ma è stata una scelta - di non voler neppure dialogare, seppure il Governo avesse voluto dare inizialmente un'apertura anche su questo punto, decidendo di mettere sul tavolo della discussione l'elezione del *Premier* anziché, come inizialmente previsto, quella del Presidente della Repubblica. L'affermazione che la sovranità popolare non possa essere concepita con l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio riflette una comprensione limitata, secondo me, sia del principio stesso di sovranità popolare sia delle dinamiche democratiche contemporanee. Per prima cosa, la sovranità popolare è un principio fondamentale delle democrazie moderne che prevede che il potere dello Stato derivi dalla volontà del popolo. La modifica prevista al sistema di Governo, che introduce appunto l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, non solo non erode questo principio, ma anzi lo rafforza offrendo ai cittadini un ruolo più attivo e diretto nella scelta del loro *leader*. In secondo luogo, la critica secondo cui l'elezione diretta del Presidente del Consiglio concentrerebbe eccessivo potere nelle mani di un singolo individuo trascura il contesto più ampio del sistema politico italiano, caratterizzato da meccanismi di controllo e di bilanciamento tra i vari organi dello Stato, che garantiscono il mantenimento di un equilibrio efficace tra i poteri. Per terza cosa, l'elezione diretta è una pratica già adottata nella sostanza in diverse democrazie mature, dove non ha pregiudicato la sovranità popolare, ma ha spesso contribuito a una maggiore stabilità governativa e a un rafforzamento della legittimità democratica dei *leader* eletti. La scelta di puntare sull'elezione del Presidente del Consiglio e non sul Capo dello Stato riflette non solo la volontà di aprire al confronto con le forze dell'opposizione, ma anche al criterio di creare un sistema ancora più democratico di altri Paesi e anche di garanzia. Il Presidente del Consiglio italiano nella riforma sarà eletto direttamente, ma non avrà anche, come succede per esempio in America, la funzione di Capo dello Stato, mantenendo un ruolo più limitato rispetto agli omologhi americani e anche a quello francese; rimarrà inoltre dipendente dalla fiducia del Parlamento. In Italia la proposta conserva un equilibrio di poteri, confermando il ruolo del Presidente della Repubblica come garante istituzionale, che rimane fondamentale; non è come dicono dall'opposizione. Non subisce poi limitazioni rispetto alla sua funzione più importante, che è quella appunto di garante delle istituzioni. I suoi poteri non sono minimamente diminuiti da questa riforma. Al contrario, il Presidente della Repubblica mantiene cruciali prerogative come il comando delle Forze armate e la nomina dei giudici della Corte costituzionale. Contrariamente alle critiche emerse dall'opposizione, non si tratta quindi di un depotenziamento, ma di un'adeguata separazione dei poteri, che mira a una maggiore efficienza e responsabilità dell'Esecutivo. Questi poteri assicurano che il Presidente continui a esercitare un ruolo di equilibrio nel nostro sistema politico e anche il Parlamento, dopo l'adozione della riforma Casellati, manterrà un ruolo centrale e influente nel sistema politico italiano: non solo rimarrà l'organo primario per la formulazione e l'approvazione delle leggi, garantendo che l'agenda del Governo rifletta il consenso parlamentare, ma il Presidente del Consiglio dovrà ottenere e mantenere la fiducia. Il Parlamento continuerà inoltre ad esercitare il controllo sul Governo attraverso interrogazioni, Commissioni d'inchiesta e altre forme di supervisione. Questa struttura assicura il sistema politico italiano continuerà a offrire un robusto sistema di controllo e di bilanciamento, fondamentale per prevenire l'accentramento autoritario del potere. Il Presidente degli Stati Uniti, per esempio, è capo dello Stato e del Governo, con ampi poteri esecutivi, incluso il veto sulle leggi e la nomina dei giudici della Corte suprema. Il Presidente della Francia unisce il ruolo di capo dello Stato a quello di figura chiave nel Governo, guida la politica estera e ha il comando delle Forze armate. La proposta di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio risponde all'esigenza di maggiore stabilità e rappresentatività, riflettendo anche l'evoluzione democratica di altre Nazioni. Stabilità governativa che non solo rafforzerà il sistema politico, migliorandone l'efficacia, ma potrebbe anche, come ha detto giustamente la ministra Alberti Casellati, anzi lo farà certamente, stimolare la crescita economica e promuovere una società più coesa e prospera. Concludo ribadendo il nostro pieno sostegno a questa riforma costituzionale, essenziale per garantire stabilità, efficacia e responsabilità del nostro Governo. È un cambiamento necessario, che rispetta la nostra storia, un ritorno a princìpi che sono fondamentalmente e profondamente italiani: l'elezione diretta è radicata nella tradizione politica dalla Roma repubblicana e delle città-stato del Rinascimento, con l'idea che il popolo debba avere un ruolo centrale e attivo nella scelta dei governanti. È un cambiamento necessario, perché prepara il terreno per un futuro in cui la volontà popolare trova la sua più piena espressione. Questa riforma è una risposta diretta ed essenziale alle esigenze dei nostri tempi, ma anche e soprattutto un invito a rafforzare la nostra democrazia, non ad indebolirla. Ecco perché merita il nostro sostegno. *(Applausi)*. docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Alfano da Termoli» di Termoli, in provincia di Campobasso,

avevano un obiettivo ben chiaro, quello di proteggere la democrazia e l'Italia da possibili distorsioni del principio democratico, da possibili derive autoritarie. Avevano la piena consapevolezza dei disastri che erano stati appena compiuti dalla dittatura fascista, dalla scellerata alleanza con i nazisti delle deportazioni e delle camere a gas; avevano capito quale fosse il pericolo della eccessiva concentrazione del potere in una sola persona. Fu per questo che decisero di inserire degli equilibri democratici, che funzionavano con la precisione di un orologio. La democrazia, lo Stato di diritto erano difesi da una netta divisione dei poteri e dalla presenza di figure di garanzia, come il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Sono proprio questi equilibri che hanno garantito la democrazia, lo Stato di diritto e la libertà dei cittadini. Ora, colleghi, questa riforma sul premierato sta distruggendo questi equilibri, questa riforma sta spostando l'ago della bilancia democratica soltanto verso uno dei poteri dello Stato, anzi verso una sola persona dello Stato. Con la pretesa di un rafforzamento dell'Esecutivo voi state smantellando quella che era una Costituzione democratica antifascista, una Costituzione che avrebbe impedito qualsiasi tipo di distorsione del principio Ora se è questo che veramente volete, potete farlo. Però, vedete, voi avete il dovere di essere onesti nei confronti dei cittadini, di dire chiaramente quello che state facendo, perché a sentire i vostri *slogan* sembrerebbe quasi che si tratti soltanto di una questione di elezione diretta del *Premier* e allora i cittadini immaginano - perché questo voi dite - che si tratti della stessa persona che sono abituati ad avere oggi.

Presidente, bisogna che la gente questo lo sappia, non è più il *Premier* che siamo abituati a conoscere. Voi state inserendo la figura di un *Premier* che avrà dei poteri enormi,

E invece noi no, noi vogliamo un *Premier*, che si sveglia da un giorno all'altro e può decidere di dimettersi e mandare tutti alle elezioni; può deciderlo da solo e il Presidente della Repubblica, che doveva essere una figura di garanzia, non potrà dire nulla. Vi ricordate la formulazione dell'emendamento del Governo che diceva che il *Premier* può proporre al Presidente lo scioglimento delle Camere? Peccato però che dopo questo Presidente non poteva avere il potere di rifiutare. Era una proposta che non poteva rifiutare.

non per motivi politici, ma perché magari ci accorgiamo che questo Presidente del Consiglio è legato alla malavita, alla criminalità organizzata oppure che è finito in uno scandalo internazionale di corruzione internazionale di corruzione ed è inadeguato a coprire il suo ruolo, per farlo dovrà andare a casa, si dovrà suicidare. Non avete previsto correttivi perché alle dimissioni sono associati i poteri di chiedere e ottenere lo scioglimento delle Camere. Questo, Presidente e colleghi, non succede in nessuna delle democrazie occidentali. Prima il collega Lisei si chiedeva perché dobbiamo copiare gli Stati Uniti o la Francia. Dovete copiare da loro perché non sapete farlo. *(Applausi)*. La democrazia deve sempre garantire la separazione dei poteri. Gli Stati Uniti sono una grande democrazia, ma i poteri sono separati. Il Presidente americano non può sciogliere il Parlamento, ma può finire lui sotto *impeachment* se commette dei gravi crimini.

in Costituzione. La Costituzione contiene i valori fondanti. I valori costituzionali sono quelli in cui la nostra società crede. Il premio di maggioranza, però, colleghi, è questione di legge elettorale, è un correttivo. Significa che voi avete dato costituzionalità dato costituzionalità al principio secondo cui la maggioranza è fittizia. Capite che non può essere un principio costituzionale? Se proprio lo volete inserire lì, in mezzo ad altri valori del nostro Paese, volete dire almeno come e quando questo premio viene assegnato o lo lasciamo così, senza neppure indicare una percentuale minima per poterlo avere? Il Il premio di maggioranza risponde ad esigenze contingenti e non si può mettere senza indicare anche alcuni paletti. Guardate che c'è un precedente storico in cui il primo partito, senza bisogno di alleanze, poteva garantirsi la maggioranza dei seggi in Parlamento; la legge Acerbo che consentì a Mussolini di avere una solida maggioranza in Parlamento. Ora capite che, se inserite il premio di maggioranza, dovete anche dire come, quando e quali sono i limiti minimi e noi dobbiamo fidarci che forse correggerete questo errore con una legge elettorale. Ma francamente mi fido poco di un Governo che nella prima stesura, addirittura, aveva fissato un premio di maggioranza al 55 per cento per la forza politica più grande: sarebbe bastato un 25 per cento per avere il 55 per cento Aspettiamo con fiducia che questo errore sia corretto quantomeno nella legge elettorale. Parliamo anche della stabilità, adesso, perché mi pare che tutta la motivazione a fronte di quella che considerate la madre di tutte le riforme sia la stabilità. Come volete garantire la stabilità? Ci state dicendo che porrete un limite al Parlamento nel votare la sfiducia. Benissimo. Quindi, la stabilità poggerà sul fatto che voi credete che i parlamentari, piuttosto che mandare via un *Premier* incapace, corrotto o che fa parte della malavita organizzata, faranno una scelta non di merito,

a cosa serve la stabilità. La stabilità, colleghi, serve perché le imprese e gli investitori hanno bisogno di regole certe; hanno bisogno di evitare che si cambino le regole del gioco strada facendo. parte di un Governo che è riuscito a bloccare i cantieri in tutte le città d'Italia, comprese le zone terremotate del Centro Italia, perché avete cambiato le regole anche a quelli che stavano lavorando sul superbonus? La stabilità che vogliono le aziende è la certezza che le leggi non cambino e che, quando si insedia un Governo, non vada a smantellare tutto quello che hanno fatto i Governi precedenti. E poi, se ci tenete davvero alle imprese, vi siete resi conto che le imprese per investire in Italia vogliono anche un contesto di legalità? Guardate le vostre politiche sulla giustizia: cancellate il reato dell'abuso d'ufficio; spuntate le armi alla procura; rendete più difficili le intercettazioni. E questo secondo voi favorisce il clima di legalità che favorisce, a sua volta, gli investimenti nel nostro Paese? Quella che state seguendo - badate bene - è una linea politica che condurrà l'Italia sul baratro, che la condurrà nella direzione opposta a quella verso cui voi state promettendo di volerla indirizzare.

Colleghi, state commettendo un grave errore, perché state facendo il contrario di ciò che la ragione ci indurrebbe a fare. State cedendo al fascino dell'uomo forte, un fascino nostalgico verso un padre che ci comanda. noi italiani siamo un popolo di maggiorenni e non abbiamo bisogno di chi ci comanda. Dobbiamo poter ancora credere che ci si può difendere, che possiamo insieme risolvere i problemi, che ci possiamo difendere insieme dalle paure, che non abbiamo bisogno di eroi. Noi Noi non potremo sapere se il super *Premier* sarà di destra o di sinistra, ma possiamo essere sicuri di una cosa, ovvero che non c'è peggior potere di quello che si nasconde dietro una sola facciata di democrazia.

per più di quattro mesi le sedute della Commissione affari costituzionali, molte delle quali anche serali, non hanno trattato altro che la riforma costituzionale del premierato. Eppure, dobbiamo constatare che un vero confronto politico di merito non si è purtroppo mai avviato, perché il Governo, signora Ministra, e la maggioranza che lo sostiene non lo hanno mai voluto avviare. Abbiamo proposto di iniziare con il condividere un'analisi dei principali problemi della nostra democrazia, dall'astensionismo alla crescente sfiducia dei cittadini nella partecipazione nelle istituzioni politiche; dallo spostamento della funzione legislativa dal Parlamento al Governo alla pessima qualità della produzione normativa; dal ridursi dei luoghi della partecipazione critica e riflessiva al contestuale diffondersi di movimenti e pratiche populiste. Abbiamo insomma proposto di fare insieme una fotografia della situazione esistente e, una volta individuati i problemi e gli scostamenti dal dover essere costituzionale, di provare a discutere delle soluzioni che appaiono, anche alla luce dell'esperienza di altri Paesi, più ragionevoli ed efficaci per ridurre tali scostamenti e dare così più piena attuazione al modello di democrazia pluralista ed emancipante descritto e prescritto dalla nostra Costituzione. La risposta sono stati il silenzio, l'accelerazione dei lavori con la moltiplicazione delle sedute - come ben sa il presidente Balboni e l'indisponibilità a mettere in discussione un testo contraddittorio che, man mano che lo si analizza, appare sempre più problematico e incompatibile con i fondamentali princìpi della democrazia pluralista e della separazione e della limitazione del potere sanciti nella nostra Costituzione e in tutte le Costituzioni europee approvate all'indomani della tragica esperienza delle due guerre e delle diverse dittature nazionali. Vi abbiamo cioè proposto, anche attraverso la presentazione di specifici emendamenti e di diversi disegni di legge ordinari e costituzionali, di discutere sul come dare oggi, nell'attuale contesto economico e sociale, una più piena ed effettiva attuazione alla Costituzione e al modello di democrazia che essa delinea e prescrive, che significa innanzitutto garantire a ogni persona le condizioni materiali e culturali per poter tutti i giorni partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Voi avete risposto proponendo di risolvere lo scarto tra l'essere e il dover essere costituzionale che i cittadini e tutti noi qui sperimentiamo abrogando il dover essere costituzionale, rinunciando alla più grande conquista di libertà individuale e collettiva del secondo Dopoguerra, che è appunto la democrazia partecipativa e pluralista e i suoi corollari, che sono - come è noto - la limitazione e la separazione del potere, la primazia del Parlamento e la costruzione dell'unità, attraverso processi partecipativi diffusi, animati e organizzati dai corpi intermedi e dai partiti politici. Signora Ministra, con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e la contestuale elezione di una sua maggioranza parlamentare eletta per trascinamento si passerà dalla primazia del Parlamento e del pluralismo, che in esso trova rappresentanza e composizione, alla primazia del Governo e in particolare dell'uno o dell'una; una primazia di legittimazione e una primazia di poteri del Presidente del Consiglio che modifica e stravolge la natura e la funzione del Parlamento. La composizione di quest'ultimo dipenderà, infatti, dalla elezione del Presidente del Consiglio e la sua durata in carica dalla volontà del Presidente del Consiglio eletto. La composizione delle Camere - come vi abbiamo più volte sottolineato e come ci hanno sottolineato tutti gli esperti che abbiamo audito - non dipenderà più solo dal voto che i cittadini esprimeranno per eleggere i deputati e i senatori; questi saranno non più eletti direttamente, in conseguenza di un voto espresso dai cittadini su di loro, come prescrivono gli articoli 56 e 58 della Costituzione, ma in conseguenza di un voto espresso sul Presidente del Consiglio. Anche la durata del mandato parlamentare dipenderà non più dalle stesse Camere, ma dalla volontà del Presidente del Consiglio, che potrà in qualsiasi momento chiedere e ottenere dal Presidente della Repubblica il loro scioglimento. Si determinerà così, onorevoli colleghi, una concentrazione del potere in una sola figura, il Presidente del Consiglio, che non ha eguali in nessuna democrazia costituzionale contemporanea. L'elezione del Parlamento per trascinamento, come riflesso del Presidente del Consiglio, consentirà a quest'ultimo di disporre di una maggioranza in grado di eleggere anche il Presidente della Repubblica, i cui poteri - come dirò fra breve - saranno comunque inevitabilmente ridotti.

avranno più potere, perché potranno, appunto, scegliere direttamente il Presidente del Consiglio, e che le istituzioni politiche saranno così più stabili e più forti. Onorevoli colleghi, noi crediamo che sia esattamente il contrario. I cittadini avranno meno potere e le istituzioni politiche saranno più rigide, meno rappresentative, meno capaci, quindi, di comporre democraticamente i conflitti sociali e, di conseguenza, saranno più fragili e più deboli. La riforma, nel disporre la fine della centralità del Parlamento e il superamento della forma di governo parlamentare, certifica l'esplicita e definitiva rinuncia alla costruzione dell'unità dal basso, attraverso il protagonismo organizzato dei cittadini e un processo di continue mediazioni e sintesi; una rinuncia radicale alla fatica della mediazione che, in un contesto plurale, finisce inevitabilmente con il ridurre, anziché ampliare, il potere politico dei cittadini e la loro possibilità di partecipare, sostanzialmente e quotidianamente, alla determinazione dell'indirizzo politico. I cittadini, ogni cinque anni, saranno solo chiamati ad eleggere - anche se dovremmo forse dire acclamare - un capo o una "capa" e a conferirgli o a conferirle quasi ogni potere, fissando, al contempo, un indirizzo politico che non potrà, nel corso del tempo, essere ridefinito, ripensato, adeguato ai mutamenti e alle trasformazioni sociali, se non attraverso un nuovo passaggio elettorale e una nuova investitura del capo. Ci sarà un vincitore o una vincitrice e ci saranno molte persone sconfitte; in realtà quasi tutte, perché anche chi avrà votato per il Presidente del Consiglio eletto si sarà spogliato, come cittadino, di quasi ogni potere politico. La famosa considerazione di Rousseau sulla democrazia inglese sembra descrivere proprio ciò che la riforma rischia di determinare. Gli inglesi - osservava Rousseau - che pure conoscono perfettamente i rappresentanti della loro contea, della loro città e dei loro borghi, credono di essere liberi. Si sbagliano di grosso. In realtà - diceva sempre Rousseau - lo sono solo nel giorno in cui votano, perché subito dopo sono servi di coloro che hanno votato. L'effetto di ridurre la partecipazione politica e la democrazia rappresentativa alla scelta del capo e il Parlamento ad una proiezione di quest'ultimo è proprio quello di ridurre ulteriormente la sovranità politica dei cittadini e la loro possibilità di far valere i molteplici e diversi punti di vista e interessi che esprimono e che caratterizzano ogni società libera e pluralista. Onorevoli colleghi, la riduzione della partecipazione democratica alla scelta del capo rischia appunto di rendere le istituzioni politiche non solo meno plurali, meno rappresentative e quindi meno democratiche, ma anche più fragili. L'elezione diretta del Capo del Governo rischia, infatti, di incentivare pratiche populiste e demagogiche che, nell'immediato, possono dare l'impressione di sopperire alle difficoltà della partecipazione organizzata e alla frammentazione politica, alla fine, si dimostrano incapaci di conferire alle istituzioni quella forza e quella legittimazione di cui necessitano per governare e orientare le dinamiche economiche e sociali all'interesse generale e alle ragioni del pieno sviluppo della persona umana e dell'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La forza e la capacità di governo effettivo delle istituzioni politiche dipendono dalla loro capacità di interpretare attese e domande sociali, dal loro radicamento, dalla loro capacità di promuovere processi di integrazione politica reali e sostanziali. Istituzioni politiche che si reggono su un consenso immediato, sulle paure, sulle emozioni e sulle pulsioni più irrazionali, più irrazionali, difficilmente sono in grado di governare davvero i processi economici e sociali e di orientarli all'interesse generale e al pieno sviluppo della persona umana. Le considerazioni e le preoccupazioni che ho appena sintetizzato abbiamo cercato come senatori del Partito Democratico

e far emergere le molte contraddizioni, i presupposti culturali, inequivocabilmente illiberali e organicisti, e soprattutto i molteplici effetti negativi della proposta di riforma. Qual è stata la risposta? Sempre il silenzio o, peggio, il rivendicare la forza dei numeri e il diritto di approvare ciò che volete, perché lo avevate promesso ai vostri elettori e avete vinto le elezioni, come se la posta in palio delle elezioni potesse essere la Costituzione e i suoi fondamentali principi che disciplinano la democrazia. Perché ricorrere a un simile argomento che contrasta in maniera evidente con la natura di qualsiasi vero confronto costituzionale? Perché una così radicale indisponibilità a ridiscutere e a riconsiderare gli aspetti più contraddittori, irragionevoli e pericolosi della riforma? La risposta - o, se vogliamo, il silenzio alle nostre critiche e considerazioni - sta probabilmente nello scambio tra autonomia differenziata e premierato, che avete siglato. un patto che vi ha impedito e vi impedisce di discutere liberamente e nel merito di ciascuno dei due provvedimenti. mesi fa avete votato un testo senza ascoltare il rilievo degli esperti, delle parti sociali, della Banca d'Italia, dell'Ufficio parlamentare di bilancio e dei diversi componenti del *club* che pure si sono dimessi, perché quello era il testo pattuito, così oggi state per votare un testo contraddittorio e di difficile applicazione che - come abbiamo cercato di evidenziare e hanno evidenziato quasi tutti gli esperti - viola fondamentali principi costituzionali, perché questo è il testo che avete pattuito. un testo che peraltro - come ben sapete - oltre a violare fondamentalissimi principi costituzionali, contiene varie sgrammaticature e contraddizioni interne, dalla distinzione, ad esempio, degli effetti della rottura del rapporto di fiducia, a seconda che ciò avvenga a seguito di una mozione di sfiducia oppure a seguito della bocciatura di una proposta su cui il Governo ha posto la questione di fiducia - come tuttora parrebbe prevedere l'articolo 4 alla possibilità che nasca un Governo sostenuto da una maggioranza diversa da quella originariamente collegata al Presidente del Consiglio direttamente eletto oppure che nasca un Governo presieduto da un Presidente del Consiglio che nessun cittadino ha eletto, come consente lo stesso articolo 4. 4. E non dimentichiamo l'incertezza degli effetti dell'eventuale proposta di scioglimento della Camera, avanzata dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica. Il secondo comma prevede, infatti, che il Presidente del Consiglio possa proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, signora Ministra, è obbligato a sciogliere? A rigore, una proposta può ricevere anche una risposta negativa, altrimenti non è una proposta. Se si dovessero prendere sul serio le sue parole, Ministra, e le parole del Governo, con le quali avete sostenuto che la riforma non intacca in alcun modo gli attuali poteri del Presidente della Repubblica, la risposta allora sarebbe obbligata e il Presidente della Repubblica potrebbe tranquillamente respingere la proposta del Presidente del Consiglio dimissionario. In realtà, sapete bene che non è così. La *ratio* della riforma è esattamente opposta e, al di là delle numerose sgrammaticature, è chiara nel sottoporre il Parlamento al Presidente del Consiglio e nell'attribuire a quest'ultimo il potere di determinare la composizione, e quindi la nascita e la durata del primo. Il testo giunto qui in Aula lascia poi senza risposta l'interrogativo che abbiamo più volte sollevato sul come si possa garantire, in entrambe le Camere, la maggioranza almeno assoluta dei seggi alle liste collegate al Presidente del Consiglio eletto e, al tempo stesso, garantire che le medesime liste non ottengano un numero di seggi sproporzionato, e dunque incostituzionale, rispetto ai voti ottenuti. Così com'è rimasto senza soluzione il problema dell'incidenza del voto dei cittadini italiani che stabilmente, o da sempre, vivono all'estero, il cui numero, in forza dell'attuale legge sulla cittadinanza, è destinato a crescere, e il cui voto potrebbe diventare determinante per eleggere il Presidente del Consiglio e, di conseguenza, l'intero Parlamento. Al Governo - mi rivolgo a lei, signora Ministra - e alla sua maggioranza diciamo dunque: fermatevi, non abusate della forza dei numeri. La democrazia pluralista e partecipativa, che con tanti sacrifici è stata conquistata, attraverso la lotta di liberazione e il compromesso costituzionale, da tutte le forze politiche, democratiche e antifasciste *(Applausi)*, al nostro Paese di rimanere unito anche nei momenti più difficili e di crescere e progredire. Ad essa, alla democrazia pluralista, a un bene così prezioso, non credo che gli italiani vogliano rinunciare tanto facilmente. Noi, per parte nostra, a una simile riforma ci opporremo con tutta la determinazione necessaria e ci adopereremo per dare alla Costituzione e ai fondamentali principi che in essa sono sanciti, a tutela del pluralismo, della partecipazione critica e riflessiva e della separazione e limitazione del potere, una più effettiva e solida attuazione. Come ben sappiamo, se tali princìpi non sono garantiti, alla fine non c'è libertà, non ci sono diritti e non c'è neppure la possibilità di un giusto e duraturo benessere economico.

il 3 novembre il Consiglio dei ministri, su proposta di Giorgia Meloni e del ministro Alberti Casellati, ha approvato il disegno di legge di modifica costituzionale recante l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. Oggi, dopo cinque mesi di dialogo, di ascolto, confronto, audizioni e miglioramento del testo base, giunge in Aula il testo n. 935 di iniziativa governativa, approvato nella Commissione affari costituzionali di cui faccio orgogliosamente parte. Una riforma costituzionale ha per definizione un tempo lunghissimo: un tempo del dialogo, del confronto e di un approfondimento, innanzitutto tra le forze politiche, con i sindacati, gli investitori, gli imprenditori, le Regioni, i sindaci, cosa che il Ministro ha fatto. Un secondo passaggio è quello del confronto nelle sedi istituzionali, quali la Commissione e il Parlamento. Il Ministro ha svolto tutto questo, come da manuale, nel primo anno di legislatura e dopo è arrivato il testo in Commissione. In Commissione, il presidente Alberto Balboni, che è anche relatore del provvedimento, con grandissima competenza e soprattutto massima disponibilità verso tutti, ha guidato i lavori,

Nell'articolo 2 abbiamo modificato l'articolo 83, terzo comma, dove viene previsto l'abbassamento del *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica a partire dal sesto scrutinio e non più dal terzo. L'articolo 3 modifica il primo comma dell'articolo 88 e sopprime la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due Camere. Un emendamento approvato in Commissione aggiunge un comma che modifica il secondo comma dello stesso articolo e stabilisce che il divieto di procedere allo scioglimento delle Camere nell'ultimo L'articolo 4 sostituisce il primo comma dell'articolo 89 e riguarda la controfirma degli atti del Capo dello Stato, cioè gli atti saranno controfirmati dai Ministri che se ne assumono la responsabilità e si lascia l'elenco degli atti che non necessitano di controfirma. L'articolo 5 sostituisce l'articolo 92 della Costituzione e, mantenendo il primo comma, si introduce la previsione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri a suffragio universale e diretto per cinque anni. Si pone un limite di mandato (due mandati), e solo in un caso possono diventare tre: qualora nelle precedenti legislature si sia svolto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi.

In base all'ultimo comma del nuovo articolo 92, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico a formare il Governo al Presidente del Consiglio eletto e quindi, su proposta di quest'ultimo, nomina e revoca i Ministri. L'articolo 6 è stato inserito in sede di Commissione e integra il primo comma dell'articolo 57. L'articolo 7 modifica l'articolo 94 e introduce una disposizione alla lettera *a)* in base alla quale, nel caso non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo e, qualora non lo ottenga, procede allo scioglimento delle Camere. Alla lettera *b)* si aggiunge che, nel caso di revoca di fiducia al Presidente del Consiglio con mozione motivata, il Presidente può sciogliere le Camere. In caso di dimissioni del Presidente, previa informativa parlamentare, può proporre entro sette giorni lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica. Qualora però il Presidente del Consiglio non voglia esercitare tale facoltà, il Presidente della Repubblica può, per una sola volta nel corso della legislatura, conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente dimissionario o ad altro parlamentare collegato al Presidente eletto; facoltà peraltro prevista anche in caso di morte, di impedimento permanente o decadenza del Presidente del Consiglio eletto. L'articolo 8 prevede che restino in carica i senatori a vita eletti prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale e, al secondo comma, si prevede che la legge si possa applicare dalla data del primo scioglimento o cessazione delle Camere successive all'entrata in vigore della stessa. Ho elencato tutti gli articoli innanzitutto per entrare nel merito del provvedimento e per sintetizzare che questa riforma ha dei chiari obiettivi: stabilità dei Governi, consolidamento della democrazia, coesione degli schieramenti elettorali e cancellazione del fantomatico trasformismo parlamentare. che dal 1948 ad oggi abbiamo avuto sessantotto Governi guidati da trentuno Presidenti del Consiglio. Chiaramente ci sono stati un'instabilità per la nostra Nazione, un indebolimento dell'Italia e del sistema Paese e soprattutto l'impossibilità, per qualsiasi Governo e qualsiasi Presidente, di mettere in atto una politica estera e industriale che ovviamente non è mai decollata. Serve uno sforzo maggiore da parte di tutti per modificare le norme. In Commissione, in realtà, abbiamo ascoltato tantissimi interventi da parte dei membri delle opposizioni e, insieme ai miei colleghi di maggioranza, che siamo stati veramente sempre presenti, vorrei dire che molti di questi interventi sono risultati solo delle prese di posizione ideologiche. Noi, come Gruppo Fratelli d'Italia e come maggioranza, crediamo fortemente nelle istituzioni e abbiamo un grandissimo senso di responsabilità verso quei cittadini che ci hanno affidato questo compito. Vorrei ricordare che da adesso in avanti comincia un lavoro importante, parallelamente a tutti i comitati civici che sono già nati in maniera spontanea. Vorrei ricordare che negli ultimi quindici giorni abbiamo presentato il comitato civico di Roma, di Rimini, di Ferrara, di Campobasso e tanti altri che stanno nascendo. Insieme a a loro abbiamo la responsabilità di fare informazione, di informare i cittadini non con le *fake news*, come è avvenuto negli ultimi diciotto mesi. Abbiamo la responsabilità di parlare non solo a quei cittadini che hanno il dovere di votare e che esercitano anche un diritto, ma soprattutto a quelli che non si sono recati alle urne, perché troppo spesso ascoltiamo delle ricostruzioni creative e fantasiose. In conclusione, Presidente, ribadisco con chiarezza l'importanza di questa riforma, per il semplice motivo che abbiamo bisogno di stabilità, di credibilità in Italia e anche all'estero e soprattutto, non cambiando i poteri del Presidente della Repubblica - come le opposizioni raccontano - abbiamo bisogno di maggiore democrazia. Con questa riforma mettiamo al centro l'elettore, che avrà la possibilità di scegliere da chi farsi rappresentare. Presidente, il mio è il primo intervento del Gruppo Fratelli d'Italia in discussione generale. Le considerazioni politiche ovviamente le farà il capogruppo Marco Lisei in dichiarazione di voto. Però mi consenta di soffermarmi su alcuni aspetti che mi hanno molto colpito e soprattutto di rispondere, per il suo tramite, al senatore Boccia per l'intervento di ieri. Il senatore Boccia non fa parte, ovviamente, della Commissione affari costituzionali, ma ha esordito dicendo che noi membri di maggioranza, di cui faccio parte, siamo stati supini durante i lavori d'Aula. Due considerazioni vorrei condividere innanzitutto con l'Aula, ma soprattutto con gli italiani a casa. Innanzitutto gli interventi dei membri di opposizione sono stati tanti, è vero, l'ha detto poco fa il senatore Giorgis - sono stati interventi che hanno avuto il *focus* solo sul tema dell'accordo-scambio con l'autonomia, quasi fosse un *mantra*. Vorrei ricordare 76 sedute di Commissione, 2.600 emendamenti, cinque mesi di discussioni. Questi sono fatti documentati. Cosa avremmo dovuto fare? A novembre il testo è stato approvato dal Consiglio dei ministri e, solo perché ci sono le elezioni europee, avremmo dovuto lasciare stare tutti i lavori e fermarci? Non credo: gli italiani ci hanno eletto per altro.

Il vero impegno, tra i nostri alleati, è rispettare la volontà degli elettori. Una seconda considerazione mi preme condividere. Mi dispiace, soprattutto come essere umano, ma anche come donna delle istituzioni e oggi anche come mamma, aver ascoltato ieri dal Capogruppo del Partito Democratico interventi nei quali si sono usati termini squalificanti per tutti. *(Applausi)*. Quindi mi chiedo, il Partito Democratico, oggi a guida di Elly Schlein, si ricorda delle battaglie di civiltà solo in occasione delle giornate ufficiali? Usare il termine "supino" - cito la frase testuale: "siete stati assenti, silenti e supini" - in questa autorevole Aula offende tutti. Mi scuso io per tutti con gli italiani, soprattutto per il messaggio sbagliato che abbiamo mandato alle giovani generazioni. Noi dovremmo essere i primi a dare un esempio, anche nel linguaggio. conclusione che in ogni campagna elettorale abbiamo sentito dire da tutte le forze politiche che l'Italia ha bisogno di riforme, che l'Italia ha bisogno di tante riforme per uscire dall'immobilismo. Concludo, con orgoglio, citando le parole di Giorgia Meloni: questa è la riforma madre di tutte le riforme. Noi siamo pronti, Fratelli d'Italia è pronta e gli italiani lo

la mia contrarietà e la contrarietà di Azione a questa riforma costituzionale sul premierato è sia nel metodo che nel merito. il metodo, nella saggezza dei nostri Padri e delle nostre Madri costituenti la procedura di revisione rinforzata, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, impone una doppia deliberazione di entrambi i rami del Parlamento, con un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi. La *ratio* di questa rigidità costituzionale era quella di richiedere scelte largamente condivise, meditate, equilibrate, con la più ampia partecipazione possibile sul procedimento che tocca la Costituzione non solo delle forze politiche e parlamentari, ma anche dell'opinione pubblica, con il coinvolgimento dei costituzionalisti, della società e dei corpi intermedi. Voglio essere chiaro: io credo fermamente che il ruolo parlamentare che oggi ognuno di noi *pro tempore* riveste sulla base del principio della rappresentanza, in nome e per conto del popolo italiano, ci richieda in primo luogo di rispettare la Costituzione. che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti e nelle forme previste dalla nostra Costituzione e dalla legge. La forza della democrazia liberale, prevista nella nostra forma repubblicana di tipo parlamentare, si misura, da un lato, nella tutela delle minoranze contro la tirannia delle maggioranze e, dall'altro, nella tutela della capacità della maggioranza di decidere senza essere ostaggio della tirannia delle minoranze. Questo è l'impianto pluralista della nostra democrazia e il ruolo di custode della democrazia rappresentativa è affidato al Parlamento. Il Parlamento, non il *Premier*, è il custode della sovranità popolare. La sacralità della Costituzione non va confusa con la sua immutabilità. Tutte le forze politiche hanno cercato di cambiare la Costituzione, sia il centrodestra che il centrosinistra; non sarebbe intellettualmente onesto dire che la Costituzione è sacra e non va modificata solo quando la cambiano gli altri, mentre invece andava bene modificarla quando nel passato l'ha fatto o ha cercato di farlo il centrosinistra quando era al Governo. La Costituzione è sacra, ma non è immutabile. La Costituzione si può cambiare, anzi si deve cambiare, ma bisogna farlo insieme, non a colpi di maggioranza. Le regole della nostra casa comune si cambiano e si scrivono insieme, non si cambiano in corsa, mentre il Paese è distratto, con una campagna elettorale alle porte, caricando il messaggio dei pieni poteri, il vecchio vizio, il peccato di *hybris*, la tracotanza come la chiama la letteratura greca, che ci ricorda come ubriaca sempre e da sempre chi è al potere. Noi siamo contrari a questa riforma costituzionale, non perché sia illegittima o incostituzionale, ma perché è sbagliata nel metodo e nel merito. Fermatevi, fermiamoci, perché siamo ancora in tempo. Noi come Azione ci opporremo con tutte le nostre forze, ma come sempre non ci limitiamo a dire solo no, non va bene, noi abbiamo il dovere morale, quando diciamo di no, di proporre un'alternativa. Nel metodo noi riteniamo che ci sia una via maestra per riformare l'impianto costituzionale in modo organico. Una via maestra garante di una discussione accesa e animata, ma alta, meditata e plurale. Questa via si chiama Assemblea costituente. Fermiamoci ed eleggiamo insieme un'Assemblea costituente in grado di coinvolgere le migliori energie del costituzionalismo italiano, che non abbia il tema della propria rielezione, ma che abbia il compito di elaborare in sei mesi un testo organico e condiviso di riforma costituzionale. Vengo al merito: la riforma del premierato che ci proponete è sbagliata perché definisce una forma di governo ibrida, fuori dagli schemi della dottrina costituzionale e comparatista. Voglio farvi una domanda. Ma se in tutto il mondo non esiste un solo Paese che abbia adottato la forma di governo che voi state proponendo, siamo noi gli unici geni oppure la verità è che questo sistema ibrido è claudicante ed è per questo che non funziona? Guardate cosa è successo in Israele dove, quando è stata adottata questa misura, ha dimostrato un voto separato tra il voto al *Premier* e il voto nel Knesset, che ha aumentato la frammentazione. frammentazione. L'errore di fondo di questa proposta è che confondete un problema giusto e condivisibile perché strutturale del nostro sistema italiano, cioè la stabilità del Governo, con una soluzione fuorviante e sbagliata, cioè la stabilità del *Premier*, la stabilità del Capo del Governo. C'è una grande differenza di fondo che è valoriale: per voi, la forza della democrazia si misura nella forza della maggioranza e del *Premier*, mentre per noi la forza della democrazia decidente si misura nella forza dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti, nella tutela delle minoranze dalla tirannia della maggioranza, nella maggioranza, nella tutela della maggioranza anche rispetto alla tirannia delle minoranze. Ricordiamoci sempre che in fisica la forza di una catena si misura dal grado di resistenza del suo anello più debole.

restituisce la dignità al Parlamento attraverso l'introduzione del meccanismo della sfiducia costruttiva; vi proponiamo di introdurre una nuova legge elettorale proporzionale che restituisca ai cittadini la possibilità di scegliere, non alle segreterie dei partiti, dei partiti, con una soglia di sbarramento alta (al 5 per cento) per coniugare il principio della rappresentanza senza favorire l'eccessiva frammentazione e il trasformismo; vi proponiamo di salvaguardare le prerogative del Presidente della Repubblica, dal momento che voi continuate a dire che la riforma del premierato non tocca i poteri del Presidente della Repubblica, la figura più autorevole, il garante dell'unità del Paese, la figura in cui tutti gli italiani hanno più fiducia. Come fate a dire che non si toccano le prerogative del Presidente della Repubblica, se abrogate il potere delle consultazioni presidenziali attraverso l'elezione diretta del *Premier*, se cancellate il potere di scioglimento anticipato delle Camere, se eliminate la nomina dei senatori a vita? Pensate veramente che continuando a raccontare una bugia possiate trasformarla in una verità? Gli italiani non vi crederanno per questo. Fermatevi, fermiamoci, apriamo un dibattito per eleggere un'Assemblea costituente in grado di presentare una riforma della Costituzione alta, organica, condivisa. Apriamo il dibattito sul cancellierato alla tedesca per garantire la stabilità del Governo ma salvaguardare le prerogative del Parlamento e della Presidenza della Repubblica. Fermatevi nell'interesse generale, ma vi dirò di più:

Avrete la forza di approvare la riforma in seconda lettura? Sì, ce l'avrete, ma non riuscirete ad approvarla con il *quorum* dei due terzi previsto dalla Costituzione per evitare il *referendum*, perché su questo le opposizioni, anche se sono divise, devono marciare unite, e devono farlo quando tra un anno gli italiani saranno chiamati a esprimersi e vi dimostreremo, anzi, ve lo dimostreranno loro quanto costa caro il peccato dell'arroganza e della tracotanza di chi ha il potere, perché la sovranità popolare vince sull'idea dei pieni poteri e vince sulla tirannia di tutte le maggioranze. Fermatevi, fermiamoci, oggi siamo ancora in tempo, altrimenti a fermarvi saranno gli italiani con un *referendum* abrogativo del premierato.

ho ascoltato gli interventi dei colleghi e delle colleghe che mi hanno preceduto e ho letto con particolare attenzione l'atto Senato 935 in merito alle modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. Ebbene, più approfondisco la tematica, più mi viene in mente un famoso proverbio latino: *mors non est finis*, al peggio non c'è mai fine, che suggerisce che, sebbene non importi quanto grave possa sembrare una situazione, vi è sempre il potenziale per peggiorare ulteriormente. Devo dire che, quale Capogruppo in Commissione giustizia per il Movimento 5 Stelle, sono già abituata ad essere testimone (e sono testimone, vista la aprioristica riluttanza di questa maggioranza e di questo Governo ad accogliere qualche nostro preciso quanto fondato suggerimento)

che effettivamente renda la giustizia veloce, efficiente e certa, nel rispetto dei diritti di tutti. Questo Governo, che è come un gambero che fa passi indietro, proponendo una giustizia che calpesta i diritti delle vittime dei reati, ma anche degli indagati e degli imputati, diventa sorprendentemente una lepre quando c'è da creare, di converso, una giustizia debole con i forti, con i colletti bianchi e con chi detiene le leve del potere. *(Applausi)*.

fumo, un pericoloso fumo. Giorgia Meloni ha definito il premierato come la madre di tutte le riforme, è una scelta disastrosa e pericolosa per il Paese. Si tratta di un'alterazione dell'equilibrio dei poteri costituzionali che mina il sistema di controlli e bilanciamenti previsti dai nostri Costituenti. Questa proposta, signora Presidente, enfatizza il ruolo del *Premier* a discapito del Parlamento e del Presidente della Repubblica, indebolendo così le istituzioni democratiche. La riforma del premierato promette stabilità elettorale e governativa, ma in realtà può portare ad instabilità e incertezza. Molti costituzionalisti stanno criticando aspramente questa proposta, in quanto la riforma erode i poteri del Parlamento, lasciando il Paese praticamente guidato da un *Premier* con pochi controlli. è un serio pericolo per la democrazia e i princìpi costituzionali. Si ridisegna il quadro istituzionale per favorire un ritorno a un potere politico centralizzato e autoritario. Con uno sguardo al passato e ai Paesi esteri, perdendo di vista il nostro impianto e l'equilibrio tra i poteri, si intende distruggere la nostra Costituzione, concentrando tutto il potere nel Presidente del Consiglio, che potrà decidere del destino delle Camere. Il Parlamento sarà assoggettato al *Premier*, perché è chiaro che se stanno insieme cadono insieme. Sarà il *Premier* a poter esercitare un potere di ricatto sul Parlamento. Stiamo andando verso una prospettiva che non porterà stabilità, ma solo più poteri al Presidente del Consiglio, che già ne ha tanti. Ricordo che oggi, con la decretazione d'urgenza e i decreti legislativi, la funzione legislativa è in capo al Governo. Di certo non potremo più avvalerci della funzione di garanzia attribuita al Presidente della Repubblica, che assurgerà a mero passacarte o cerimoniale. solo, quindi, di un *Premier* eletto dai cittadini e chiaramente più forte al cospetto del Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento, che quindi potrebbe far valere questo suo peso ogni volta che lo ritenga; tuttavia, circostanza ancora più importante, i cittadini perderebbero la loro autorevole figura di riferimento e garanzia, volta a intervenire per arginare in modo imparziale quelli che potrebbero essere gli interventi posti in essere in disprezzo dei nostri ad oggi tutelati e garantiti diritti. Al *Premier* viene assegnato il potere di chiedere e ottenere lo scioglimento delle Camere, togliendo così una prerogativa fondamentale al Quirinale, dandola a chi ha già grandi poteri. È veramente pericoloso indebolire questa figura di riferimento, tanto più in una fase di particolare fragilità sociale, tensioni e conflitti, determinata anche dalle radicali trasformazioni in corso. Non solo, quindi, viene svilita la figura del Presidente della Repubblica, ma consideriamo anche il fatto che le Camere sono sotto scacco del *Premier.* infatti, un palese colpo all'equilibrio tra i poteri il fatto di prevedere che sia il capo del Governo a decidere lo scioglimento del Parlamento, che così diventa un organo perennemente sotto ricatto; inoltre, il Parlamento verrebbe letto al traino del *Premier,* creando una maggioranza al guinzaglio del Governo che, invece di essere un'espressione della sovranità popolare, diventa una mera appendice del Governo. Qualsiasi riforma si voglia prendere in considerazione, non dovrà mai mortificare la funzione del Parlamento, che è molto utile per garantire l'inclusività e la composizione dei conflitti. il Parlamento ha bisogno di alcuni correttivi che abbiano la capacità di restituire la centralità e l'operatività che la Costituzione gli assegna *(Applausi)*; attività in questa legislatura più volte svilita da una facile decretazione d'urgenza.

non è da sottovalutare, poiché, oltre a mortificare la figura del Presidente della Repubblica ed il Parlamento, si incastra perfettamente con altre proposte che mirano a limitare l'indipendenza della magistratura e a depotenziarla e a concentrare il potere decisionale nelle mani dell'Esecutivo. Basti semplicemente pensare alla proposta in merito alla separazione delle carriere o piuttosto a quella relativa alla composizione del CSM. In merito alla prima proposta, al netto della circostanza della riduzione delle garanzie per gli imputati, se i pm escono dal perimetro comune con i giudici, se si allontanano dalla cultura della giurisdizione, se perdono interesse rispetto all'esito del processo e diventano una figura unicamente deputata al sostegno dell'accusa, dell'accusa, saranno ridotti al terminale processuale della Forza di polizia giudiziaria, a sua volta sottoposta al comando e all'impulso del Governo. Avremmo, chiaramente, un pubblico ministero prevalentemente radicato nella cultura e nella prassi di polizia. Quindi, diventa chiaro che l'intento vero è un altro: quello di sganciare i pm dalla magistratura autonoma e indipendente, dal potere terzo rispetto all'esecutivo e al legislativo, e di portarli sotto l'influenza diretta del Governo e del Ministero della giustizia in particolare. Non a caso, tra gli altri loro intendimenti più volte annunciati vi è il superamento dell'obbligatorietà dell'azione penale, lasciando che sia la maggioranza di turno a decidere su cosa si deve indagare. In merito alla composizione del CSM, che sappiamo essere l'organo di autogoverno del potere giudiziario, oggi autonomo e indipendente, viene da questa maggioranza prevista, di riflesso, tenuto conto dell'intento di procedere alla separazione delle carriere, l'istituzione di due differenti Consigli superiori della magistratura. Questi due organi di autogoverno, invece di essere composti per un terzo da laici e per due terzi dai togati, saranno composti al 50 per cento da membri togati e al 50 per cento da laici, cioè i membri scelti dalla politica. Ecco un altro tassello dell'influenza del potere politico sulla magistratura. cento dei laici sarebbe scelto per metà dal Parlamento e per metà dal Presidente della Repubblica. Quest'ultimo è garanzia di terzietà: oggi sì, ma domani, con la riforma del premierato, che prevede un *Premier* eletto dai cittadini, con al suo rimorchio una maggioranza parlamentare preconfezionata del 55 per cento, è chiaro che al Quirinale ci sarà una persona eletta dalla sola maggioranza di turno in base a convenienze di parte. Ecco come tutto si regge insieme. L'elezione diretta del *Premier* comporterebbe uno stravolgimento della Carta e dell'assetto istituzionale. Non è quello di cui l'Italia ha bisogno e non serve questo per risolvere le criticità del sistema. Un *Premier* è inamovibile. Stiamo andando verso una soluzione che non esiste in nessun altro Paese del mondo e vi sarà una ragione se questo esempio non viene accolto da nessun altro Paese. Noi non ci stancheremo mai di illuminare i cittadini, ai quali è stato gettato il fumo negli occhi, al fine di evidenziare i fondati timori e rischi. La necessità di intervenire con interventi mirati e chirurgici perché siamo convinti che i Governi debbano avere più stabilità. Questo risultato, però, può raggiungersi solo con il rafforzamento del Parlamento e con una maggiore partecipazione democratica dei cittadini. Presidente, per questo noi abbiamo presentato una serie di proposte. La sfiducia costruttiva, la fiducia del Governo a Camere riunite, il potere al *Premier* di proporre al Presidente della Repubblica la revoca dei Ministri: sono tre soluzioni che darebbero stabilità al Governo, mettendolo al riparo da crisi al buio e giochi di palazzo. Se a ciò aggiungiamo i limiti all'uso dei decreti-legge, che diventerebbero veramente provvedimenti emergenziali e dal contenuto omogeneo, il vaglio obbligatorio preventivo della Corte costituzionale sulle leggi elettorali e i diritti dell'opposizione inseriti in Costituzione, in Costituzione, arriveremmo a rafforzare il ruolo del Parlamento nel rapporto con il Governo e a tutelare il pluralismo e lo spazio delle minoranze nelle Camere. In conclusone, signor Presidente, la situazione richiede una forte mobilitazione e un'opposizione compatta, per contrastare questa deriva autoritaria che stanno proponendo questo Governo e questa maggioranza. Il MoVimento 5 Stelle c'è

colleghi, siamo qui oggi a discutere di una questione molto seria, perché è importante che i cittadini a casa e gli studenti che ci ascoltano capiscano cosa c'è in gioco oggi: non è in gioco una cosa qualsiasi, ma stiamo discutendo di una modifica della legge costituzionale che è la legge fondamentale, su cui si fonda il patto costitutivo tra la Repubblica, i suoi cittadini e l'equilibrio delle istituzioni, quindi è un elemento che andrebbe trattato con grande attenzione e con grande delicatezza. Va anche ricordato con forza che la Costituzione non è fatta di due parti, come spesso si è sentito dire, ma è un *unicum*, nel senso che i principi e i doveri i contenuti nella prima parte poi trovano una loro realizzazione e una loro applicazione concreta nella seconda parte. Pensare quindi di modificare la seconda parte dicendo che tanto si stanno facendo modifiche che non riguardano i diritti e i doveri è una falsificazione della realtà. I diritti e i doveri - come il diritto alla sussidiarietà e il diritto al protagonismo delle autonomie, sanciti nella prima parte - vengono garantiti da passi successivi, che si trovano nella seconda parte, quindi la declinazione

come purtroppo stiamo facendo in questo momento, senza tenere presente che il principio dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica è contemplato in maniera forte nella prima parte. Altrimenti, se si pensasse di ridurre questa discussione a un fatto tecnico ad esempio la modalità di elezione del Presidente del Consiglio - si commetterebbe un grande errore politico. La Costituzione non va giudicata a pezzi, ma nel suo insieme e la responsabilità delle modifiche della seconda parte ha conseguenze rilevantissime rilevantissime sulla prima. In primo luogo, di cosa stiamo parlando? Parliamo della legge fondamentale della Repubblica, che come obiettivo fondamentale ha il fatto di promuovere una democrazia sostanziale dei cittadini, cioè la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica il fatto che la Repubblica cresce, è fondata sul lavoro e sui diritti e i doveri dei cittadini e cresce man mano che il cittadino diventa sempre più consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri e dà il suo contributo fattivo nei mezzi, con le possibilità che ha, per la costruzione di questa grande casa comune che è la nostra Repubblica. Perché fu scelta questa strada? Esattamente perché il fascismo e la guerra avevano mostrato come la manipolazione dei cittadini, l'uso del popolo - non la crescita del popolo nella sua consapevolezza democratica

potessero rappresentare un pericolo gravissimo non solo appunto per la libera espressione delle persone (abbiamo ricordato recentemente l'omicidio di Giacomo Matteotti), ma anche e soprattutto per la pace e per il mantenimento dei diritti fondamentali. Allora questo elemento fondativo della Prima Repubblica, che è appunto la democrazia sostanziale, come la chiamava Giuseppe Dossetti, cioè il fatto che in tutti i modi si promuovessero forme di partecipazione, oggi viene riportato indietro.

c'è la consapevolezza della complessità della democrazia e dei suoi processi decisionali, che non possono essere affidati a un capo. Per questo la seconda questione fondamentale della nostra Costituzione è l'equilibrio tra i vari poteri. È l'equilibrio tra i poteri del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica, l'equilibrio tra i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri. Come sapete, il Presidente del Consiglio non ha potere sopra i Ministri e questo modello fu scelto allora ed è peraltro

ma a me interessa relativamente poco, perché se fosse un grande slancio italiano di innovazione, potremmo compatirlo. In fondo, la nostra Costituzione, insieme alla Costituzione tedesca, ha aperto la strada al costituzionalismo in

l'equilibrio dei poteri e l'equilibrio tra le varie articolazioni della Repubblica. noi, dinanzi a questa riforma che appare molto semplice e che viene raccontata ai cittadini italiani in maniera molto semplice, vogliamo semplicemente farvi decidere:

che giustamente è in Aula ad ascoltare questa discussione, tramite lei Presidente - noi andiamo a modificare gli equilibri dei poteri tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Noi avremo un Presidente del Consiglio eletto dal popolo: l'abbiamo sentito risuonare diverse volte qui e lo sentiamo risuonare diverse volte in una propaganda da cui - mi permetto di dire - dovrebbe essere preservata la legge fondamentale. La propaganda non dovrebbe usare la Costituzione o le riforme costituzionali; sarebbe un buon costume che la tenessimo fuori dalla propaganda di partito. La semplificazione e la propaganda di partito non fanno bene alla Costituzione. Allora dire ai cittadini che conteranno di più che conteranno di più e che non intaccherete i poteri del Presidente del Repubblica è dire una bugia, perché non è così. I cittadini non conteranno di più, perché il potere dei cittadini non si esprime semplicemente nella scelta di un capo, ma si esprime nella scelta della partecipazione, della consapevolezza, della crescita democratica e quindi anche attraverso i partiti, le associazioni, le articolazioni della Repubblica eccetera. La difesa La difesa dei cittadini e dei loro diritti non può essere affidata alla scelta del Presidente del Consiglio, perché altrimenti vorrebbe dire - se questo fosse vero, signora Ministra - che tutte le altre democrazie in giro per il mondo non stanno esercitando una vera democrazia, perché nessuna di loro ha scelto di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio. Quindi, non so cosa vi è saltato in mente, io non riesco a capire cosa vi sia saltato in mente. Qual è il motivo per cui partiamo da lì? da lì? Volete dimostrare che c'è una nuova rifondazione del patto costituzionale? Perché partite da lì? Non si capisce. Si poteva parlare di rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio, che era una cosa non solo legittima, ma auspicabile, secondo me. secondo me. Si è parlato qui di sfiducia costruttiva, si è parlato di potere di revoca dei Ministri eccetera, tutte cose su cui si poteva ragionare, ma l'elezione diretta dice: attenzione, amici cari che verrete a votare, noi abbiamo il Presidente del Consiglio che verrà eletto direttamente da voi e quindi ha una grande legittimazione e avremo un Presidente della Repubblica eletto dalla casta, da quelli che stanno in Parlamento e che, teoricamente, sarebbero i vostri rappresentanti, secondo la Costituzione repubblicana. Però questo Presidente è sostanzialmente il risultato degli accordi tra i partiti, non della scelta dei rappresentanti del popolo, perché questa è la narrazione, su questo contate per vincere il *referendum*. Allora, così facendo, la conseguenza ovvia e diretta è che c'è un indebolimento sostanziale, vero e profondo dei poteri del Presidente della Repubblica, perché se c'è un'istituzione rispettata nel mondo, rispettata in Italia, amata dai cittadini e che rappresenta fisicamente, da sempre, la fiducia e quel patto fondamentale che è la Costituzione italiana, se c'è una figura che ha rappresentato sempre un fattore di protezione e di difesa della Costituzione, al di là di ogni Governo che si è succeduto, questa è esattamente la Presidenza della Repubblica.

il susseguirsi di Governi e posso testimoniare che il Presidente della Repubblica ha esercitato un ruolo fondamentale per le istituzioni italiane, molto al di là dei ruoli che potevano esercitare, con tutto il rispetto, i Presidenti del Consiglio che hanno cercato di fare il loro dovere il loro dovere in maniera adeguata. Quindi questa bugia va tolta dal tavolo, perché il Presidente della Repubblica sarà in secondo piano rispetto al Presidente del Consiglio. Se volete fare questa modifica, dovete dire la verità ai cittadini, perché devono sapere la verità:

e anche al potere di difesa delle istituzioni che il Presidente della Repubblica ha sempre egregiamente esercitato durante gli anni della vita repubblicana. Vorrei concludere, visto che abbiamo la Ministra in Aula. Tutte queste considerazioni potrebbero Aula. Tutte queste considerazioni potrebbero essere derubricate al fatto di fare della filosofia o del patriottismo costituzionale a buon mercato. Sarà così vero che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio darà stabilità ai Governi? Sarà così vero, signora Ministra? Penso che invece proprio lei dovrebbe sapere - e le leggo la scheda - che che abbiamo avuto un Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana che si chiamava Silvio Berlusconi, che si è presentato ai cittadini. Nessuno lo ha votato direttamente. Lei ha votato direttamente per Silvio Berlusconi? Io no sicuro, ma neanche lei. Lei ha votato invece per il partito di Silvio Berlusconi.

No, il suo partito aveva preso la maggioranza e Silvio Berlusconi ha governato la Repubblica senza bisogno di essere eletto direttamente dal popolo. Allora questa operazione non è un'operazione tecnica, perché non è vero che gli italiani non hanno potuto scegliere Berlusconi o Prodi, e non è vero che non hanno scelto Giorgia Meloni; l'hanno scelta. A meno che voi non diciate che il Presidente della Repubblica vuole fare cose contro la democrazia sostanziale dei cittadini. Se voi assumete questo principio, allora avete ragione, e cioè c'è un Presidente della Repubblica che è contro la volontà dei cittadini. Invece no: il Presidente della Repubblica rimedia ai pasticci che i partiti di quella maggioranza hanno combinato, rimedia per dare stabilità alle istituzioni, rimedia per dare dei Governi che continuino a governare. Chi ha mandato a casa Silvio Berlusconi nel 2011? Sono state delle trame di potere? No, la situazione economica internazionale e il fatto che non si governavano i processi. Lasciamo perdere, per favore. È stato eletto sempre dal popolo Silvio Berlusconi, così come Romano Prodi e anche Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Se è così, che bisogno avevate di tutta questa roba? Perché non mettersi a sedere per ragionare sul rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio? Perché non mettersi a sedere e ragionare degli equilibri dei poteri e di un Parlamento che venisse deciso direttamente dai cittadini con una forma di legge elettorale, intanto che si preparava anche la riforma? Se lei, signora Ministra, non è convinta di quello che ho detto, si vede che ha memoria cattiva, mi spiace. Ripeto, lei mi spiace. Ripeto, lei non ha votato per Silvio Berlusconi, eppure Silvio Berlusconi ha fatto il Presidente del Consiglio. Il motivo per cui è caduto non è stato perché non era chiara l'indicazione, ma perché la sua maggioranza è mancata. Questa legge impedirà questa cosa? La risposta è no, perché, se questa maggioranza si sfalda, che Giorgia Meloni venga eletta direttamente dal popolo o non venga eletta direttamente dal popolo, il Governo va a casa. Questo è il punto. Quindi non si capisce, o forse si capisce troppo bene, cosa state cercando di fare. State cercando di modificare l'unità sostanziale della Costituzione e l'equilibrio dei poteri e di diminuire i poteri del Presidente della Repubblica, cosa che noi non vogliamo e non possiamo permettervi.

continuare il discorso appena fatto dal senatore Delrio. Noi oggi siamo qui per una riforma che sicuramente non è voluta dal popolo. Non ho mai sentito, nei vari presidi che hanno riempito le nostre piazze,

dei giochi da tavolo, sembra chiuso nelle sue stanze e si discosta da quelle che sono le vere necessità degli italiani. Gli italiani chiedono ben altro.

diritto ad avere una vita salubre in un ambiente sano, il diritto ad avere infrastrutture. Tutto questo viene inficiato da lavori parlamentari che invece si occupano di giochi da tavolo, si occupano di dimostrare quanto si è bravi a giocare ai Padri costituenti. Siamo molto lontani dall'essere in grado di difendere la nostra Costituzione e dal portare davvero qualcosa di utile ai nostri cittadini e alla nostra Italia. Questo è un gioco di bandiere: il premierato contro l'autonomia differenziata. Vanno di pari passo, devono arrivare di corsa. Qui stiamo facendo esercizio di oratoria, perché, a quanto già si dice, non ci sarà dato modo di cambiare una virgola di questo disegno di legge. Dunque già oggi i nostri diritti di parlamentari sono quasi aboliti, visto che si va avanti a decreti-legge e visto che questa maggioranza sfrutta sfrutta i suoi numeri per schiacciare completamente la voce delle opposizioni. Se guardiamo bene cosa vorrebbe il popolo, sicuramente vorrebbe eleggere i parlamentari, come il Presidente del Consiglio, ma tra la gente comune, non tra i politici, che nei listini bloccati sono sempre gli stessi. Perché non parliamo di riforma elettorale? Quella sì che è una riforma voluta dai cittadini, perché si vorrebbero sicuramente eliminare i listini bloccati. Allora che facciamo? Il Presidente del Consiglio lo scegliamo sempre tra le stesse persone, sempre tra gli stessi politici? E così anche i senatori a vita. Dove ci porta la modifica costituzionale che stiamo portando avanti? Semplicemente Semplicemente a eliminare la possibilità di dare questo onore ai cittadini meritevoli, invece lo si potrà dare solo agli ex Presidenti della Repubblica; quindi sempre e solo alla politica. Una politica che schiaccia tutto il resto e schiaccia anche queste figure che danno che danno onore e lustro alla nostra Italia. Sinceramente leggendo questo testo, come del resto ultimamente mi capita, mi rendo conto davvero che quello che viene detto è sempre fallato. Il compito delle opposizioni è quindi quello di essere la voce dell'informazione. Questo facciamo in quest'Aula oggi e questo faremo nelle piazze da ora in avanti, perché serve

soltanto un signor sì, in mano al Presidente del Consiglio, quindi un politico che fa parte della maggioranza, che poi sarà in grado di ricattare i suoi parlamentari perché andranno via tutti insieme. *Simul simul*: la sorte del Presidente del Consiglio sarà la sorte dei parlamentari. Quindi quale democrazia? Quale possibilità

questo *diktat*? Il Presidente del Consiglio potrà dire o da questa porta o per la finestra, come si suol dire. Una

legislativo, che dovranno definire i livelli essenziali delle prestazioni, non potremo noi stabilire una linea netta, ma a noi sarà concesso solo fare delle osservazioni per nulla vincolanti. Noi non ci stiamo a tutto questo. Mi appello a tutti i colleghi invitandoli ad essere obiettivi nell'analisi del testo, concreti nel rappresentare fuori quello che si sta facendo ed anche umili nell'accettare i consigli dai tantissimi costituzionalisti che si sono avvicendati in Commissione, che tutti unanimemente hanno rappresentato le difficoltà di questo scellerato disegno di legge che dovrà finire con un *referendum* abrogativo. Questo sì sarà il *boomerang* che arriverà su di voi perché chiaramente la verità viene sempre a galla. Nel limite di quelle che sono ora le vostre esigenze elettorali, riuscirete magari a illudere e

la separazione dei poteri è incostituzionale e gravissimo. Gli organi di garanzia verranno nominati dalla maggioranza che si costituisce e quindi non ci saranno parti terze, cosiddette *super partes*. È necessario che ci sia una regola chiara su quella che sarà la legge elettorale. Noi qui stiamo facendo precisamente come è stato fatto per il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Si dice sì, poi si farà. Quindi si rispetta la Costituzione su qualcosa che non c'è. non sono finanziati e nemmeno quantificati e indicati i livelli essenziali delle prestazioni che renderebbero il disegno di legge costituzionale, e qui non c'è il riferimento alla legge elettorale che andremo a mettere in campo

chiaro. Essere al buio non fa parte del lavoro parlamentare. I cittadini vorrebbero che noi fossimo informati su tutto per essere quindi utili e portare delle risposte portare delle risposte chiare e confacenti a quelle che sono le necessità dell'Italia e degli italiani. Nel terzo comma dell'articolo 92 si esclude in modo esplicito che possano essere Presidenti del Consiglio

non soltanto di controllo e di confronto vero, ma chiaramente può anche essere un luogo in cui il confronto è talmente ricco ricco e variegato che può portare ad un allungamento dei tempi decisionali. Infatti spesso - siamo di meno, tra l'altro, in quest'Aula, rispetto al numero previsto all'inizio dalla nostra Costituzione si sono fatte tutta una serie di riforme, anche quella del Regolamento di questa Assemblea, per accelerare e rendere più efficaci i nostri lavori. Ora, però, quello che ci insegnano quando studiamo la Costituzione e la divisione dei poteri, come raccontiamo spesso anche agli studenti che vengono qui a trovarci, è che esiste questa invenzione della modernità della distinzione dei diversi poteri, per cui c'è il potere del Governo, c'è il potere del legislatore e poi c'è anche il potere di chi effettua il controllo. Sono delle distinzioni che fanno della nostra democrazia certamente un ordine complesso, ma un ordine che ci avvicina alla complessità che è presente nella società. È inutile ricorrere alle scorciatoie come quella di questa riforma,

sia con riferimento alle motivazioni - e spiegherò perché - sia con riferimento alle modalità con cui la proposta di riforma si inserisce nel contesto internazionale. Quando si fa l'analisi comparata - è stato detto prima da un collega della maggioranza - non la si fa perché si vuole scopiazzare, ma perché i sistemi delle democrazie liberali sono sistemi complessi e cercano, con diverso ordine, a seconda delle diverse soluzioni culturali,

facciamo una forzatura, una curvatura nella nostra Costituzione che effettivamente elimina il ruolo significativo del Parlamento, oltre a quello, come dirò, del Presidente della Repubblica. Qui il parlamentare, nel momento in cui

Non è semplicemente un tema di povertà del parlamentare, ma è un tema che ha a che fare con il tipo di mandato che il parlamentare riceve perché il parlamentare nella nostra Costituzione non riceve un mandato che è associato alla vita del Governo, ma riceve un mandato che è associato alla sua capacità di rappresentare il territorio che lo ha votato e gli elettori e quindi una volontà diversa da quella del Governo, che poi si ricongiunge a quella del Governo nel momento in cui si dà la fiducia. fiducia. Questo non significa, come è stato detto, che noi - e quando dico noi non intendo soltanto noi della minoranza, ma tutti i costituzionalisti che sono stati ascoltati, come sa bene il Presidente, nella 1a Commissione, su questo tema - abbiamo una visione del parlamentare opportunista o del parlamentare che non ha una sua autonomia di giudizio e una sua capacità anche di dire no al Governo sapendo che dopo va a casa. Noi abbiamo un'idea per la quale il parlamentare deve poter esercitare la sua libertà, legge in esame viene privato esattamente dello spazio di libertà del mandato parlamentare. Abbiamo anche qualche sospetto. Io sono un semplice parlamentare alla prima legislatura, però, proprio nell'esperienza della 1a Commissione, ho avuto, da parte dei parlamentari di diverse forze politiche di questa maggioranza, una strana esperienza, perché ho avuto dei sussurri nei corridoi da parte di una forza politica che mi incoraggiava a presentare emendamenti contro quando si votava l'autonomia differenziata e dei sussurri contrari da parte di un'altra forza politica, quando si votava il premierato. La forza del Parlamento, l'autonomia dei parlamentari, consiste nel fatto che si parla qui e si parla nelle Commissioni e non si sussurra nei corridoi. Il parlamentare che ha una sua dignità, una sua autonomia non dice "vorrei, ma non posso", ma cerca di esercitare la propria autonomia e la propria libertà. Nel momento in cui si approva una proposta di riforma parlamentare in cui il destino del mandato del Parlamento e del parlamentare è legato al destino del Presidente del Consiglio, noi stiamo completamente cancellando il ruolo dell'autonomia del parlamentare e stiamo rivedendo il rapporto fra libertà, potere e rappresentatività. Un parlamentare eletto deve essere libero di poter dire di no ad un provvedimento, senza che questo comporti a cascata una decisione di scioglimento delle Camere, come è quanto previsto dal disegno di legge in discussione. Allo stesso modo, il Presidente della Repubblica, che esercita la sua libertà costituzionale attraverso la propria discrezionalità, deve essere libero di valutare anche come cambia nel tempo la rappresentatività nel Parlamento e la volontà politica. Allo stesso modo persino il Presidente del Consiglio o la Presidente del Consiglio indicata deve poter avere la libertà di rinunciare, per qualunque ragione, nel corso del suo mandato parlamentare a quel mandato ed esercitare questa libertà senza per questo pensare che si porta a casa tutto il Parlamento e tutti i parlamentari. In sostanza, quello in esame è un disegno di legge che mette insieme cose diverse che, dal punto di vista della razionalità politico-istituzionale, non dovrebbero necessariamente stare insieme, perché se si cerca la rappresentatività, allora si punta all'idea che il cittadino deve poter scegliere il Presidente del Consiglio che lo governa, ma si mette da parte il tema della stabilità. Se invece si cerca la stabilità, allora si mette da parte il tema della rappresentatività e si punta sulla riforma istituzionale. Se si cerca di evitare quello che avete scritto nella parte di accompagnamento di questo disegno il ribaltone, si insiste, per esempio, come abbiamo sempre sostenuto, con la riforma dei Regolamenti parlamentari, per quello che riguarda la formazione dei Gruppi, introducendo dei disincentivi a questa azione. Il combinato disposto di tutto questo assieme è la cosa fondamentale che non convince. Non è un caso che questo sia l'unico premierato, l'unica ipotesi di legge che non trova nessun tipo di riforma simile in nessuna democrazia Ci sarà un motivo ed è che non si possono mettere superpoteri, non si può mettere un Presidente del Consiglio che deve per forza essere eletto, indicato dai cittadini, per forza ricevere l'incarico e che, se non riceve la fiducia, fa cadere la prospettiva del Governo e si va immediatamente a votare. Non esiste, in questo impianto di potere già così forte, che si inserisca una legge elettorale a maggioranza e non esiste neanche il fatto che non ci sia una libertà di via d'uscita, perché se c'è una via d'uscita del Presidente poi si deve andare ad elezioni, tranne che nel caso di morte. Questa legge così forte e così abnorme, così inutilmente e pericolosamente accentratrice dei poteri su un unico partito, su un'unica coalizione, su un'unica persona, a questa opposizione potrebbe anche convenire. Noi siamo convinti, infatti, signora Ministro, che sul prossimo Governo vinceremo noi. Nonostante questo, noi respingiamo questa ipotesi, perché ci rendiamo conto che chiedere ai cittadini un *referendum* su una persona, rendendo i parlamentari meri esecutori di una volontà non meglio definita, così come il Presidente della Repubblica, privato di quelle che sono le sue prerogative costituzionali, crea un disegno complessivo di architettura istituzionale che è veramente preoccupante. Mi ricorda un discorso, fatto tanti decenni fa, da una persona che disse alla Camera: io avrei potuto comunque fare un Governo senza senza passare dalle Camere, ma non l'ho fatto e quindi ringraziatemi per il fatto che sono qui, chiedendo comunque il sostegno ai miei parlamentari. Ovviamente era una fase storica diversa, una fase che noi abbiamo cancellato, ma vi assomiglia nell'idea del potere, della personalizzazione del potere, dell'autonomia degli eletti e della loro libertà. Un altro tema che viene fuori da questa discussione è quello delle implicazioni dei rapporti istituzionali internazionali. Noi leghiamo la rappresentatività di questo Paese non più al Parlamento come luogo di autonomia, ma ad una sola persona. Questo non è soltanto un tema di per sé pericoloso, ma è un tema che può anche cambiare la postura della politica, la postura della nostra capacità di confronto. Noi oggi viviamo in un mondo fortemente polarizzato, fortemente personalizzato, e non è affatto garantito che una personalizzazione ulteriore, che abbia nelle istituzioni un sistema sbilanciato di poteri e rappresentatività, possa migliorare le condizioni o ridurre determinati pericoli. In conclusione, questa proposta è una proposta che non ha una sua razionalità, non ha una razionalità politica, non ha una coerenza istituzionale. Per la prima volta riduce in modo fortemente drastico il ruolo del singolo parlamentare, la sua libertà, la sua discrezionalità. Riduce la discrezionalità, il potere e la rappresentatività del Presidente della Repubblica. Affida a chi ha vinto le elezioni il compito di essere non il sindaco d'Italia, ma il padrone dell'Italia ed è in aperta violazione con quello che i Padri costituenti hanno scritto. Visto che spesso si fa riferimento, da quella parte lì, al concetto di Patria, ricordate che il concetto di Patria significa terra dei padri. Questa proposta di legge non ha nulla a che fare con i nostri Padri costituzionali. È un disegno di legge orfano e, soprattutto, è orfano

partiamo da una situazione in cui il ruolo di una Repubblica parlamentare come la nostra è ridotto ai minimi termini. Noi siamo ormai dei notai. Voi quasi ci quasi ci riservate almeno questo compito di ratificare le scelte del Governo. Quindi, già c'è un organo collegiale che decide, che si è appropriato del potere legislativo e legifera in nome per conto del Parlamento. Ormai è una prassi, che si è consolidata sempre di più con l'attuale Governo.

ai cacicchi del proprio partito per cercare poi di diventare innanzi tutto il *leader* di quella coalizione ed essere eletto. Capite quindi la pericolosità di questa riforma,

che magari avevano causato danni di tipo bellico e autoritario, un po' come sta facendo oggi il Governo Netanyahu in Israele, che causa migliaia di morti fra bambini, civili e innocenti;

venivano da diverse sensibilità. Proprio il lavoro di intelligenza collettiva aveva portato questo risultato straordinario, una Costituzione bellissima, che ci ha dato libertà e democrazia. Siamo un Paese libero e democratico grazie alla nostra Costituzione, che volete rendere sempre

quindi spero che questa riforma non passi e che non abbiate i numeri per farla passare, perché è veramente pericolosa, come ci insegna la storia: un uomo solo al potere mi ricorda i tempi che furono ed è sicuramente anacronistico un uomo forte al potere, magari che grida dal balcone, e un po' come il Piano Mattei mi ricorda le campagne in Africa; mi ricorda questo passato di una novantina di anni fa, che è un po' preoccupante. Noi dovremmo invece capire che i nostri difetti e i nostri problemi secondo me sono altri. Innanzi tutto, secondo me dovremmo imporre programmi elettorali

con un *click* sarebbero costati 20 miliardi al mese. Questo è quello che proponete, la spesa improduttiva: oggi criticate il superbonus e volevate 1.000 euro con un *click*. Queste cose ve le dovete ricordare: magari quei 1.000 euro con un *click* un po' di voti ve li hanno portati, perché sull'onda della disperazione della pandemia, qualcuno vi ha creduto e poi vi ha votato. Noi dovremmo fare altro, secondo me: dovremmo fare programmi elettorali che siano supportati da numeri, quindi dovremmo imporci che ogni forza politica abbia un programma elettorale che dica dove prende i soldi quando promette qualcosa. Lì saremmo già più credibili.

più di mille disegni di legge, questa è intelligenza collettiva; dobbiamo fare un lavoro in cui il Parlamento riprenda il ruolo legislativo e si veda all'interno delle nostre proposte di legge quali siano le migliori idee e le migliori soluzioni per risolvere i problemi che attanagliano oggi il nostro Paese, ma soprattutto quelli che mettono a rischio il futuro dei giovani. Dovremmo quindi lavorare su questo, su questo, valorizzare quello che abbiamo prodotto: abbiamo migliaia di disegni di legge depositati e non perdiamo il tempo - che sarebbe tempo utile - per discuterne e vedere cosa c'è di buono, ma poi stiamo magari mesi a discutere una riforma costituzionale autoritaria, che mina il futuro democratico di questo Paese. Questo è un ruolo del Parlamento assolutamente sbagliato. Noi stiamo solo perdendo del tempo, quando abbiamo tanti disegni di legge utili che oggi potremmo discutere, però c'è l'arroganza di un Governo che pretende di sapere tutto e di voler decidere tutto. Poi abbiamo visto le decisioni; voi criticate una misura che ha fatto rilanciare l'economia e oggi vi accorgete che quella misura è insostenibile, ma il ministro Giorgetti la gestisce da tre anni e mezzo.

Questo chi lo doveva fare? Lo dovevamo fare noi, che non abbiamo responsabilità di Governo, o voi? Oggi state cambiando le leggi in essere, facendo passare i crediti da cinque a Questo è assolutamente anticostituzionale e antidemocratico. Abbiamo fatto delle leggi e oggi state agendo in maniera retroattiva. Vi rendete conto dei disastri che state combinando a questo Paese? *(Applausi)*.

chi doveva monitorare il superbonus? Il Ministro. Chi doveva fare degli scenari costi-benefici? Il Ministro. E oggi scopre che la manovra è insostenibile e ce lo dice quando ormai dall'insediamento del Governo Meloni, quando il superbonus pesava 50 miliardi, oggi è arrivato a 120 miliardi; 70 miliardi sono stati scatenati dal panico di Giorgetti, dove tutte le imprese per finire hanno accelerato i lavori, quando quella misura doveva essere resa strutturale con un *décalage*. La misura del 110 per cento era infatti pensata per la pandemia, ma finita la pandemia doveva passare al 90

per un periodo limitato per riuscire ad avere quel salto nel nostro PIL che c'è stato. Però, poi, è logico che quella misura andava resa strutturale. Questi sono gli uomini forti al potere che stanno distruggendo il Paese. I risultati sono questi perché voi non leggete le nostre proposte, non usate l'intelligenza collettiva, ma lavorate in maniera saccente e arrogante. Pensate di essere competenti in ogni materia, ma così non è. La vera forza, quella da cui poi il MoVimento 5 Stelle è nato, è la forza collettiva. Ha un ruolo fondamentale, perché noi pensiamo che il confronto ci arricchisca, non l'uomo forte dal balcone che urla «mille euro con un *click*», o la donna in questo caso. Fatevi Fatevi un esame di coscienza, capite che fino adesso state facendo un errore dietro l'altro, state accumulando solo sbagli e purtroppo questi sbagli non li pagherete voi, perché se fosse stato così, si dice che ognuno è causa del suo male, ma li pagheranno quei li pagheranno quei ragazzi che oggi studiano e assistono a questo disastro. Tornate indietro e prendete esempio dai nostri Padri costituenti, le cui sensibilità hanno realizzato una Costituzione bellissima. Noi non ci sentiamo inclusi in questo progetto. State cambiando le regole del gioco da soli in maniera univoca. Siete voi a decidere il destino, il futuro e le regole del gioco di tutti. Questo è

rappresentanti del Governo, permettetemi di affermare che la nostra Costituzione è l'affresco principe della nostra democrazia. È il capolavoro della politica italiana su cui è rinata l'Italia dopo anni bui di regime e di guerra. In un certo senso, è la Cappella Sistina della Repubblica, su cui sono impressi con parole chiare, semplici ed incisive i princìpi fondanti del nostro Stato di diritto, valori universalmente riconosciuti e regole democratiche con cui le nostre Madri e i nostri Padri costituenti hanno dipinto il ritratto di quella che sarebbe diventata una delle democrazie più avanzate al mondo. E lo hanno fatto con una visione a lungo termine che non si basava su umori o opportunità del momento o sulle percentuali di questo o quel partito *leader*, ma con la consapevolezza che chi doveva uscirne vincitore era lo Stato *(Applausi)*, nel suo insieme di istituzioni e cittadini. La nostra Costituzione è nata attraverso una discussione che ha coinvolto tutto l'arco costituzionale, perché la democrazia è confronto, mediazione, condivisione in particolare dei pilastri chiamati a reggere tutto l'impianto democratico, che fino ad oggi non ha mostrato crepe proprio grazie al modo con cui la Costituzione italiana è stata studiata e approvata. Oggi invece si propone di cambiare quello stesso impianto senza che vi sia stato alcun confronto preventivo e condiviso, auspicabile, anzi essenziale, per una modifica così incisiva e stravolgente dal nostro sistema politico e istituzionale. Signora Presidente, noi siamo qui in quest'Aula chiamati a rappresentare il popolo italiano e a garantire che le differenti visioni della società e della politica siano considerate, rispettate e soddisfatte. Quale momento più alto di una modifica costituzionale richiederebbe il confronto e la sintesi fra noi eletti? Su cosa dobbiamo ragionare di comune accordo se non sulle modifiche costituzionali di quella Carta che è la garanzia reale e duratura della Repubblica italiana? Dovremmo essere chiamati a una condivisione dei princìpi di riforma per mantenere intatto quel ritratto di democrazia realizzato nella Costituzione con pennellate semplici ma cariche di valore, senza dover far ricorso a contorsioni linguistiche. I 139 articoli della Costituzione non lasciano spazio a dubbi e, conservando i propri colori freschi e vivaci dopo quasi ottant'anni di di età, sono ancora attuali oggi come lo erano ieri. Ad esempio, l'articolo 94, quello che racchiude l'essenza del rapporto fra Governo e Parlamento, ovvero l'esercizio del voto di fiducia, è composto da sole 88 parole. Fra l'altro, che questo sistema di fiducia funzioni bene il Governo lo sa molto bene, visto che nel corso di questa legislatura ne ha fatto abbondante ricorso *(Applausi)*, bloccando di fatto il lavoro legislativo di competenza delle Camere. torniamo all'articolo 94: 88 parole nella sua stesura attuale. Questo articolo, con le modifiche che il Governo e i Gruppi di maggioranza ci propongono, passerebbe da 88 a ben 246 parole, quasi il triplo. Potrebbe sembrare una banalità, ma non è così, perché è nella chiarezza del tratto delle parole e del linguaggio che viene definita la trasparenza di una legge, di un articolo, di un comma. E da questa trasparenza ne deriva forza e quella genuinità legislativa che portò il capo dello Stato provvisorio Enrico De Nicola ad affermare: «Possiamo firmare con sicura coscienza». Si riferiva proprio alla nostra Costituzione. Signora Presidente, questa frase dell'allora Capo dello Stato, che non a caso è utilizzata sui canali di comunicazione ufficiale del Senato della Repubblica, deve far riflettere, oggi più che mai. Il gioco democratico fu studiato perché ci fossero pesi e contrappesi, perché la Repubblica avesse nel suo DNA gli elementi per risolvere i conflitti interni fra organi dello Stato e soprattutto perché ci fosse quel bilanciamento necessario fra le attività del Governo e del Parlamento che vede nel Presidente della Repubblica il massimo punto di equilibrio, e vorrei sottolineare la parola equilibrio. Le Madri e i Padri costituenti, che pur venivano da partiti ed esperienze diverse, mai hanno immaginato uno Stato in cui ci fosse una concentrazione di potere maggiore in una delle sue componenti, ben consapevoli che per storia, tradizione, cultura ed esperienza era l'equilibrio l'essenza democratica che avrebbe garantito il futuro della Repubblica. La modifica dell'articolo 94 della Costituzione introdurrebbe una rigidità eccessiva nei rapporti fra Parlamento e Governo, attraverso automatismi procedurali che inciderebbero sul vincolo fiduciario e concentrerebbero i poteri nelle mani del Presidente del Consiglio, in nome della stabilità di Governo. Ma la stabilità va ricercata nelle alleanze basate su una condivisione della visione del Paese, sulle strategie da adottare perché il Governo e il Parlamento lavorino sugli stessi obiettivi. Non si può sacrificare la pluralità della nostra cultura politica per una stabilità che null'altro sarebbe che la concentrazione di un potere eccessivo nelle mani di una donna o di un uomo impegnati probabilmente più alla ricerca di consensi *social* che ad operare per il bene comune, cose che purtroppo troppo spesso sono in contrapposizione e non collimano. Noi, signora Presidente, ci opponiamo a questa visione *social* delle istituzioni. La responsabilità della politica non è quella di navigare le onde degli umori popolari, ma è quella di riuscire, nella tempesta, a tenere la barra dritta verso quelli che sono gli obiettivi a lungo termine; obiettivi da raggiungere basandosi su analisi reali delle opportunità, dei doveri e degli accordi internazionali, non su *like* e*follower*, perché il Paese deve contare su una guida forte nelle idee e nei progetti, a prescindere da chi in quel momento sia a capo del Governo. È questa la stabilità che dobbiamo ricercare, non quella effimera di numeri basati su seggi distribuiti, più che sul consenso elettorale, su degli artifizi matematici messi in essere per premiare una persona, alimentando un alto rischio di plebiscitarismo. L'elezione diretta del *Premier* potrebbe, anzi può trasformare le elezioni in un plebiscito, focalizzando l'attenzione solo sul *leader* e non sui partiti o sulle questioni politiche. Lo stesso Gianni Letta, non certo esponente di opposizione, ci ha messo in guardia, sottolineando come questa modifica costituzionale ridurrebbe i poteri del Presidente della Repubblica. Fra i tanti motivi, vi è anche quello della legittimità che deriva dall'investitura popolare, che è certamente maggiore di quella che deriva dall'investitura del Parlamento. Ciò porterebbe squilibri in quella che è oggi la dialettica istituzionale, senza fra l'altro risolvere l'annoso problema della scarsa partecipazione alle elezioni; una disaffezione al voto, quella del popolo italiano, che purtroppo raggiungere livelli sempre più alti. Un eventuale *bonus* di maggioranza potrebbe quindi essere assegnato a chi in realtà rappresenterebbe una piccola minoranza degli aventi diritto al voto. Altro che stabilità politica. L'approvazione di questa proposta del premierato equivarrebbe al lancio di un secchio di vernice sul capolavoro del Giudizio universale di Michelangelo. Sarebbe la vandalizzazione della Cappella Sistina. Ecco perché, signora Presidente - mi avvio a concludere - il mio invito è di accantonare questa riforma dannosa e vandalica per il Paese e di avviare un confronto *bipartisan* che parta dall'esigenza di coinvolgere un numero maggiore di cittadini nelle scelte relative alle riforme istituzionali. Solo dopo sarà possibile esplorare cambiamenti alle regole, in modo che garantiscano non la stabilità di un Governo, non la carica di un *leader*, non la maggioranza di un partito, ma lo Stato, le istituzioni e i cittadini. Tramite lei, signora Presidente, mi appello ai partiti di maggioranza. Fermatevi: siamo ancora in tempo per avviare una nuova Costituente dove tutti insieme - così come disse il presidente De Nicola - potremo poi votare eventuali cambiamenti con sicura coscienza. Grazie. colleghi, siamo qui oggi per discutere ampiamente di una legge che rivoluzionerà nei fatti l'ordinamento democratico di questo Paese. Eppure, a parte numerosi colleghi

il parere delle minoranze: un numero stratosferico di otto parlamentari. Devo dire che l'attenzione per un momento così cruciale della nostra democrazia è sconvolgente. Oltretutto vediamo che ci sono solo parlamentari di Fratelli d'Italia, quasi come se le altre forze di maggioranza volessero sfilarsi dalla riforma. Chissà come mai non sono qui a difenderla insieme ai colleghi. Tornando al merito di questa legge, partiamo dalla bugia più grande che avete raccontato in questi mesi ai cittadini italiani, ossia che in alcun modo questa riforma andava ad investire i poteri del Presidente della Repubblica. Basta guardare la relazione che accompagna in Aula il provvedimento per leggere, per leggere, partendo dall'articolo 1, che si abroga il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, ossia la previsione in base alla quale il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita. E la prima prerogativa se ne è andata. Passiamo all'articolo successivo e arriviamo all'abbassamento del *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica. Al primo comma primo comma dell'articolo 88 si sopprime la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due Camere. E un'altra prerogativa esce dalla finestra. Passando poi all'articolo successivo, vediamo che gli atti del Presidente della Repubblica vengono controfirmati dai Ministri proponenti

intellegibili. Andiamo avanti e vediamo ancora che il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo al Presidente eletto e, quindi, un incarico *pro forma*, perché non lo nomina più lui dopo le consultazioni, attraverso una valutazione personale in base a quello che dicono le forze politiche, ma fa quanto gli è stato confezionato dai partiti che hanno ottenuto la maggioranza alle elezioni. Ricordo che ciò non vuol dire che rappresentino necessariamente la maggioranza del Paese, esattamente come avviene ora con questo Parlamento. Praticamente avete già iniziato la campagna pubblicitaria di questo disegno di legge con delle bugie vere e proprie. *(Applausi)*. Archiviamo poi la questione che non toccate i poteri del Presidente della Repubblica perché abbiamo visto che

La nostra Repubblica si fonda su tre poteri - legislativo, esecutivo e giudiziario - che tra di loro devono essere indipendenti e bilanciati, ma con questa riforma l'indipendenza non c'è più. Ci giochiamo anche il ruolo di arbitro del Presidente della Repubblica, come abbiamo visto poc'anzi, perché egli non ha più il potere di sciogliere le Camere laddove manchi una maggioranza. Automaticamente, se non c'è più una maggioranza che

senza un battito di ciglia, senza minimamente preoccuparvi di quello che state facendo al nostro ordinamento e alla democrazia. Non vi rendete conto o ritenete superfluo che vi state auto relegando e state relegando tutti i parlamentari, anche quelli che si oppongono a questa scellerata riforma, al mero ruolo di correttori di bozze, che più o meno è quello che fate già adesso. Già oggi, infatti, se andiamo a guardare i grandi interventi migliorativi o correttivi approvati con i decreti e i disegni di legge che arrivano dal Governo, vediamo che vengono accolti emendamenti *pro forma* che cambiano una virgola, un aggettivo, un articolo, ma nulla di sostanziale. Sono mesi che non vediamo approvare nulla di sostanziale che arrivi dall'iniziativa parlamentare e questo accade una democrazia che si regge sul potere del Parlamento, con le fiducie che vengono approvate e senza un Presidente del Consiglio eletto. Ma un domani che cosa pensate di fare più che gli schiaccia bottoni? bottoni? Questo è quello che state decidendo. O non ve ne rendete conto o non ve ne frega niente, perché tanto a voi interessa solo che ci sia qualcuno a tutelare gli interessi che vi portano qua, null'altro. Eppure, è evidente che già oggi non rappresentate la maggioranza dei cittadini italiani e avete costruito una legge per cui ci sarà una persona che comanda indipendentemente dal fatto che rappresenti o meno la maggioranza, essendo

rappresenta il 43 per cento dei votanti. Non siete la maggioranza neanche oggi. Solo per effetto di una legge elettorale avete la maggioranza in questo Parlamento, perché più del 50 per cento ha votato per qualcun altro. Il 40 per cento degli aventi diritto non è neanche andato a votare. Se facciamo i conti, in realtà voi rappresentate meno del 30 per cento degli aventi diritto e pensate di mettere mano a quella

si possano ricordare, dopo una dittatura che ci ha portato alla guerra e ha portato alla guerra civile il nostro Paese. E voi volete ripercorrere quei passi e riportarci nelle stesse condizioni. Siete degli sciocchi che non si rendono conto

Mi scuso per il termine, e mi rivolgo a lei, Presidente. Penso che chiunque abbia partorito questa riforma non si renda conto dei danni che farà al Paese e l'ha fatto con scarsa capacità di comprendere le conseguenze di quello che stava per fare, oppure con un lucido disegno che ci vuole riportare ai fasti di un ventennio sciagurato, nefasti per i cittadini e brillanti solo per qualcuno che doveva garantire i propri interessi. *(Applausi).* Ripeto che questa riforma è mera merce di scambio: da una parte chi voleva l'autonomia, da una parte chi voleva distruggere il potere giudiziario e dall'altra chi vuole accentrare il potere in una sola persona al comando. Non imparate mai dai vostri errori. Non si impara mai dalla storia, dovremmo tutti studiare di più e non ripetere quegli errori invece di perpetrarli. il progetto che stiamo discutendo in una situazione un po' surreale non è parte di un disegno organico di modernizzazione delle nostre istituzioni; non viene dopo un dibattito vero, profondo, largo nel Paese sul cambiamento dell'architettura istituzionale necessaria per far funzionare meglio le istituzioni e riavvicinare, attraverso questa strada, i cittadini alla politica e alla Repubblica. No, noi non stiamo discutendo di questo tipo di progetto. Il progetto di cui stiamo parlando è un pezzo di un accordo politico sottoscritto sulla testa degli italiani; un accordo di potere per consentire ad ogni forza di questa maggioranza

ad un mese dalle prossime elezioni europee e amministrative. Parlo di bandiere perché questo Governo ha smesso da tempo di occuparsi dei problemi concreti degli italiani, ossia dell'inflazione, del lavoro, delle famiglie delle famiglie che guardano con preoccupazione al loro futuro. Avete smesso di occuparvi di questi problemi e lo abbiamo visto poche settimane fa, quando avete consegnato al Parlamento un Documento di economia e finanza solo tendenziale, che ci racconta come vanno le cose per l'economia e i conti pubblici, ma non ci dice nulla di quello che avete intenzione di fare, non indica priorità per le politiche economiche e sociali. Questo Governo, che sin dall'inizio si è definito politico e di legislatura, non ha una politica economica e non ha una politica sociale. E questo Governo e questa maggioranza hanno deciso di parlare di altro di altro e di ingaggiare, con l'opposizione ma soprattutto con il Paese, una guerra di simboli, di bandiere identitarie, di provvedimenti che servono a scaldare i propri tifosi,

Paese. L'autonomia differenziata è, quindi, la bandiera della Lega. La separazione delle carriere dei magistrati è la bandiera di Forza Italia. E la bandiera di Fratelli d'Italia, che è l'azionista di riferimento di quest'avventura, è l'elezione diretta del *Premier*. è una strada - ricordiamolo in quest'Aula - radicalmente diversa rispetto a quanto avevate proposto agli elettori il 25 settembre 2022, quando nel programma della destra si parlava di elezione diretta del Presidente della Repubblica, e non del Presidente del Consiglio. Se questo patto di potere arriverà a compimento - noi speriamo di no e faremo di tutto perché non accada - provocherà danni gravi e irreversibili agli equilibri istituzionali del Paese e incrinerà in modo irreparabile un'architettura costituzionale che ha retto, nel bene e nel male, per settantasei anni, garantendo a questo Paese democrazia, libertà, equilibrio tra le istituzioni e un ruolo centrale al Parlamento della Repubblica. l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che è il cuore di questo progetto, è una soluzione assolutamente sbagliata per un problema reale. reale. Questa architettura istituzionale che abbiamo ereditato dalla Costituzione del 1948 ha avuto un limite oggettivo sul versante della stabilità dei Governi ed esiste senza dubbio un problema di stabilità degli Esecutivi in un Paese in cui in media i Governi durano meno di un anno e mezzo. Nessuno lo può negare noi certamente non negheremo questo problema. Tuttavia, questo progetto ci porta in una direzione sbagliata; propone una soluzione sbagliata per un problema reale e propone una soluzione che nessun Paese al mondo oggi ha adottato. O meglio, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio - come hanno ricordato tanti colleghi - è stata adottata dallo Stato di Israele con la riforma approvata dalla Knesset nel marzo del 1992, è entrata in vigore con le elezioni del maggio 1996 e abolita subito, dopo cinque anni, abbandonata nel marzo del 2001. Se voi andate nello Stato di Israele, non troverete una persona che rimpiange l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che lo Stato di Israele adottò nel 1992. E non troverete un costituzionalista, a livello mondiale, nelle altre grandi democrazie che proponga questa scelta di riforma dell'architettura istituzionale. Colleghi e colleghe, l'esperienza israeliana

è destinata a non funzionare ed è destinata a portarci su un binario morto. Questa riforma non funzionerà perché parte da un presupposto falso, e cioè l'investitura popolare diretta del Presidente del Consiglio che - lo ripeto - non è prevista in nessuna democrazia al mondo. Secondo questa riforma, l'elezione diretta dovrebbe garantire la stabilità e la governabilità, in realtà, è una soluzione che aggraverà gli squilibri e le disfunzioni del nostro sistema istituzionale. Le radici della crisi delle istituzioni repubblicane, del problema dell'instabilità dei Governi, sono innanzitutto politiche; sono radici legate alla crisi dei partiti, legate alla fragilità e alla conflittualità delle maggioranze che, di volta in volta, si sono susseguite in questo Paese. Sono radici legate alla degenerazione di un sistema, a fenomeni involutivi di che si presentano di fronte agli elettori cerca di conquistare il consenso con proposte demagogiche e irrealizzabili; attori che propongono una classe dirigente di bassa qualità, selezionata per la fedeltà nei confronti dei capi di turno più che per il merito. Questi fenomeni degenerativi portano all'instabilità e a Governi che franano di fronte alla realtà, che non sono in condizione di mantenere le promesse dei demagoghi e dei populisti e che saltano per aria, per poi dare vita a quell'instabilità che ha segnato gli ultimi decenni. Il risultato di questi fenomeni degenerativi, che ripeto essere legati ad una crisi politica più che istituzionale, è sotto gli occhi di tutti. Gli italiani vanno sempre meno a votare. L'astensionismo cresce in modo dilagante negli ultimi anni e non sarà certo questa riforma, la scorciatoia che ci state proponendo, a recuperare la disaffezione dell'elettorato, che è il problema numero uno Questa riforma non funzionerà, signor Presidente, perché l'elezione diretta del Capo del Governo introduce una personalizzazione senza precedenti della *leadership* istituzionale: un uomo o una donna soli al comando. Questa personalizzazione esasperata non è compatibile col sistema disegnato dai nostri Padri costituenti; non è compatibile con un sistema di tipo di tipo parlamentare come quello delineato dalla Costituzione del 1948. E questa personalizzazione ci porta dritti verso una deriva plebiscitaria, che noi dobbiamo evitare a tutti i costi in un Paese con una democrazia fragile come il nostro. Questa riforma, signor Presidente, non funziona, perché prevede l'elezione diretta del Capo del Governo ed un sistema elettorale previsto in forma maggioritaria nella Carta costituzionale, ma con una legge elettorale che tuttora affida alla *leadership* dei partiti la selezione degli eletti, in tal modo privando gli elettori del diritto di scegliere le donne e gli uomini da mandare in Parlamento. Questo combinato disposto porta a un radicale svuotamento della funzione del Parlamento, ancor di più se pensiamo all'assenza di pesi e contrappesi che caratterizza altri sistemi. Penso, tipicamente, al modello degli Stati Uniti d'America, che elegge direttamente il Presidente, ci sono una rigorosa separazione dei poteri e un ruolo altrettanto forte del Congresso. Nulla di tutto questo è la risultante di questa riforma, signor tutto questo finisce per indebolire drammaticamente il principio di rappresentanza e i diritti delle minoranze. Questa riforma non funzionerà se passerà, perché attraverso un meccanismo rigido, rigidissimo, di formazione del Governo si indebolisce il ruolo di garanzia e di mediazione del Presidente della Repubblica, che ha aiutato enormemente il Paese a superare momenti particolarmente difficili e ha risolto crisi alle quali i partiti non sapevano dare risposta. Ridurre il Presidente a un ruolo decorativo - questa è la risultante di tale riforma - è una regressione democratica inaccettabile e pericolosa. La riforma non funzionerà anche per il meccanismo bislacco e barocco - scegliete voi l'aggettivo - che avete introdotto nel caso di dimissioni del Presidente eletto dai cittadini con il meccanismo di subentro che - i costituzionalisti me lo confermeranno - non credo abbia soluzioni paragonabili in nessun altro Paese del mondo. Ed è comunque la premessa per il logoramento del Presidente plebiscitariamente eletto dai cittadini ad opera dei membri della sua stessa maggioranza. *(Richiami del Presidente).* Ho concluso, signor Presidente. Non vogliamo conservare l'esistente e abbiamo presentato le nostre proposte in Parlamento e nel Paese, guardando alle migliori esperienze europee e alle democrazie che hanno garantito Esecutivi stabili. Abbiamo proposto una razionalizzazione del nostro sistema parlamentare attraverso un meccanismo di sfiducia costruttiva che ha funzionato molto bene nell'esperienza tedesca, garantendo stabilità, ma anche la tutela delle prerogative del Parlamento. Abbiamo proposto l'autoriforma dei partiti, che è un nodo cruciale delle problematiche che investono la democrazia italiana. E ci battiamo per una diversa legge elettorale, che, questa sì, è un nodo estremamente importante della crisi del rapporto tra i cittadini e le cittadine e le istituzioni democratiche. Voi - avete deciso di ignorare queste proposte, di andare dritti per la vostra strada e di adempiere a un patto di potere che avete scritto sulla testa degli italiani: è un grave errore. Troverete il Partito Democratico di traverso. Ci troverete di traverso in Parlamento, ci troverete di traverso nel Paese.

questo: elezione diretta, più premio di maggioranza, più riduzione delle prerogative del Capo dello Stato, più poteri esagerati al *Premier* a discapito del Parlamento, uguale stravolgimento della democrazia parlamentare *(Applausi)*. È questo che succederà. Presidente, equivale a un colpo di grazia che arriva dopo aver ferito più e più volte la nostra democrazia parlamentare. Basti pensare all'esercizio sconsiderato della legge delega della *premier* Meloni, che, modificandolo, ha ridotto il Parlamento a un mero passacarte. Ora questo strapotere viene reso strutturale. Quindi, se prima era possibile chiedere con ragione il rispetto e la tutela della nostra attività parlamentare - inutilmente, tra l'altro - d'ora in poi sarà ancora più inutile farlo, perché questo Governo, con siffatta riforma, sta addirittura la previsione di questa tutela. Avete l'urgenza di arrivare a ridosso delle elezioni europee con qualcosa in mano da sbandierare in campagna elettorale, capace di catturare l'attenzione dell'elettorato e distoglierlo dal pensiero dei problemi reali del Paese, che sono sono sempre lì; problemi che, grazie a una straordinaria capacità comunicativa manipolatoria, nascondete con numeri strampalati, condoni vari e mancette da infilare nel sacco della Befana 2025. Ed è un'urgenza che obiettivamente non aveva e non ha ragione d'essere. avete posto in essere una serie di pasticci nella formulazione del provvedimento, tant'è che la stessa *Premier* - lo ricorderete tutti - aveva sollevato dubbi e perplessità sul contenuto, lasciando spazio alle correzioni. E vediamo queste correzioni: tra le varie, quella che sicuramente mi è piaciuta di più è relativa al premio di maggioranza, ma in realtà non è per niente migliorativa. L'articolo 3, norma cardine della riforma che riscrive l'articolo 92 della Carta, nella sua prima versione prevedeva che la futura legge elettorale avrebbe garantito il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste dei candidati collegati alla o al *Premier*. Questa previsione, lo ricorderete tutti, sollevò per la sua grande arroganza molte critiche, anche perché non specificava alcuna percentuale minima di consenso per far scattare il premio. Questo succedeva a novembre. Dopo qualche mese viene depositato il nuovo testo, che vede scomparire la percentuale dei seggi da assegnare, prevedendo più semplicemente - ma "più semplicemente" è un modo di dire, che evidentemente vale per chi lo ha scritto che la coalizione vincente vedrà garantita una maggioranza in ciascuna Camera, nel rispetto dei principi di rappresentatività, rimandando la definizione specifica della percentuale a una futura legge elettorale. In questo modo, furbescamente, è stato spento lo sconcerto provocato da cento, mantenendo però ferma la vera gravità di questa previsione, ossia la costituzionalizzazione del premio di maggioranza. In questo modo, infatti, si sta costituzionalizzando la trasformazione radicale del rapporto tra Parlamento e Governo. Questa è la vera arroganza, grave e preoccupante, che elimina la separazione dei poteri, che è invece necessaria in una democrazia vera, non apparente. Costituzionalizzando il premio di maggioranza, il Governo in Parlamento avrà una maggioranza ovviamente superiore al 50 per cento, che potrà essere del 52, del 54 o del 55 per cento, ma che in ogni caso darà la possibilità - ma chiamiamolo pure "il potere" - di incidere nelle votazioni in Parlamento. Pensiamo all'incidenza nel far eleggere in Parlamento, ad esempio, quelle figure che la Costituzione definisce organi di garanzia: pensiamo allo stesso Presidente della Repubblica, o ai giudici della Corte costituzionale. signora Presidente, credere che tutti i colleghi della maggioranza abbiano chiare le conseguenze di questa riforma e che con questa consapevolezza le abbiano condivise e supportate. Con rispetto parlando, diamo per scontato che tutti conoscano gli effetti di questo provvedimento, però che in molte parti manca di specifiche, rimandando alla legge elettorale che ancora non esiste. È quindi improbabile che si conoscano tutti gli effetti della riforma, ma già quelli che possiamo dedurre dalla lettura sono comunque gravi e, quindi, preoccupano decisamente e profondamente. Dando quindi per scontata questa conoscenza precisa, possiamo affermare che siamo davanti ad un preciso disegno che mira a ledere i principi fondamentali che stanno alla base dell'equilibrio dei poteri. Tornando all'arroganza di cui sopra, questa si mostra in tutta la sua bellezza, quando supera anche ciò che abbiamo visto fare con il Governo Renzi, che affiancò alla riforma costituzionale una riforma della legge elettorale orientata a supportare la trasformazione istituzionale. Qui si va ben oltre e si è arrivati a mettere nella riforma della Carta delle regole del gioco scritte su misura. Che dire poi della possibilità per gli elettori di far sentire la propria voce? È una possibilità presentata su un bellissimo piatto d'argento, che si rivelerà essere di argento finto. oltre ai rapporti tra poteri, a essere indebolita sarà anche la capacità dell'elettorato di vedere rappresentate le proprie istanze. Si potrà scegliere solo tra opposti *leader* e le loro liste di fedelissimi, concentrando sempre più nelle mani dei primi e sempre meno in quelle della rappresentanza popolare la scelta dei rappresentanti. Altro che stabilità dei Governi, signora Presidente! A questo Governo interessa solo la propria stabilità e occupare velocemente tutto ciò che si può occupare, per rafforzare questa bella stabilità. Alla base di una democrazia vera e sincera, che non prende in giro il proprio Paese, ci dovrebbe essere un'azione legislativa a favore del mantenimento dell'equilibrio dei poteri, ma il Governo sta facendo esattamente il contrario: sta colpendo a morte la nostra democrazia.

piuttosto riduce la partecipazione democratica. Oggi siamo chiamati a decidere su un provvedimento che cambia la natura del Parlamento, un provvedimento che di fatto ne esautora il potere. Siamo chiamati quindi a difendere l'organo pilastro nella nostra Costituzione, che viene invece svilito sia dall'autonomia differenziata, che dal premierato. Si passerà dalla primazia del Parlamento alla primazia del Governo: è un cambiamento radicale del modello di democrazia che determina una concentrazione del potere che non ha eguali, consegnando alla maggioranza anche la possibilità di eleggere il Presidente della Repubblica. Abbiamo più volte evidenziato, come d'altra parte ha fatto anche parte della maggioranza, la necessità di conoscere ed esaminare insieme la legge elettorale per fugare i dubbi di illegittimità che abbiamo e che temiamo, ma la ministra Casellati ci ha detto che scopriremo la legge elettorale solo dopo aver votato il premierato, una dichiarazione poco rispettosa del nostro ruolo e del nostro lavoro. Con la Carta del 1948, i nostri Costituenti intesero costruire, dopo l'esperienza autoritaria, una democrazia a impianto pluralista garantista, ritenendo che questa forma di governo fosse la più adatta a favorire la convivenza pacifica e lo scambio tra le diverse forze in campo che si contrapponevano e che erano espressione di un sistema politico caratterizzato da un livello molto elevato di frammentazione e conflittualità. È chiaro che ancora oggi il nostro sistema politico appare caratterizzato da diverse forze in campo che dovrebbero dialogare in un'ottica di scambio e compromesso politico. Con questa riforma viene irresponsabilmente spezzato l'equilibrio tra la funzione di indirizzo politico e la funzione di controllo costituzionale, attraverso la riduzione dei poteri sia del Parlamento che del Capo dello Stato. Si affianca ad un Capo dello Stato, rappresentante dell'unità nazionale, ma eletto in secondo grado dal Parlamento, un Presidente del Consiglio, rappresentante della maggioranza, ma eletto in primo grado direttamente dal popolo e, di fatto, investito di una legittimazione e di un peso costituzionale costituzionale superiore a quello riconosciuto al Capo dello Stato. Si tenta di creare una forma di governo che non ha precedenti e che mira a combinare elementi non combinabili del governo presidenziale con elementi del governo parlamentare, sottraendo però la loro impostazione impostazione originaria voluta dai Padri costituenti, dal momento che al governo parlamentare si sottrae il valore sostanziale della fiducia e al governo presidenziale si sottrae il limite insuperabile espresso dalla divisione dei poteri, introducendo un vincolo di dipendenza, sin dalla fase costitutiva, del potere legislativo dal potere esecutivo. Il Partito Democratico si oppone con fermezza a questo tentativo di attentato alla democrazia del nostro Paese, democrazia che non è la libertà di acclamare un capo, ma la libertà di scegliere di essere rappresentato in un sistema di pesi e contrappesi che non permetta al singolo, singolo, all'uomo o donna al potere, di stravolgere l'assetto istituzionale. Non riteniamo di poter trovare in questa riforma possibili linee di compromesso, che invece, con buona volontà, sarebbe possibile raggiungere, ove si volessero implementare strumenti costituzionali già sperimentati efficacemente in altri Paesi, in grado di perseguire con minori rischi, rispetto a quelli che questo disegno prospetta, quegli stessi obiettivi di rafforzamento della stabilità dei Governi che con questa riforma si dichiara di voler perseguire. In relazione all'articolo 4, in Commissione è stato bocciato il nostro emendamento che prevedeva la sfiducia costruttiva. Ci sembra evidente, a questo punto, che c'è il tentativo di affossare il reale problema costituzionale a tutti noto da tempo: la debolezza del Parlamento. Una revisione consapevole della Costituzione, allora, dovrebbe innanzitutto rafforzare il Parlamento e, in tal modo, indirettamente, ristabilire i giusti rapporti con gli altri poteri, tanto il Capo dello Stato quanto lo stesso Governo. È questo l'unico modo per riconoscere davvero ruolo e protagonismo dei cittadini, dando loro maggiore possibilità di scelta per eleggere i propri rappresentanti, cambiando la legge elettorale per superare le liste bloccate e contemporaneamente dare piena attuazione all'articolo 49 della Costituzione, che vede nei partiti politici gli organismi attraverso i quali la volontà popolare incide sulle scelte, a cominciare dalla definizione delle liste elettorali fino agli indirizzi da esprimere in Parlamento. Si tratta di scelte che con ogni evidenza non si compiono, come vorrebbe questa riforma, una volta ogni cinque anni. Abbiamo tentato di inserire il tema del *quorum* per tutelare le prerogative della minoranza e quindi cominciare a delineare dei contrappesi allo strapotere del *Premier*. Ma la destra è sorda a questa esigenza di riequilibrare i poteri, che è fondamentale in una democrazia. In particolare, il fatto che il Parlamento sia eletto a trascinamento del *Premier* eletto, mette nelle disposizioni del *Premier* lo stesso Parlamento e anche il Presidente della Repubblica, visto che il *Premier* lo potrebbe eleggere da solo con la propria maggioranza. nessun peso e contrappeso, come invece prevede il semipresidenzialismo alla francese, separando l'elezione del Presidente della Repubblica da quella del Parlamento. Uno dei limiti più gravi del disegno di legge costituzionale in esame è proprio il mancato riconoscimento in Costituzione dei diritti e delle garanzie delle opposizioni. Abbiamo a più riprese proposto l'inserimento in Costituzione - e non nei Regolamenti parlamentari, che sono una fonte del diritto di diverso livello - della facoltà di deputati e senatori di adire la Corte costituzionale, come avviene in Francia, Germania e Spagna; della previsione dello statuto delle opposizioni; dell'innalzamento delle maggioranze richieste per l'elezione degli organi di garanzia, come i Presidenti delle Camere e il Presidente della Repubblica, e per l'approvazione dei Regolamenti parlamentari; della riserva di spazi dedicati alle iniziative delle opposizioni nel calendario dei lavori, nonché di limiti più rigorosi per la decretazione d'urgenza. A fronte di tali proposte, la maggioranza ha opposto un atteggiamento di totale chiusura, peraltro senza motivare la sua contrarietà. Questo tentativo di accentramento del potere configura una società dove l'individuo assume un ruolo più passivo, inserito in una struttura che svaluta la pluralità e promuove un'organizzazione quasi organicistica. Tale impostazione trova riscontro e coerenza in una serie di politiche e misure già intraprese o annunciate dal Governo, che interessano ambiti critici quali immigrazione, istruzione e giustizia. In questo quadro si colloca quasi incongruamente la proposta di legge sull'autonomia differenziata, che tuttavia condivide la tendenza a ridurre il ruolo del Parlamento.

ulteriore dimostrazione di un allontanamento dal modello di democrazia parlamentare verso una concentrazione di poteri esecutivi. La nostra responsabilità è far recuperare ai cittadini una percezione positiva della funzione democratica della rappresentanza. È imperativo impegnarsi con determinazione per una piena attuazione dei princìpi sanciti dalla nostra Costituzione, al fine di superare l'attuale contesto che vede una predominanza del potere esercitato individualmente da sindaci e governatori regionali, ma soprattutto la centralità del decisionismo esercitato da Palazzo Chigi, che si manifesta attraverso un ricorso eccessivo a decreti e alla richiesta di voti di fiducia. Questa riforma aggredisce alcuni dei pilastri costitutivi dello spirito costituente, dello spirito dei nostri cittadini e del nostro Paese. Noi ci opponiamo duramente oggi, continueremo ad opporci con fermezza e ad organizzare la resistenza dell'opinione pubblica, a difendere il nostro ruolo, il ruolo ruolo delle istituzioni e a difendere una società aperta e plurale. Presidente, oggi ci troviamo di fronte a un bivio: scegliere tra la difesa della nostra Costituzione o l'abbandono dei suoi princìpi fondanti.

Questa forzatura giunge proprio alla vigilia - come sempre vediamo - di un'importante competizione elettorale, mettendo in discussione addirittura i fondamenti della democrazia e anche del nostro continente. Il premierato della presidente Meloni, come proposto in questo disegno di legge, non solo concentra eccessivi poteri nella figura del Primo Ministro, che li rivendica continuamente, ma svuota di fatto il significato del Capo dello Stato, in un momento storico così delicato, in cui l'Europa si trova ad affrontare sfide cruciali future. È inaccettabile, in questo momento, indebolire la figura di garanzia che rappresenta l'unità nazionale e la sovranità popolare. Contrariamente a quanto dichiarato dai suoi proponenti, questa riforma non porta alcun beneficio al Paese, non garantisce il rispetto della volontà popolare, ma anzi istituzionalizza il ribaltone elettorale e annichilisce il ruolo del Parlamento. Inoltre non incentiva la partecipazione dei cittadini, come dimostrato anche dai drammatici

questo disegno di legge, sembra veramente che il Parlamento stesso viva di una sindrome di Stoccolma del Presidente. Siamo arrivati - ve lo dico, colleghi oltre le fiducie del Governo Draghi, siamo arrivati oltre quello che era stato un Governo di unità nazionale, l'abbiamo sorpassato. Il vostro ruolo in questo momento è completamente esautorato da questo Governo; voi venite qui esclusivamente a ratificare quello che decide il Governo. *(Applausi)*. C'è stato, in questo Paese, un momento di unità di intenti e il Presidente della Repubblica, a garanzia di tutti i Gruppi politici del Paese, aveva chiesto quel Governo.

La scelta di inserire in Costituzione un premio di maggioranza, che addirittura avevate anche quantificato e che poi avete ridotto in maniera indefinita, supera l'indecenza della legge Acerbo. È un atto inaccettabile e arrogante. Inoltre, questo meccanismo per la scelta del successore del Presidente del Consiglio ricorda norme adottate in un passato che ci siamo lasciati alle spalle e che ha minato la democrazia di questo Paese. Tutto questo è sintomo della visione autoritaria di una destra che considera la gestione del potere come unica gestione del Paese. La maggioranza con la sua forza, con la sua arroganza e con il suo disprezzo delle istituzioni democratiche sta umiliando questo Parlamento. Utilizza solo la forza dei numeri per imporre delle scelte. Quella forza gli è derivata in particolare da un momento drammatico per questo Paese. Il momento più drammatico è stato quello della pandemia; durante quel momento e durante quei Governi, questa forza politica ha preso una maggioranza all'interno del Paese su due principi. Il primo era quello della pandemia, il secondo era quello dell'immigrazione; ma nessuna di queste cose ha insegnato nulla alla maggioranza. La pandemia ha insegnato una cosa, cioè che la sanità doveva essere messa al primo posto, Presidente. E invece stiamo vedendo che, dopo due manovre di bilancio, continuate a tagliare e a investire il meno possibile sulla sanità, raccontando continuamente menzogne a questo Paese. Il secondo era quello dell'immigrazione, che avete miseramente fallito, raddoppiando le entrate dell'immigrazione e spendendo milioni di soldi degli italiani in presidi in Albania, che stanno dando risultati pessimi e che non funzioneranno. Con queste false promesse avete raggiunto questa forza dei numeri. L'atteggiamento del Governo è l'ulteriore dimostrazione dell'arroganza dimostrata rispondendo a metà delle interrogazioni presentate da questo Parlamento. Quello che chiedono i cittadini e i parlamentari non ha praticamente avuto risposte; è un segnale di chiara mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e dei cittadini.

nel raggiungere i propri obiettivi, quali saranno le sue reali conseguenze? I cittadini devono porsi questo interrogativo e ricordare che la sovranità appartiene al popolo, come recita la nostra Costituzione. Presidente, per queste ragioni questa mattina molte forze politiche hanno presentato delle pregiudiziali di costituzionalità contro questo disegno di legge, ma ovviamente il meccanismo della maggioranza relativa di questo Paese ha imposto per l'ennesima volta una linea che dal nostro punto di vista appare sbagliata. Non possiamo permettere che la nostra democrazia sia svuotata di significato e che i principi fondanti della nostra Costituzione vengano calpestati. Dobbiamo difendere il Parlamento, il Capo dello Stato e la sovranità del popolo italiano. Respingiamo questo disegno di legge con fermezza e invitiamo - tutti quanti lo faremo in tutte le sedi possibili - a difendere la nostra democrazia. Non vogliamo e non possiamo permettere che questo premierato

ho preso parte anch'io nelle scorse settimane e negli scorsi mesi a diverse sedute della 1a Commissione, così come hanno fatto tanti colleghi e colleghe del Partito Democratico. Non sono un membro permanente di quella Commissione, ma sono stata mossa dalla convinzione che su una materia così importante e cruciale per il funzionamento del Paese come è una materia che mette mano alla Costituzione - sia dovere, oltre che diritto di ogni singolo parlamentare, intervenire nel merito, secondo le proprie competenze, la sensibilità propria e della parte politica e sociale che si rappresenta. ovviamente sempre nell'interesse prioritario del Paese che, come è noto e come noi siamo convinti essere, viene prima di quello di ogni singola parte politica. Chiunque di noi abbia avuto modo non dico di studiare, ma almeno di guardare i resoconti dei lavori dell'Assemblea costituente avrà senz'altro potuto apprezzare come i Padri e le Madri costituenti abbiano sentito abbiano sentito il dovere di contribuire alla scrittura di quel testo, ciascuno e ognuno in prima persona. Giudicherà ovviamente chi verrà dopo di noi se il percorso che ci ha condotto sin qui sia stato all'altezza dell'afflato costituente di cui tutti noi siamo figli. È probabilmente vero che siamo tutti nani sulle spalle dei giganti, ma io sono convinta che a noi spetti almeno la responsabilità di conservare l'ambizione di meritare la parte di storia migliore che ci ha condotto fino a qui. Non ho potuto avere il piacere di conoscere il punto di vista di diversi colleghi della maggioranza, per esempio sugli emendamenti che abbiamo presentato in 1a Commissione con uno spirito sinceramente e genuinamente costruttivo, come spesso ha rappresentato il nostro Capogruppo, il collega Giorgis. Colleghi, spero che almeno il dibattito che ancora abbiamo davanti in Aula ci consentirà questo scambio di opinioni e di punti di vista con ciascuno di noi e di voi. In realtà, il dibattito che è stato svolto fino a questo momento è stato dominato da interventi di esponenti delle opposizioni, ma abbiamo ancora tempo - auspico molto, spero sia sufficiente ad approfondire questa materia per poter ascoltare anche i colleghi delle forze di maggioranza. Noi crediamo fermamente nel valore della democrazia parlamentare ed è questo uno dei principi che ha ispirato tutto il percorso che il Partito Democratico ha svolto anche in Commissione e la sua strategia emendativa. È per questo che il modello di premierato che ci proponete non ci convince affatto, non solo perché si tratta, come è stato rilevato da altri colleghi, di un modello che non ha simili in nessuna democrazia europea, ma perché altera l'equilibrio dei poteri non tra il Parlamento e il Presidente della Repubblica, come avviene nelle forme di governo che vedono l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma perché altera l'equilibrio tra Parlamento e *Premier*, colui cioè che dovrebbe essere un *primus inter pares* nell'ispirazione della nostra Costituzione. Questa operazione schiaccia la complessità dell'esercizio della rappresentanza all'elezione di un solo capo, che si porta poi dietro pattuglie di eletti al seguito, non di pari con cui confrontarsi - alla pari, appunto - nel dibattito parlamentare. Per questo gli emendamenti che il Partito Democratico ha presentato alla prima parte del testo della riforma, che viene perciò definita del premierato, sono tutti accomunati dall'intento di ripristinare come prioritaria la legittimazione del Parlamento sul *Premier* e di razionalizzare il potere presidenziale di scioglimento del Parlamento, chiarendone i presupposti, senza tuttavia svilirlo e senza subordinarlo rigidamente alle dinamiche del rapporto fiduciario e quindi senza far venire meno la necessaria flessibilità fisiologica di ogni forma di governo parlamentare. La conseguenza più diretta dell'elezione del Presidente del Consiglio dalla legittimazione popolare è proprio quella di irrigidire in una serie di automatismi il il rapporto tra Parlamento e *Premier*, facendo venire meno, anche in situazioni di eccezionale difficoltà non solo politica, la possibilità di formare in Parlamento altri Governi. Questo dispositivo, almeno così è il racconto che le forze di Governo e di maggioranza ne fanno, ha l'obiettivo di garantire una maggiore stabilità del *Premier* e dei Governi in carica. Presidente, mi lasci dire che questa idea della costruzione della stabilità assomiglia più alla costruzione di una forma di vassallaggio che ad un'idea degna di una democrazia matura, dove la creazione e la gestione del consenso avvengono intorno a progetti politici e di Governo, non secondo meccanismi di ingegneria istituzionale che legano il *Premier* al suo seguito di parlamentari eletti. Garantire la stabilità prendendo una scorciatoia nella storia non è mai stato compatibile con la democrazia, la democrazia è un esercizio più complesso che ha a che fare con la costruzione di processi che sono di natura politica e la stabilità del *Premier* e delle maggioranze deve essere una stabilità garantita dal consenso politico, dalla serietà e condivisione di un progetto di Governo, non da un meccanismo istituzionale ingegnerizzato a tavolino, come prova a fare questo testo. Per ragioni di tempo, non potrò soffermarmi a lungo su altri aspetti che hanno acceso il dibattito anche in Commissione e nel Paese, *in primis* lo svilimento del ruolo del Presidente della Repubblica. Questo - Presidente, mi lasci fare una riflessione di buonsenso va contro tutto quello che i cittadini italiani da anni ci suggeriscono quando rispondono ai sondaggi demoscopici indicando nel Presidente della Repubblica l'istituzione che gode del maggior grado di fiducia. Non si capisce qual è la ragione per cui smontare questo rapporto di fiducia che è un rapporto di fiducia, ancorché non mediato dal voto diretto di natura popolare. Checché ne dicano diversi esponenti di Governo e di maggioranza, questa riforma intacca profondamente il ruolo del Presidente della Repubblica, non solo perché gli sottrae diverse prerogative (non ultima la nomina dei senatori a vita), ma perché ne consente l'elezione attraverso una maggioranza meno qualificata di quella attuale e intorno alla quale è più difficile costruire un consenso trasversale tra le forze, che è l'elemento che ha garantito e preservato il Presidente della Repubblica anche agli occhi dei cittadini. Non dirò a lungo del grave *vulnus* rappresentato dal fatto che noi ci apprestiamo a votare e a discutere questa riforma in in mancanza di chiarezza su quale sarà la legge elettorale che sarà alla base e che farà da sostrato alla riforma stessa, cambiandone la natura a seconda del modello elettorale adottato. Non lo farò e desidero soltanto concludere con una riflessione di altra natura, cioè sul contesto complessivo in cui questa nostra discussione si svolge; un contesto che, a partire dal ritorno della guerra nel cuore dell'Europa, per arrivare alla crescita galoppante delle disuguaglianze tra i cittadini, tra i gruppi sociali e anche tra i territori, è probabilmente quanto di più lontano dall'idea di pace, uguaglianza e prosperità che i nostri predecessori in queste Aule avevano in mente per il futuro del Paese e dell'Europa. Questo mi porta a ritenere che l'agenda che la maggioranza e il Governo ci stanno proponendo, tutta concentrata sulla sbilenca coppia premierato-autonomia, sia quanto di più distante quello di cui i cittadini, il Paese e anche l'Europa hanno bisogno. Avrei preferito che le nostre energie, oggi pomeriggio e nei pomeriggi che verranno, fossero impiegate nella spasmodica costruzione di un'Italia e di un'Europa capaci di farsi attori di mediazione e di pace nei conflitti conflitti che ci circondano, per esempio nella ricerca di una via per una crescita capace di chiudere il *gap* tra chi ha sempre di più e chi ha sempre di meno, tra le donne e tra gli uomini, tra chi riesce a tornare la sera dal lavoro e chi invece non riesce a farlo. veramente alla conclusione, il sospetto che noi abbiamo e che io desidero rappresentare in quest'Aula è che non solo questa riforma sia sbagliata nel merito e nel metodo con cui siamo arrivati alla discussione di oggi, ma anche che ci porti ben lontano dal cuore dei problemi che oggi il Paese e i cittadini italiani hanno di fronte.

prendo la parola con gravi difficoltà su questo disegno di legge di revisione costituzionale, perché più che essere di revisione costituzionale è di eversione costituzionale nasce da una serie di gravissimi equivoci, il primo dei Ne do documentazione puntuale e storica. Nell'accordo di programma intitolato «Per l'Italia», presentato il 12 agosto 2022, a firma di Meloni, Salvini e Berlusconi, figurava, prima tra le riforme, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Successivamente si è perduta per strada. Dopo una gestazione di ben dodici mesi, quale quella dell'asina, in un accostamento che non è oggetto di mio *copyright*

tranne il breve caso, peraltro presto abortito, di Israele. Se volessimo utilizzare le categorie della biologia applicandole al diritto costituzionale, dovremmo dire che è una mutazione genetica della Costituzione su base quasistica. L'elezione del *Premier* è per metà popolare e per metà parlamentare. Il modello è quasi presidenziale ed è quasi parlamentare, senza essere né l'uno né l'altro. Quindi, è un ircocervo, un ircocervo giustificato da che cosa? Se leggiamo la relazione che accompagna il disegno di legge, sentiamo decantare le qualità in termini di efficienza, di decisionismo, di sveltezza dei procedimenti deliberativi. Tutti principi che non trovano conforto nella prova storica e fanno rabbrividire, perché io ho notato, con grande apprensione, una identità concettuale e una somiglianza persino lessicale, con un celebre discorso fatto nel 1924, in occasione il Governo deve essere un istituto atto a risolvere nel modo più rapido, fermo e univoco tutte le molteplici questioni che nell'azione quotidiana si presentano, non impacciato da preventive compromissioni, non impedito da divieti insormontabili, non soffocato da dissidi. Così Benito Mussolini. Ma è proprio necessario varare questo ircocervo giuridico, responsabile di questa mutazione genetica ed eversiva della Costituzione, per raggiungere questi traguardi di efficienza e di incisività della produzione normativa?

cinque e tre Governi e abbiamo varato la disciplina del *referendum*, lo statuto dei lavoratori, l'istituzione delle Regioni, la riforma del diritto di famiglia, la legalizzazione dell'aborto, la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi, l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. Dunque, non è vero Le scorciatoie sono percorsi che piacciono ai *caudillos* sudamericani non sono consone ad una democrazia effettiva che, per essere vitale, deve essere necessariamente conflittuale. *(Applausi)*. La vitalità della democrazia, si misura sulla conflittualità e sulla capacità di mediazione. L'altro equivoco sul quale devo intrattenermi rapidamente è che la maggioranza considera la Costituzione una sorta di regolamento condominiale. Il regolamento condominiale, come si sa, è appannaggio di chi ha le maggiori carature della proprietà. Questo, però, colleghi, è un patrimonio che appartiene a tutto il Paese, a tutta la comunità, indifferenziatamente alla maggioranza e all'opposizione. Voi non potete arrogarvi questo premio di maggioranza, andando a svellere principi fondamentali della Costituzione, soltanto perché avete ricevuto dei voti in più. Voti che avete ricevuto gabbando gli elettori, perché avete detto loro di avere come programma di Governo la madre delle riforme, che andavate a modificare l'assetto del Presidente della Repubblica laddove, invece, state modificando l'assetto del capo dell'Esecutivo. Avete frodato il vostro elettorato e ne risponderete in sede di *referendum*, perché la gente capirà finalmente che avete fatto il gioco delle tre carte. Passo ad altro argomento importante: è stato detto egregiamente dai colleghi che mi hanno preceduto che il principio fondamentale della nostra Costituzione è quello dell'equilibrio tra i poteri fra gli organi costituzionali, non sono a compartimenti stagni. Sono organi in cui la sfera di potestà di ognuno coincide con i confini della sfera di potestà dell'altro: non c'è un potere che possa troneggiare sugli altri, perché, se ciò accade, si determina la tirannia di questo potere a danno degli altri e si scuote dalle fondamenta l'equilibrio costituzionale. Vedete, la Corte costituzionale ha detto chiaramente con una sentenza del 1988

Questi principi sono il principio democratico e il principio dell'equilibrio tra i poteri. State facendo l'ennesima legge incostituzionale, come quella dell'autonomia differenziata, che credo batta batta il *record* dei vizi di incostituzionalità. Ne elencai ben dieci in quest'Aula, ma poi, riflettendoci sopra, ne ho trovati anche altri due, e ne parleremo al momento opportuno.

che dice che questa riforma è proprio il rovescio di quella che avrebbe dovuto essere fatta, perché se oggi c'è un potere debole che andava avvalorato e puntellato è quello del Parlamento.

L'abrogazione è già iniziata con la riforma dell'autonomia differenziata, quando il Parlamento della Repubblica ridotto al rango di organo che esercita un blando potere consultivo sulle intese devolutive delle competenze dallo Stato alle Regioni, in violazione dell'articolo 117 della Costituzione.

è una legge suicida? Voi siete parte di questo Parlamento, state votando una legge contro il vostro *status* giuridico: è una questione di dignità e di orgoglio, ribellatevi e acquisite consapevolezza di quello che state facendo. Fate vostro il monito di Mattarella, che qualche settimana fa, quando si è incontrato con i giovani *influencer*, ha detto due concetti che dovremmo tenere presenti, perché abbiamo l'obbligo morale e giuridico di farlo: la nostra Costituzione è giovane,

Il secondo concetto è l'unità d'Italia (all'articolo 5, primo comma, della Costituzione), che avete avviato a dissoluzione con la sciagurata riforma dell'autonomia differenziata. Teniamo conto di questi moniti e abbiamo ancora il tempo di rimediare. Quest'Assemblea oggi da più parti vi ha rivolto

della follia». *(Applausi)*. Stiamo vivendo giorni di follia: cerchiamo di porvi riparo e cerchiamo di recuperare il significato vero dalla nostra Costituzione, fondata

sentimento di rispetto nei confronti dei senatori a vita, che sono stati "decapitati". Ho letto con con un senso di malessere la norma transitoria, che dice loro che saranno trattenuti in servizio

e auguro - checché ne pensi il redattore della norma, che probabilmente li ha conformati come ospiti sgraditi che si trattengono oltre il dovuto, come quando si invita un ospite a casa propria - che ci rimangano per tanti anni ancora e che si avveri il detto profetico del Libro della Genesi, quando il buon Dio disse all'uomo: Vivrai fino a centoventi

un argomento che sento ripetere molto spesso in questo periodo, a proposito di come spiegare al Paese il cambiamento della Costituzione: non lo chiamerei infatti "riforma", non trovando nessun elemento positivo che mi faccia utilizzare questo termine. Il cambiamento della Costituzione che volete proporre richiama spesso questa idea: i cittadini avranno esplicitamente la possibilità di votare il Presidente del Consiglio e questo li renderà più partecipi di questa soluzione. Già altri colleghi, intervenendo in questa sede, hanno ricordato quanto sia difficile dire che i cittadini italiani non sapessero già prima quali candidati Presidenti del Consiglio stessero votando: è una bugia che si racconta, per dare un valore aggiunto. Quello che mi preoccupa davvero è l'idea di fondo che c'è in questo messaggio e cioè che la democrazia si riduce all'espressione del voto, ovvero che è sufficiente la presenza del suffragio universale per dire che siamo dentro una democrazia compiuta. Vi suggerirei di fare qualche attenzione, perché ho presente, anche nella stessa Europa geografica, qualche Paese in cui ci sono dei veri e propri brutali dittatori, che pure godono del suffragio universale e lo utilizzano. Se c'è una Se c'è una ricchezza della nostra Costituzione, è esattamente il fatto che non riduce la democrazia alla sola partecipazione al voto, ma immagina e pensa che siamo una Repubblica democratica, fondata sulla democrazia parlamentare, che risponde a una sovranità del popolo, che non si riduce al minuto del voto, ma che si traduce attraverso la partecipazione. Se dunque pensiamo - credo che dovremmo pensarlo e in verità mi stupisce che se ne discuta troppo poco - che una delle crisi politiche del Paese è esattamente quella della poca partecipazione dei cittadini alla politica - e mi permetto di sottolineare anche della poca partecipazione al voto e se l'argomento è quello che, se i cittadini possono nominare il Presidente, allora parteciperanno, basta guardare tutti i risultati delle ultime elezioni regionali per scoprire che non è l'indicazione del Presidente che porta o non porta al voto, ma è il rapporto che c'è tra i cittadini e la politica, il rapporto che c'è in termini di fiducia nelle istituzioni e il sentirsi o meno coinvolti e rappresentati dal voto.

dell'accentramento dei poteri nel ruolo di qualcuno, ma nel domandarsi invece come si ricostruisce un'idea di rappresentanza. Se c'è un indebolimento della partecipazione dei cittadini alla vita politica, forse una delle risposte che dovremmo darci è quale ruolo e spazio hanno oggi i corpi intermedi nel nostro Paese, che sono stati progressivamente ridotti dal punto di vista della loro possibilità di rappresentare e interloquire con il potere politico. La seconda domanda che forse dovremmo farci è se democrazia è tutela delle maggioranze o è invece tutela delle minoranze e quanto più si afferma l'idea che la democrazia sia solo quella delle maggioranze, più le persone si sentiranno escluse e non incluse, si sentiranno in qualche modo giudicate e tagliate fuori. E se noi proviamo a guardare e a domandarci chi sono quelli che non partecipano al voto, scopriremmo - e lo sappiamo in realtà da tempo - che sono spesso coloro che fanno più fatica ad essere centrali nella società. Sono quelli che magari hanno un lavoro povero, quelli che magari non trovano casa, quelli per cui le periferie sono l'unico mondo possibile, quelli che magari non riescono a curarsi o hanno difficoltà ad affermare i loro diritti. Allora la prima risposta che bisognerebbe dare loro per ricoinvolgerli in una partecipazione democratica è esattamente quella di poter usufruire dei diritti. Ma come si fa a dire a delle persone che si può usufruire dei propri diritti, diritti, se i corpi intermedi di rappresentanza non ci sono e se il potere si accentra progressivamente, in un misterioso conflitto tra autonomia e accentramento in cui non si capisce? Ma in fondo si capisce, perché poi nel Presidente del Consiglio si radunano tutte le possibilità e le risposte. A me verrebbe in mente di ricordarci che il 2 giugno del 1946 questo Paese ha votato per la Repubblica. Aveva la possibilità di scegliere un modello accentrato di potere e un modello di comando, invece che di governo. Scelse il governo e la democrazia. Forse dovremmo ricordarcelo e proprio per questo è giusto, il 2 giugno, discutere profondamente di quale deve essere il nostro modello. modello. Però è evidente che se non si affrontano i temi della rappresentanza e della partecipazione dei corpi intermedi e non si affronta la fatica che la politica fa e i partiti politici fanno a interfacciarsi con la pluralità delle opinioni, con la volontà di partecipazione, con la capacità di dare se non si risponde in questo modo, ma si sceglie la strada che voi definite del premierato e che a me pare quella del capo senza contraddittorio da questo punto di vista), allora bisogna dire che la strada che invece bisognava seguire era quella di pensare se, per esempio, una delle ragioni della solitudine delle persone e della non volontà di partecipare, non sia anche figlia di un modello elettorale che progressivamente ha ridotto il senso del loro Ha ridotto, cioè, quella vicinanza tra coloro che eleggi e le persone che conosci nel territorio; ha ridotto quella vicinanza tra chi vorresti che facesse, per esempio, attività nelle amministrazioni o in Parlamento e la possibilità di esprimere quel voto. voto. In realtà, i cittadini ci hanno già detto che i modelli di accentramento e di scarsità di equilibrio di poteri a loro non piacciono. Allora questa non è la risposta alla crisi della politica e alla crisi della partecipazione. È forse la risposta alla crisi del Parlamento? Sento di nuovo dire che c'è un problema di funzionamento di velocità e di attuazione del volere governativo da parte del Parlamento. Evidentemente io sto su un'astronave e non in questa Camera, perché in verità posso dire che in questi due anni noi abbiamo votato decreti, atti di governo e non siamo ancora riusciti a fare una discussione vera su un progetto di iniziativa parlamentare. *(Applausi)*. Questo non aiuta la fiducia del Paese, non aiuta l'idea dei cittadini che noi stiamo in questa Assemblea legislativa perché stiamo lavorando per loro. La sensazione è quella che si voglia tenere il Paese nella perenne emergenza. Ci sono sempre un decreto e un'emergenza da risolvere, mai un elemento di prospettiva o un elemento di visione. Vorrei dire che il fatto che si lavori così indica una propensione al comando che ha per il momento la sua apoteosi nel fatto che si ripete il voto se non va come vuole il Governo. Guardate che questa è una violazione straordinaria della democrazia *(Applausi)* e dice innanzitutto ai cittadini che non ha importanza il loro voto, perché poi chi è qui non può esercitare il suo mandato, non può decidere quali sono le sue opinioni. Sono abituata a pensare che un Paese che ha bisogno degli eroi, che ha bisogno dei gesti dimostrativi per affermare i più banali diritti è un Paese che ha qualche problema e qualche malattia. malattia. L'idea che ci sia un Parlamento che è eletto per trascinamento del Presidente del Consiglio, un Parlamento dentro il quale non si può decidere di avere un'opinione diversa dal Governo perché bisogna acconsentire a ciò che il Governo chiede, sia o una domanda di eroismo ai futuri eletti oppure la sanzione che in realtà non si vuole una democrazia parlamentare. È la sanzione, in realtà, che si immagina che le difficoltà che ci sono non si superano con la dialettica, con l'autonomia del pensiero, con la capacità di confrontarsi - d'altra parte, questo dibattito rischia sempre di più di essere un monologo invece che un dibattito in Parlamento - ma si affronta invece esclusivamente obbedendo agli ordini di qualcuno. Credo che questo Paese non meriti una scelta di questo tipo. Peraltro l'esperienza recente ci dice che quando si propone un cambiamento così radicale, senza aver fatto una discussione nel Paese, senza averla fatta maturare, senza aver ragionato delle possibilità alternative, le risposte non sono mai state positive; anzi, i cittadini ci hanno sconsigliato dal manomettere ciò che pensano giustamente sia un loro diritto di partecipazione. Guardate Guardate che nella politica, nel nostro Paese come in qualunque altro Paese, la ruota gira e chiunque abbia immaginato e pensato di costruire degli esperimenti di accentramento del potere che non avessero equilibri, non solo ha peggiorato la democrazia, non solo l'ha resa più fragile, ma poi se ne è - credo e temo - amaramente pentito quando non è più toccato a lui stare al timone. Non si può immaginare una riforma della Costituzione e un cambiamento della democrazia del Paese in ragione del fatto che ci si immagina che si sarà quelli che governeranno da qui all'eternità. Non si può pensare questo altrimenti ciò risponde non al fatto che stiamo immaginando quali sono le forme migliori di partecipazione, quali sono le forme migliori di Governo, come possiamo dare la stabilità, ma perché si sta in realtà immaginando che c'è una possibilità di comandare. La possibilità di comandare determina alcune delle distorsioni che stiamo già vedendo: è quella che poi richiede che ci sia un'informazione che è al servizio di quel comando e che non rappresenta più la realtà per quella che è; è quella che ha bisogno di scelte che, dal punto di vista del rapporto con la questione sociale, non si occupino dei problemi dei lavoratori, dei salari e della loro condizione, ma invece affermino che c'è sempre un altro altro colpevole, che è fuori da noi e dalle responsabilità che abbiamo. Si continua ad affermare, se si continua a eccedere nella logica del comando invece che del Governo, che chi è in difficoltà è un colpevole, invece di essere una persona che deve poter esercitare i suoi diritti e partecipare. Vorrei unirmi unirmi alla richiesta che hanno fatto molti colleghi negli interventi precedenti: provate a fermarvi; provate a non pensare che si può fare una prova di forza perché così si afferma; provate a domandarvi come farete a rispondere ai cittadini che pensano che il Presidente della Repubblica sia la figura migliore che abbiamo in questo Paese (lo dicono da anni). Che cosa direte loro nel momento in cui toglierete la possibilità a quella figura di esercitare il suo ruolo? Provate a immaginare che cosa potrete rispondere a chi vi dirà: dopo il voto, come esercito la mia partecipazione e la mia possibilità di essere rappresentante? *(Applausi).* Che effetto ho rispetto al futuro e alla prospettiva di sapere che magari i Governi durano un po' di più, ma non rispondono alle esigenze esistenti? Vorrei anche dire che i Governi sono durati poco non in ragione del fatto che i meccanismi costituzionali non funzionavano; anzi, ciò che ha salvaguardato esattamente la Repubblica e il suo andamento è stato che i meccanismi costituzionali funzionavano. Ciò che ha causato le crisi dei Governi era la relazione nelle coalizioni o l'insufficiente consenso politico rispetto alle scelte che si facevano. Eppure, in tutti quegli anni a nessuno è venuto in mente di sostituire la necessità di costruire il consenso con l'idea di imporlo; quando si impone il consenso, vuol dire che non si ha nulla da proporre davvero a chi si vuole rappresentare.

Grazie, Presidente, colleghe, colleghi, membro del Governo. Sottosegretaria, la vedo annoiata mi dispiace per la mancata presenza dei Ministri, in particolare della ministra Alberti Casellati, che è stata qua un po' e poi ha preferito abbandonare il campo, anche perché avrò la possibilità in ogni caso, per il suo tramite, Presidente, e anche per il tramite del rappresentante del Governo, Mi dispiace dire che, in un'Aula vuota, vedo vuoti anche gli scranni o i posti riservati ai giornalisti. Qua abbiamo però una rappresentanza delle future generazioni, che possono - ahinoi - assistere un esercizio di mera retorica. Purtroppo stiamo trattando di un tema importantissimo: parliamo di una modifica costituzionale. E come l'affrontiamo? In un'Aula vuota, dove Fratelli d'Italia ha una buona rappresentanza, nell'assenza totale di Forza Italia e con qualcuno della Lega; comunque il vuoto quasi assoluto. Le opposizioni sono qua presenti a far sentire forte la propria voce e il grido d'allarme per quello che è un potenziale attentato alla vita democratica del Paese. un invito accorato anche a chi ci permette di ricoprire questi importanti ruoli. Mi rivolgo, per il suo tramite, Presidente, ai cittadini italiani, agli elettori: ponete la massima attenzione a questo disegno di legge, a questo terribile disegno di legge, che rischia di ribaltare alcuni dei fondamenti della nostra bella Carta costituzionale.

e la chiamo il grande inganno. *(Applausi)*. Questo è un grande, enorme inganno nei confronti degli italiani e degli elettori. Abbiamo più volte sentito, a giustificazione di questa terrificante legge, che loro, quelli bravi, quelli preparati, quelli che due anni fa dicevano di essere pronti a trovare le soluzioni, avevano già in tasca ogni soluzione per i problemi degli italiani. Secondo voi i problemi degli italiani li risolviamo in questo modo, portando una donna o un uomo solo al comando con una riforma costituzionale che voi, mentendo agli italiani, non avevate promesso in campagna elettorale? Presidente - ahinoi - invito i cittadini italiani ad andare a visitare il sito di Fratelli d'Italia, delle

Perciò giù le tasse dal lavoro: legge di bilancio 2024. Nel programma di Fratelli d'Italia 2022 poi, giù in basso, troverete "scarica il programma in PDF". Cliccate italiani e andate a trovare la grande truffa, il grande inganno. La pagina non può essere trovata, hanno cancellato pure il loro programma elettorale. *(Applausi)*. Andate italiani, andateli a vedere questi mentitori seriali. Qua ci sono le prove del grande inganno. Noi vi portiamo le prove. Italiani andate sul sito dei parenti d'Italia, cognati compresi per trovare il programma. Ora, ahinoi, il programma del centrodestra sono andato a cercarlo in giro per il *web*. I grandi mentitori seriali, al punto 3 del loro programma (accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra, tra cui, ben in vista i simboli di Berlusconi, Forza Italia e famiglia, Lega, Salvini, Meloni and *company*, Noi Moderati),

portando avanti una promessa fatta ai vostri elettori, al di là del fatto che - ribadisco - voi dimostrate di essere soltanto dei prepotenti, utilizzando una maggioranza che, come hanno detto bene tanti colleghi, non rappresenta la maggioranza degli elettori italiani e del Paese. *(Applausi)*. Voi volete modificare la Costituzione con l'inganno senza avere i numeri.

minano quella che è la credibilità di tutta la politica italiana. Noi dobbiamo fondare il rapporto con gli elettori sulla verità, non sulla menzogna. *(Applausi)*. Pertanto, al di là degli esercizi retorici o della semantica, mi dica lei qual è il termine appropriato per aver mentito all'Italia e agli italiani. Mi dica. Imbroglio è meglio? Piace alle maggioranze?

completare il suo intervento. I colleghi di maggioranza possono iscriversi in discussione generale e intervenire. *(Commenti)*. Ho ripreso il senatore quando ha usato un termine non consono, ora mi sembra che il suo intervento sia assolutamente

a loro fa male, mentre gli italiani devono conoscere con attenzione *(Applausi)* e vi invito nuovamente ad andare a vedere. Avete cancellato dal vostro sito internet il programma elettorale. Vi vergognate pure di quello che avete scritto. Vi vergognate anche di questo. Tornando al tema, voi state minando i fondamenti della democrazia costruiti dai Padri costituenti dopo un ventennio terribile di dittatura.

Senatore se vuole intervenire, la iscrivo in discussione generale. Colleghi, il senatore Lorefice completa il suo intervento. Se il senatore Zedda vuole iscriversi in discussione generale, la iscriviamo così può replicare. Prego, senatore Lorefice, vada avanti. Presidente, riparto da quello che stavo dicendo. I Padri costituenti, dopo un ventennio terribile di dittatura assoluta e dopo milioni di morti, hanno costruito una Costituzione mettendo dei bilanciamenti, degli equilibri che questa maggioranza vuole totalmente sovvertire, relegando il Presidente della Repubblica al ruolo neanche di un normale notaio. Pertanto, consegnare nelle mani di una sola persona le sorti di una Nazione e il futuro delle nuove generazioni

Presidente, visto che si sono tanto accalorati, finisco dicendo soltanto che noi, insieme a tutte le forze di opposizione, continueremo a batterci e ad avere sempre una voce chiara a difesa dei tanti elettori e cittadini italiani che credono ancora nella libertà, perché è anche a rischio la libertà della Nazione italiana e di tutte

senatrici e senatori, con l'arrivo in Aula di questa proposta di riforma costituzionale siamo ad un passaggio che io voglio definire con forza drammatico della nostra storia repubblicana. Mai si era visto uno scambio politico-elettorale arrivare a mettere in discussione la nostra Costituzione. La riforma del premierato non nasce per affrontare i problemi della nostra democrazia, primo tra tutti il crescente astensionismo, ma per consolidare una visione dei sistemi di Governo schiacciata sulle *leadership*, con il rischio di produrre danni ancora peggiori in termini di partecipazione dei cittadini alle scelte politiche. Ad un mese dalle elezioni europee, con i manifesti "vota Giorgia" che stanno tappezzando il Paese *(Commenti)*, date avvio a un dibattito su modifiche costituzionali che hanno il preciso compito di snaturare i poteri del Parlamento, il vero luogo della democrazia pensato e voluto dai nostri Madri e Padri costituenti, dopo la tragedia del ventennio fascista che anche in quest'Aula molti senatori dimenticano quasi ogni giorno. *(Applausi)*. Siamo qui a Siamo qui a discutere di una riforma costituzionale che in nessun modo affronta i problemi urgenti e le difficoltà in cui versa il Paese e anzi ne preannuncia l'aggravamento per la confusione istituzionale che comporta. Una riforma ispirata esclusivamente ad una concezione della politica propria della destra, che in questi ultimi anni ha tentato più volte, con diverse alleanze politiche, di modificare, se non sovvertire, le fondamenta del nostro sistema democratico. Il premierato in versione Meloni svuota il ruolo e le prerogative del Presidente della Repubblica e annulla la centralità del Parlamento quale sede della rappresentanza democratica del popolo. Questa frase l'hanno ripetuta praticamente tutti i miei colleghi. Siamo anche andati a ripeterla continuamente nella Commissione preposta, perché siamo convinti che ripetendola in quest'Aula qualcuno ci ascolti e qualche germe di quello che diciamo diciamo entri come consapevolezza nei loro cervelli. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio, come sostengono autorevoli commentatori, prosciuga la figura, le funzioni e l'autorevolezza del Presidente della Repubblica, elementi essenziali nel nostro sistema per garantire l'equilibrio e la tenuta del sistema costituzionale e - voglio sottolinearlo con forza - per l'unità del Paese. Non è sfuggito ai più che la ministra per le riforme Alberti Casellati insiste ad affermare che si può eleggere direttamente il *Premier* senza indebolire il Presidente della Repubblica come figura *super partes* e di garanzia. Debbo rilevare con rammarico che dire questo significa semplicemente arrampicarsi sugli specchi e sostenere l'indifendibile. La ministra Alberti Casellati lo ripete ogni giorno, così come voi,

è che le due cose non possono stare insieme e la ragione è molto facile da capire: l'elezione diretta del *Premier* fa saltare l'equilibrio costituzionale oggi esistente tra Capo dello Stato e Presidente del Consiglio, eliminando il voto di fiducia iniziale del Parlamento al Governo e comportando la non sostituibilità del Primo Ministro ad opera del Parlamento. State cercando di creare un sistema istituzionale che non esiste in nessun Paese al mondo e che mortifica fortemente sia il Presidente della Repubblica che il Parlamento, perché priva di fatto e di diritto entrambi questi organi di funzioni essenziali per salvaguardare il delicato Siamo rammaricati, perché ci eravamo detti disponibili a ragionare insieme su una riforma complessiva del sistema di governo. Del resto le regole si fanno tutti quanti insieme. Avevamo avanzato disponibilità su un rafforzamento che garantisse maggiore stabilità ai Governi, ipotizzando l'introduzione della fiducia costruttiva, oltre che la possibilità che le liste elettorali recassero addirittura anche anche l'indicazione del Presidente del Consiglio proposto. Tuttavia nessuno ha mai neanche immaginato che si potesse arrivare a discutere di una proposta che prevedesse di togliere funzioni al Capo dello Stato e neutralizzasse il Parlamento. Nessuno di noi lo avrebbe mai pensato. La riforma della Presidente del Consiglio, invece, risponde esclusivamente a un desiderio che soverchia ogni riflessione costituzionale. È una riforma che asseconda il desiderio peggiore,

i princìpi con cui si esercitano i poteri democratici. La destra sta tentando di farlo già adesso, con l'aumento della forbice tra poveri e benestanti, annullando la maggior parte delle garanzie per le classi svantaggiate. In questo sì del Consiglio Meloni sta truffando i suoi elettori, perché è vero che noi stiamo assistendo alla riduzione dei diritti dei lavoratori. Penso, per esempio, alla scelta disumana di favorire la sanità privata affossando quella pubblica, gratuita e universalistica, anche se non c'era scritto nulla sul programma di Meloni sulla sanità; alla negazione del diritto all'aborto, ai manganelli contro chi dissente, come è avvenuto a Pisa, la mia città: quelle ferite non si sono ancora rimarginate. alle compressioni della libertà di stampa invocate per legge e all'appropriarsi del servizio pubblico televisivo, ormai da noi e da tutti soprannominato tele-Meloni. alla sottomissione del potere giudiziario a quello politico, a partire dalla separazione delle carriere. Tutto ciò è comandare e non governare, sottraendo spazio a quella cultura del dialogo che ha segnato positivamente il nostro sistema istituzionale dal Dopoguerra ad oggi. Comandare, un verbo caro anche al vice presidente del Consiglio Salvini, che non molto tempo fa chiedeva per sé pieni poteri, mentre si divertiva a suon di musica e *mojito* in spiaggia. Pieni poteri che gli italiani, con il voto, giustamente non gli hanno concesso. Siamo qui a discutere di una riforma che la destra vuole approvata in Parlamento prima del voto europeo, per poter sbandierare ai propri simpatizzanti, a quelli cui piace l'uomo - ora la donna soli al comando, il raggiungimento di un risultato identitario. Ricordo, però, a questa maggioranza che nel Paese siete minoranza, indiscutibilmente minoranza. Vi ricordo che la somma delle opposizioni in Parlamento e i tanti che non sono andati a votare alle ultime elezioni politiche è ben più consistente del consenso che avete ricevuto e che è già in parabola discendente.

ostacolando il lavoro delle Camere, accelerare il voto, per poter dire che avete ottenuto quel che volevate. Quanto ci costerà questa pervicacia, finalizzata esclusivamente a un interesse di parte? Con contraccolpi negativi sui nostri equilibri costituzionali costituzionali e quindi sulla nostra democrazia, rilevati da quasi tutti gli esperti e studiosi della nostra legge primaria. passerà al vaglio del *referendum*, ma, per garantire l'appoggio di tutto il centrodestra in Parlamento, essa è stata barattata, dal partito del Presidente del Consiglio, con l'approvazione, da parte delle Camere, della legge ordinaria sull'autonomia differenziata, promossa dalla dalla Lega ed elaborata dai suoi teorici della prima ora, per affermare la supremazia del Nord sul resto d'Italia. L'autonomia differenziata sarà una catastrofe, perché comporta lo smantellamento dell'unità d'Italia, aumentando il divario tra Regioni ricche e povere, tra sanità efficiente ed assenza di cure, tra risorse certe per le Regioni sviluppate, derivanti dalla fiscalità, e altre Regioni già condannate da economie al nero. Una legge pensata per cristallizzare le diseguaglianze e non per combatterle. Signor Presidente, la genesi stessa della Lega in qualche modo lasciava prevedere il progetto di dividere la nostra Nazione. Si chiamava Lega Nord, aveva il culto del dio Po, di Alberto da Giussano e, senza vergognarsi, invocava la secessione. Sono tornati lì, anche se, nel frattempo, il lemma Salvini ha sostituito la parola Nord. Per il partito del Presidente del Consiglio, però, quel che accade ha il sapore del paradosso. Il partito si chiama Fratelli d'Italia, non Fratelli del Nord Italia o Fratelli del Sud Italia; ha sempre riconosciuto e anzi esaltato l'Italia unita, un'unica Italia. Ma, allora, come fa chi è di quel partito a sopportare e ad accettare quel patto scellerato che, alla fine, non porterà a nessuna riforma costituzionale, perché il *referendum* la boccerà? lascerà le macerie di un Paese spezzettato e diseguale, per volontà di chi ha un consenso saldo e ora in declino solo in una parte del nostro Paese. Dopo il negazionismo del fascismo, volete anche la negazione del Rinascimento? Dovreste avere almeno un sussulto di dignità. Noi, invece, non permetteremo che questo accada. Continueremo a contrastare questa riforma scellerata, in quest'Aula e nel Paese, con gli strumenti della democrazia e della Costituzione, che restano il nostro riferimento e i nostri valori non negoziabili. Signor Presidente, gentile rappresentante del Governo, colleghe e colleghi senatori, pubblico che ci segue da casa e dagli spalti, per cultura e per formazione sono orientata alla concretezza, che rifugge dagli stereotipi e, quindi, non mi sono mai appassionata troppo all'importanza delle definizioni, anche a quella dell'antifascismo, non foss'altro perché - sia ben chiaro - lo ritengo un fatto scontato, che non può essere neppure messo in discussione. Un anno e mezzo di questo Governo, in realtà, mi ha fatto riflettere non poco su questo tema e mi ha fatto ricredere, partendo dal presupposto che certamente il fascismo è stato espressione di autoritarismo e che un Governo che esercita il potere in modo autoritario ben può riportare alla mente una drammatica ventennale esperienza di Governo passata e cassata dalla storia. Ciò premesso, alla luce di quanto sta accadendo negli ultimi mesi con questo Governo, devo dire di essere preoccupata. E sono preoccupata dal contenuto delle leggi approvate, dal metodo con cui vengono approvate (decretazione d'urgenza e fiducia), dall'assenza di ascolto e di un vero dialogo e di un confronto, fino alla modifica della Costituzione, nella direzione dell'accentramento del potere in capo al Presidente del Consiglio, una singola persona, invece di condividerlo con il complesso ecosistema del Parlamento. Prima ancora che nel merito, la mia critica va al metodo, perché sappiamo che soprattutto in politica la forma è sostanza. Una modifica costituzionale di cotanta portata necessiterebbe di un percorso condiviso con tutte le forze politiche in Parlamento, secondo il principio giuridico che un atto si modifica con la medesima forma con cui è nato, e la Costituzione è nata con un'Assemblea costituente, espressione di un approccio democratico. Direte che è già accaduto che una riforma costituzionale sia stata licenziata a maggioranza, ma è altresì noto che sia rimasta inapplicata. Bisognerebbe quindi saper fare tesoro degli errori del passato. Se l'intento della riforma è quello di garantire maggior stabilità ai Governi, bene, lavoriamoci insieme per partorire un progetto condiviso e ponderato da un serio confronto. Quello che vi sfugge è che state legiferando solo dal punto di vista della maggioranza, creando i presupposti affinché questa in futuro abbia la strada spianata a governare con prepotenza, eliminando gli ostacoli sulla strada e i contrappesi all'accrescimento dei poteri del Presidente del Consiglio e mettendo in discussione la separazione tra potere esecutivo e potere legislativo. Un esempio per tutti è il potere del Presidente del Consiglio di sciogliere le Camere a fronte di un voto di sfiducia, cioè o state con me o andate tutti a casa. Purtroppo abbiamo già sperimentato come l'uomo possa essere opportunista sino al punto di divenire malvagio e nella nostra Costituzione ci sono gli antidoti affinché una tale degenerazione del potere non possa accadere e non possa ripetersi. Ho l'impressione, care colleghe e cari colleghi, che questa partita vi stia già sfuggendo di mano. Questa rischia di essere una deriva antidemocratica, che crea l'ingresso in una spirale pericolosa. Quindi, rivolgo un richiamo alle colleghe e ai colleghi senatori di maggioranza ad una pausa di riflessione per ponderare l'opportunità di cambiare metodo di aprire ad un'Assemblea costituente o a un tavolo per addivenire a una proposta democraticamente condivisa dal Parlamento. Mi rivolgo al pubblico che ci segue e a tutti quegli italiani che, schifati dalla politica, non vanno a votare: attenzione, vi conviene alzarvi da quel divano e andare a votare, perché qua la situazione non è rosea. In ogni caso, questa vostra iniziativa di maggioranza dovrà passare al vaglio diretto degli italiani con un *referendum.* In più di un'occasione gli italiani hanno dimostrato di essere più attenti di quello che i governanti di turno pensavano e non credo che vogliano essere governati da un re Giorgia in delirio di potere. Grazie, credo che i colleghi senatori del mio Gruppo, ma anche quelli di altri Gruppi di opposizione, con serietà e con consistenza di argomenti, dimostrato e rappresentato le motivazioni forti per le quali ci opponiamo in maniera dura e determinata al provvedimento

punto: quello in cui stiamo facendo questa discussione, che riguarda le fondamenta dell'impalcatura democratica e costituzionale del nostro Paese, è un momento in cui la democrazia è in crisi ed è anche sotto attacco. Onorevoli colleghi, cos'è la democrazia? Lo sappiamo, lo sapete, ma ricordiamolo. È un sistema di Stato e di regolazione della convivenza che appartiene soltanto all'8 per cento della popolazione mondiale: l'8 La democrazia è un sistema giovane, a parte Atene, e non è solo minoritaria nel mondo, ma lo è anche nella storia del nostro Paese. Nel nostro Paese esiste dal 1945, nel 1946 abbiamo festeggiato la Repubblica, che continueremo a celebrare il 2 giugno, che viene dopo - è sempre bene ricordarlo, senza alcun riferimento polemico - il 25 aprile. Se non ci fosse stato il 25 aprile, non ci sarebbe stato il 2 giugno e non ci sarebbe stata neanche

La democrazia è in crisi, anche laddove esiste nel mondo. Con la precarizzazione e l'insicurezza che la parte negativa della globalizzazione ha provocato in centinaia e centinaia di milioni di famiglie nel mondo,

che, se la democrazia non le aiuta a risolvere i problemi, forse sarà meglio qualche altra soluzione semplificata. Posso capire - lo dico cercando di dare un contributo di riflessione, oltre che di dialettica tra maggioranza e opposizione - che qualcuno possa tifare per i repubblicani americani, rispetto ai democratici, in un sistema di grande democrazia come quella americana. Quello che però non è possibile è tifare per chi non c'entra niente con quel sistema e guida gli assalti a Capitol Hill, come Trump. La democrazia americana è in pericolo, anche per questi fenomeni e quelle manifestazioni, così come è in pericolo in America Latina, dove è capitato anche che abbia vinto un signore come Bolsonaro. Insomma, la democrazia è in crisi. Anche in Italia fatichiamo. Anche in Italia la democrazia deve essere irrobustita, perché non è una conquista per sempre

svolga un ruolo fondamentale, oggi di opposizione e domani di alternativa. Non sono però così cieco da non vedere che, tutti insieme, i partiti italiani non raccolgono neanche un milione di iscritti e invece aumentano fino a 7 milioni gli iscritti negli albi del volontariato. Quindi, intendo intendo dire che c'è bisogno di rinsaldare un patto tra cittadini e democrazia. E c'è bisogno di dare risposte sociali, innanzitutto, alle fragilità e alle diseguaglianze, per avvicinare i cittadini e il popolo alla democrazia, rafforzando un nuovo patto. Al tempo stesso, però, c'è bisogno che la democrazia prenda le sue decisioni, rafforzi il tema della democrazia partecipata, ma al tempo stesso insieme, non in contrapposizione della democrazia che decide. Al tempo stesso i partiti, le istituzioni devono aprirsi, rinnovarsi e far sì che quella parte di popolo che si sente esclusa possa invece ritrovare le ragioni di fiducia.

dovremmo pure fare qualcosa; dovremmo trarre le conseguenze da questa cosa; dovremmo procedere a una riforma delle istituzioni seria e a una riforma anche dei partiti. In questo senso si citava prima: noi abbiamo qui, per esempio, una proposta di applicazione dell'articolo 49 della Costituzione Insomma, è questo un momento drammatico, aggravato dal contesto internazionale di guerra. A proposito di crisi della democrazia, non ci dimentichiamo una intervista che Vladimir Putin rilasciò al «Financial Times» nel 2019, 2019, e in Italia, in due pagine lo stesso giorno, la pubblicò il «Corriere della Sera», quando il dittatore russo annunciò che la democrazia era finita, annunciando un nuovo ciclo di espansione delle democrature dell'autoritarismo, che vediamo poi anche con le armi e l'invasione in Ucraina.

una proposta seria, che avesse coinvolto tutto il Parlamento e non solo, anche aprendo un dibattito all'esterno. Il Partito Democratico sarebbe stato disponibile. Abbiamo presentato con i nostri emendamenti, con la discussione in Commissione, coerente con le decine e decine di audizioni dei costituzionalisti e di altri soggetti, delle proposte che vanno in una direzione di riformare le istituzioni, di rendere più stabili i Governi, di rendere la democrazia parlamentare più efficace e funzionale. Abbiamo presentato proposte che avvicinano il popolo alle alle istituzioni democratiche. Ma voi avete reso il confronto totalmente impossibile. Voi avete presentato in un patto - definirlo scellerato credo sia tra la Lega, con il totem dell'autonomia differenziata che renderà più deboli chi è già più debole oggi, e Fratelli d'Italia, una proposta del premierato che colpisce alla base la sovranità parlamentare e colpisce al cuore il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica e, infine, un'idea della giustizia, quella il cui vessillo è portato da Forza Italia, che francamente rischia di colpire al cuore la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura. Permettetemi di dire che ne abbiamo avuto un esempio ieri: non si è mai visto un Ministro della giustizia in carica che critica un provvedimento di una procura *(Applausi)*. Il Ministro può, se vuole, ordinare le ispezioni, ma non si deve permettere il Governo di colpire l'indipendenza della magistratura. *(Applausi)*. Ecco perché dicevamo prima che un conto è aver vinto le elezioni e un conto aver preso il potere. Voi date l'impressione di avere preso il potere e così non può esserci dialogo. Noi combatteremo con tutte le armi democratiche fino alle estreme conseguenze, eventualmente dei *referendum*, anche se anche se io sono convinto - è una convinzione mia, naturalmente mi posso sbagliare - che, passate le elezioni europee, sarete costretti a parlare in termini diversi sia di autonomia differenziata - come dicevo prima,

delle pericolose riforme annunciate nel settore della giustizia. Ne parlerete in termini diversi e non so se sarà perché i risultati delle elezioni europee non andranno nella direzione che voi auspicate, e mi auguro naturalmente che non vadano in quel modo. Penso che queste riforme sanno molto di un patto preelettorale destinato a venir meno e a sciogliersi dopo il voto, perché non ci sarà più

lo dicono in tanti più autorevolmente di me - di definire drammatico per la democrazia nel mondo e anche difficilissimo per la democrazia nel nostro Paese, si può Si può non capire a che altezza bisognerebbe lanciare la sfida? Se l'aveste fatto, il Partito Democratico ci sarebbe stato e sarebbe stato pronto a confrontarsi. Anche dal vostro interno qualcuno - penso alle posizioni del senatore Pera - ve l'ha detto, ma ve l'hanno detto anche autorevoli commentatori, non certamente della sinistra. Voi avete rifiutato questa cosa e per noi è uno schiaffo non all'opposizione, ma al Paese e di questo credo porterete una grande responsabilità. nel Meridione il tasso di occupazione è più basso rispetto al Centro e al Nord. Donne e giovani pagano un costo elevato e sono tanti coloro che a malincuore lasciano la terra d'origine, accentuando un rischio di spopolamento che andrebbe frenato. «Lo sviluppo della Repubblica ha bisogno del rilancio del Mezzogiorno» e «Una separazione delle strade tra territori del Nord e territori del Meridione recherebbe gravi danni agli uni e agli altri»: a pronunciare queste parole è stato qualche giorno fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È un segnale chiaro e inequivocabile - hanno chiosato diversi analisti politici - di come il Capo dello Stato abbia messo in guardia l'Esecutivo sui rischi connessi all'accelerazione di ulteriori forme di autonomia. Il Capo dello Stato, il nostro Capo dello Stato, non il vostro, quello che volete derubricare a semplice passacarte è il baluardo della tenuta democratica del nostro Paese, il garante dell'unità nazionale, un vero e proprio porto sicuro per 60 milioni di italiani. Oggi questa maggioranza vuole minare la sacralità di siffatta figura e la garanzia che essa offre, minando le fondamenta che sorreggono la nostra Repubblica. A tale proposito vorrei ricordare uno stralcio di un celebre discorso effettuato da Pietro Calamandrei a degli studenti negli anni Secondo il Padre costituente «(...) la costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità». Da rappresentante istituzionale mi scuso con i Padri costituenti della Patria per il vostro disegno eversivo messo in campo da questo Esecutivo, che sta letteralmente umiliando e calpestando il sudore e il sacrificio che hanno gettato le fondamenta della nostra democrazia. È infatti ormai evidente che, con l'accelerazione di ulteriori forme di autonomia e con il premierato, il Governo Meloni ha deciso di cambiare il volto della nostra Carta costituzionale nata dal sangue della Resistenza. Non posso che fare mie le parole del professore Enzo Cheli, Vice Presidente emerito della Consulta, secondo cui molti elementi del premierato indurrebbero a pensare che si tratti di un primo passo verso una svolta diametralmente opposta alla storia e allo spirito che animò il nostro impianto repubblicano e antifascista. Pertanto invito i colleghi della maggioranza a leggere le memorie depositate presso la 1a Commissione del Senato e ad approfondire i pareri, gli studi e le riflessioni dei più grandi costituzionalisti italiani, che hanno letteralmente demolito questa riforma del premierato nelle audizioni parlamentari. Ciò che traspare è un tentativo palese e pericoloso di ingabbiare il Colle. Sì, lo ripeto: l'obiettivo è di dare i pieni poteri a una persona sola al comando; lo hanno detto quasi tutti i nostri rappresentanti qui finora ascoltati. Pertanto Pertanto ciò che traspare è un tentativo palese e pericoloso di ingabbiare il Colle. Ci sono alcuni passaggi di questo testo che davvero imbrigliano il Presidente della Repubblica, relegandolo a una figura ancillare e di ratificatore. Mi chiedo se Giorgia Meloni abbia letto, ad esempio, le memorie del professor Ugo De Siervo, giurista e presidente emerito della Corte costituzionale, che, dopo aver aspramente criticato questo provvedimento, ha chiosato: sempre nel nuovo articolo 92 che il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto (...)" e successivamente che "il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo (...) quasi che egli potesse fare altrimenti"». Questo passaggio sintetizza il ruolo che andrebbe ad avere il Capo dello Stato, ovvero quello di semplice passacarte. E questo noi non lo possiamo accettare. È una vera vergogna. Fossi in voi, proverei un forte senso di imbarazzo, anche per lo scambio politico-elettorale che ha di fatto attaccato la spina a questo provvedimento, cioè il baratto tra l'autonomia differenziata e il premierato o, meglio, tra la riforma spacca Italia e la riforma spacca Costituzione. Pur di portare a casa il risultato, Fratelli d'Italia sta consentendo alla Lega di creare una nuova Repubblica Cisalpina. Vi ricordo che la Lombardia percepirà 106 miliardi in più, il Veneto 41 e l'Emilia-Romagna 43, creando cittadini di serie A e cittadini Inoltre, cito ancora a proposito le parole del professor Walter Obwexer, ordinario di diritto internazionale pubblico all'Università di Innsbruck, che, in sede di audizione parlamentare, ha riferito chiaramente che il nuovo premio di maggioranza del 55 per cento, previsto per entrambe le Camere del Parlamento a favore delle liste di candidati collegate al Presidente del Consiglio dei ministri, potrebbe ridurre il numero dei rappresentanti delle minoranze linguistiche eletti in Alto Adige in entrambe le Camere, a meno che i rappresentanti delle minoranze linguistiche non si colleghino con la lista del Presidente del Consiglio eletto. Perciò il combinato disposto autonomia regionale differenziata e premierato sono nefasti per l'intera Nazione e questo rappresenterebbe un chiaro limite nel criterio di rappresentanza delle minoranze, anche settentrionali. Onorevoli colleghi, mi rivolgo a voi con profonda preoccupazione, innanzi a questo disegno di legge costituzionale presentato in maniera affrettata e inopportuna, durante un periodo così delicato come la campagna elettorale per le elezioni europee. Questo provvedimento non solo minaccia di compromettere la struttura fondamentale del nostro Stato, ma rappresenta anche un chiaro affronto alle istituzioni democratiche, che sono il pilastro della nostra società. Il concentrarsi eccessivo dei poteri nella figura del *Premier*, come proposto da questo provvedimento, rischia seriamente di compromettere l'equilibrio delicato tra i diversi poteri dello Stato, mettendo a repentaglio la nostra democrazia. La centralizzazione e l'accentramento del potere esecutivo nelle mani di una singola figura, infatti, potrebbero portare a una perdita di controllo e di bilanciamento tra i poteri, mettendo a rischio la separazione dei poteri sancita dalla nostra Costituzione. Perciò ritengo che la maggioranza che sostiene questa proposta mostri un chiaro disprezzo per il ruolo e l'autonomia del Parlamento, indebolendo così il cuore pulsante della nostra democrazia rappresentativa. Vedete: l'accentramento del potere legislativo e l'indebolimento delle istituzioni parlamentari potrebbero compromettere la capacità del nostro sistema politico di rappresentare realmente gli interessi e le esigenze dei cittadini, minando così la legittimità e l'efficacia delle nostre istituzioni democratiche. Onorevoli colleghi, il fatto poi che un premio di maggioranza così ampio venga inserito in Costituzione rappresenta una minaccia per la nostra democrazia, superando addirittura l'indegnità di numerose leggi passate. Il rischio è di compromettere la capacità del nostro tessuto democratico di garantire una rappresentanza equa e proporzionale dei cittadini, mettendo a repentaglio la legittimità e l'efficacia del nostro sistema politico. non possiamo permettere che il nostro Paese cada vittima di manovre politiche che minano i principi fondamentali della democrazia. È nostro dovere porci interrogativi seri sulle reali conseguenze di questa riforma, mantenendo sempre presente che la sovranità appartiene al popolo, come sancito dalla nostra Costituzione, e non certo a Giorgia Meloni.

Durante i lavori di Commissione la Ministra ha reso una questione di principio il fatto di essere sempre presente e di interloquire

di aprire davvero un confronto. Non me ne voglia la Sottosegretaria, ci mancherebbe. Da un punto di vista formale - sia chiaro - non c'è violazione alcuna delle prerogative del Parlamento. Non sto facendo alcuna eccezione di carattere formale, registrando un aspetto che, vista la delicatezza del tema, meriterebbe di essere considerato. Noi, in 57 sedute di Commissione, abbiamo sentito ripetere dalla Ministra che lei intendeva ascoltare ogni intervento,

la sede della discussione della riforma è questa, e non un'altra. Io non voglio neanche immaginare che la Ministra sia assente, perché vuole confrontarsi sul premierato fuori dal Parlamento,

quelle vere, sono rispettate. Se invece si immagina che il confronto si debba svolgere in una sede extraparlamentare, io credo che i cittadini siano un po' meno sovrani e un po' meno rispettati. Chiederei a lei, Presidente, di condividere con gli altri Gruppi, in un clima naturalmente di condivisione, la sospensione dei lavori e il rinvio a quando la Ministra potrà essere presente e ascoltare - come ha detto di voler fare tutti i nostri interventi. Ciò per un problema di riguardo nei confronti del Parlamento e della fatica che fanno i senatori nell'argomentare in maniera seria e non ostruzionistica le ragioni e le preoccupazioni che abbiamo ascoltato fino ad ora nei confronti di questa riforma. Grazie, senatore. Riporterò queste sue osservazioni al presidente La Russa. Come lei ha osservato, il Governo è rappresentato in questo momento dal Sottosegretario. Il relatore è presente in Aula. Immagino che ci sarà sicuramente una replica

anch'io con quanto ha testé detto il senatore Giorgis. Ritengo che l'importanza di questo disegno di legge, senza ovviamente voler mancare di rispetto alla Sottosegretaria che è qui presente, richieda necessariamente la presenza della Ministra, che tanto ha ha sostenuto questo provvedimento in Commissione. Penso che sia fondamentale un'alta, la massima rappresentanza di chi ha voluto questa riforma e di chi l'ha firmata con il proprio nome qui in quest'Aula. Non è accettabile che i lavori procedano in questo modo, con una scarsa partecipazione dei colleghi di maggioranza, senza alcun intervento quest'oggi da parte loro, tranne poi mugugnare durante gli interventi dei colleghi dell'opposizione. Chiedo anch'io, come il senatore Giorgis, che si sospenda e si riprenda

che una delle principali critiche che viene mossa da noi e non solo da noi, ma direi da esimi costituzionalisti a questa riforma, è che essa svuota il ruolo del Parlamento

A volte non è una questione - lo dico alla senatrice che è appena intervenuta - di legittimità in base al Regolamento, ma c'è una cosa che si chiama opportunità politica, sensibilità istituzionale. E questo è il momento principe, il primo, di un dibattito che dovrebbe essere approfondito, articolato e anche franco. Non ci si spaventa nel Parlamento di un dibattito che è

e si sta gloriando di questa riforma costituzionale, la dice lunga sul rispetto nei confronti delle istituzioni parlamentari da parte ha scritto questa proposta di legge. *(Applausi)*. Questo si chiama *bon ton* istituzionale e non è una cosa per signorine: sono gli elementi e la cifra, la forchetta

nella nostra discussione. Devo dire che ho ascoltato con grande attenzione i pochissimi interventi che sono stati svolti oggi da parte della maggioranza. Ho frequentato la Commissione affari costituzionali durante il dibattito e la pur non essendo la mia Commissione. Ritengo di grandissimo interesse capire in modo approfondito e dettagliato come cambierà il nostro assetto istituzionale nei prossimi anni se mai questa legge dovesse passare, e io mi auguro di no e mi auguro che ci sia un ripensamento durante il percorso. Ma non erano presenti tutti i rappresentanti della maggioranza. Credo che sia questo, alla fine del lavoro che si fa nelle Commissioni di merito, il luogo in cui possiamo tutti renderci conto fino in fondo di qual è la nostra responsabilità nel Paese e questo è, tra l'altro, il cardine dell'articolo 67 della Costituzione che, se anche non viene toccato da questa norma, in realtà viene stravolto implicitamente. Come dicevo, ho ascoltato con attenzione gli interventi di oggi, ma anche gli interventi di ieri, quando abbiamo affrontato il tema della pregiudiziale, perché lì

il suo rappresentante, che il cittadino scelga il Presidente del Consiglio direttamente, scelga e decida chi lo governa. Ebbene, questo è il succo della domanda

Bisognerà capire se questa legge risponde veramente alle intenzioni di chi l'ha scritta o almeno alle intenzioni che sono state scritte. Mi riferisco in particolare alla alla questione che ha aperto in quest'Aula il Presidente del Gruppo Fratelli d'Italia, il senatore Malan, e che ha fatto anche adesso, da questo convegno, la ministra Alberti Casellati o che ci dice tutti i giorni la *premier* Giorgia Meloni. Io credo che questo sia l'equivoco di fondo, perché il tema di questa norma non è

vengono attribuiti di fatto poteri inimmaginabili in tutte le democrazie liberali. Tant'è vero che la forma di premierato (e questa specie di premierato all'italiana che verrà definito come il premierato Meloni) la stiamo sperimentando sul vivo della nostra pelle, con questo disegno di legge, soltanto adesso qui ora in Italia. È un *unicum* italiano, purtroppo un *made in Italy* di cui avremo poco di essere fieri. bisogna veramente vedere come è stata ribaltata la storia del dibattito istituzionale in Italia degli ultimi venti-trent'anni. È vero, infatti, che in tutte le forze politiche di questo arco costituzionale si è discusso più volte se per i cambiamenti operati in Italia, se per le trasformazioni del tessuto sociale e soprattutto per i cambiamenti politici avvenuti nel nostro Paese, anche all'indomani della riforma del Titolo V, che ha di fatto cambiato l'assetto delle istituzioni in Italia, fosse più opportuno fare un cancellierato alla tedesca, un semipresidenzialismo alla francese, oppure lavorare verso un sistema all'americana, un presidenzialismo puro, come aveva proposto durante la sua campagna elettorale la

occidentale, perché poi ci sono le cosiddette "democrature" di cui parlava prima il senatore Verini, dove la gente elegge sì, ma elegge un dittatore e questa non è democrazia, ma un'altra cosa. In tutte queste tre forme che noi conosciamo c'è una caratteristica:

ma ci sono delle forme di *check and balance* e cioè di pesi e contrappesi all'interno delle istituzioni che rafforzano il Parlamento,

queste democrazie mature, che hanno esplicato un diverso modello di rappresentanza parlamentare, con una rappresentanza di elezione diretta o facendo il Parlamento dei *Lander*, un po' in Germania, hanno tutte tenuto ben presente una distinzione del ruolo del Parlamento da quello del *Premier* o del Presidente, o il diverso rapporto tra Presidente e *Premier,* dell'autorità giudiziaria, e hanno investito il Parlamento di una forza politica e di controbilanciamento che tiene insieme l'equilibrio dei poteri e quindi garantisce la democrazia.

avete disegnato qualcosa di assolutamente inedito nello scenario delle democrazie occidentali. Questo non è un complimento vorrei che fosse molto chiaro. Non è un complimento il mio. E secondo il vostro testo, che cito, nella presentazione voi dite che l'Italia ha bisogno del premierato perché la forma di governo italiana è un modello di Governo parlamentare a debole razionalizzazione ed è ritenuta responsabile dei più variegati problemi, tra cui l'instabilità dei Governi, la eterogeneità e la volatilità delle maggioranze, il trasfughismo parlamentare.

Siccome non è sufficiente che il nemico sia la sinistra, rispetto alla debolezza della politica italiana, dell'incapacità dei partiti politici di rigenerare il sistema democratico, la maggioranza ha trovato un nemico nella Costituzione e nella forma di governo, mentre le proprie debolezze che non vengono minimamente né affrontate, né risolte in questo disegno di legge costituzionale.

al centro dell'ipotesi di modifica della nostra forma repubblicana, vi è appunto la riscrittura dell'articolo 59, che lega l'elezione del Presidente del Consiglio a quella delle nostre due Camere, che saranno formate per il 55 per cento da candidati collegati al Presidente del Consiglio. del Consiglio. I Ministri arriveranno dopo le elezioni, con nomina del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. In primo luogo, non si capisce perché il Governo debba ottenere la fiducia di una maggioranza che è formata da candidati collegati al Presidente del Consiglio, anche perché, se questa fiducia non arriva, il Presidente della Repubblica deve rinnovare l'incarico per un secondo tentativo; e se neanche il secondo atto di questa messa in scena sarà buono, il Presidente della Repubblica dovrà sciogliere le Camere. Insomma, o si ratifica la scelta del Presidente del Consiglio o i parlamentari vanno a casa. a casa. Se poi il Presidente del Consiglio cessa dalla sua carica, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo allo stesso Presidente del Consiglio dimissionario o ad un altro parlamentare a lui collegato; anche in questo caso, se la maggioranza rinnega il Presidente del Consiglio, si va tutti a casa. Questa non è una forma di governo democratica, ma è la mera introduzione di una carica collegata al successo di una tornata elettorale. A cosa servono, quindi, i parlamentari in questa forma di governo? Possono solo votare, a maggioranza, di andare a casa con il Presidente del Consiglio e null'altro. Che fine fa l'articolo 67? Come si coniuga questo con questa riforma? Il Parlamento non è più un contrappeso della democrazia, ma un'adunanza di militanti obbedienti e diligenti, che hanno un'evidente incentivo personale ad approvare l'esistenza di un Governo: altro che il principio di rappresentanza e di rappresentatività; altro che il ruolo di intermediazione tra la popolazione e il Governo; altro che ruolo di indirizzo dei partiti! Risolve forse il problema della stabilità questa riforma che avete incredibilmente messo in campo? No, essa introduce invece un elemento autoreferenziale, che incentiva i parlamentari ad assecondare il Presidente del Consiglio se vogliono conservare la loro carica: signori cari, zitti e buoni, sennò tutti a casa! E io li voglio ascoltare i dibattiti in questa sede quando ci saranno questioni dirimenti di coscienza, che coinvolgono l'etica, che coinvolgono il nostro futuro. Ma chi li farà?

i nostri Padri costituenti hanno voluto costruire una forma di governo repubblicana;

far questo servivano altri equilibri che potevano essere più o meno rigorosi e più o meno severi. alla fine questo Parlamento abbia dato delle risposte all'Italia e negli ultimi dieci anni lo ha fatto in momenti di crisi di cui non c'erano precedenti. Ora, prima di smontare tutto quello che è stato fatto di buono da gente che veniva dalla guerra e che aveva affrontato cose non banali, pensiamoci bene, non per retorica, ma per essere sicuri che stiamo offrendo gli strumenti giusti a queste nuove generazioni per affrontare un futuro molto incerto. Per affrontare questo futuro molto incerto, stiamo abbandonando delle sicurezze di diritti e libertà costituzionali che abbiamo disegnato con tanta fatica e con tanto sacrificio nella storia di questo nostro Paese. Signora Presidente, mi fa piacere che sia tornata in Aula la Ministra ad ascoltare questo dibattito che riteniamo così importante, perché riguarda il futuro dell'assetto istituzionale del nostro Paese. Penso che che avremmo potuto avere un dibattito su questo tema molto diverso da quello che stiamo affrontando oggi con questa contrapposizione così netta tra la maggioranza e l'opposizione, se solo si fosse davvero cercato un metodo di lavoro e di dialogo diverso, che penso sarebbe stato doveroso, trattandosi di una materia - quella delle riforme istituzionali - sulla quale bisognerebbe almeno fare lo sforzo di trovare un minimo di terreno d'intesa e di condivisione. Tale sforzo non c'è stato onestamente, perché non si può considerare tale un unico incontro con le forze di opposizione, dopo il quale non c'è più stata alcuna interlocuzione, perché questo è stato quello che è successo. Penso invece che si sarebbe potuto cercare di trovare un minimo di terreno d'intesa, tenuto conto del fatto che del fatto che nessuno di noi, a mio parere, contesti il fatto che sia opportuno intervenire per migliorare il sistema istituzionale del nostro Paese. Saremmo ipocriti se non lo riconoscessimo: è almeno da quarant'anni che si fa una discussione su questo, sulla necessità di ammodernare l'architettura istituzionale del Paese. Noi stessi ci abbiamo provato negli anni scorsi, come sappiamo, con una riforma che cercava di affrontare alcuni nodi pacifici del malfunzionamento del nostro sistema. Mi riferisco intanto al nostro sistema bicamerale paritario, che oggi è tanto disfunzionale da essersi trasformato in un sistema sostanzialmente di monocameralismo alternato,

una volta che l'altro ramo lo ha esaminato, l'altra Camera è costretta, di fatto, ad approvarlo così com'è, senza emendamenti. Questa è una prassi talmente invalsa

obbliga a questa navetta i provvedimenti e non garantisce la necessaria efficienza a sistema. La nostra riforma cercava di affrontare quindi quel tema, perché obiettivamente è largamente condiviso,

questo caso la nostra esperienza di parlamentari credo lo possa attestare senza discussione). Mi riferisco alla mancanza da parte del Governo di uno strumento che gli consenta di attuare il proprio indirizzo politico nelle Assemblee legislative, che comporta la necessità di abusare dell'unico strumento che oggi è utilizzabile per quell'obiettivo, che è la decretazione d'urgenza. si tratta di uno strumento che dovrebbe essere utilizzato in casi straordinari di necessità, ma oggi è diventato quasi un'abitudine legislativa dei Governi che si succedono nel Paese. Non parlo di questo in particolare, anche se sta raggiungendo dei *record* dal punto di vista numerico. Comunque anche i Governi precedenti hanno dovuto utilizzare questo strumento, perché non ci sono altri strumenti che consentano, garantendo al Parlamento di svolgere la sua funzione, di avere la possibilità di attuare il proprio indirizzo politico. Noi avevamo immaginato in quella riforma la legge a data certa, che è uno strumento che potrebbe contemperare questa necessità. Siamo arrivati al paradosso di decreti-legge che violano patentemente, in modo direi quasi esagerato, anche quei limiti che la legge, ma anche la Corte costituzionale, hanno cercato di porre a questo abuso della decretazione d'urgenza, tra cui un limite in particolare che è quello dell'omogeneità di materia. Voi sapete che la Corte costituzionale dice decreto-legge si può fare, ma deve riguardare una materia omogenea. Da questo punto di vista voglio provare a leggervi il titolo di un decreto-legge che abbiamo convertito in quest'Aula pochi mesi fa, il 4 ottobre 2023. Si trattava di un decreto-legge il cui titolo recitava: «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 105 in materia di processo penale, di contrasto agli incendi boschivi, recupero delle tossicodipendenze, salute e cultura, personale della magistratura e della pubblica amministrazione». Questo è quasi un prendere in giro i principi costituzionali che sono stati posti dalla Corte. Vuol dire che l'abuso di questo strumento è diventato talmente necessario, evidentemente, per il Governo e la maggioranza *pro tempore*, che addirittura si ridicolizzano i principi che ha cercato di porre la stessa Corte costituzionale. che c'erano e ci sono tanti temi sui quali penso che non ci sia una particolare distanza di vedute e sui quali quindi era possibile e sarebbe possibile lavorare insieme per cercare di trovare gli accorgimenti, anche di natura costituzionale, per ovviare a queste inefficienze. Voi avete affrontato invece altre questioni e vi siete concentrati sulla forma di di governo, però, come dicevo, con un metodo che penso sia profondamente sbagliato, cioè un'assenza totale di confronto, salvo un incontro unico con le opposizioni. Ricordo che

dopo che ci fu un accordo iniziale, quantomeno sullo schema di quella riforma, tra i due principali partiti di allora, ossia il principale partito di maggioranza e il principale partito di opposizione. Si tentò di fare questo questo accordo tra maggioranza e opposizione, tra i due principali partiti di allora, per condividere un impianto e una proposta. Poi per ragioni diverse e di natura politica quell'accordo naufragò, ma non tanto sul merito di quella proposta, bensì perché ci furono ragioni di dissenso politico che portarono a una decisione di non percorrere più quella strada. Questo per dire che in quella circostanza si tentò di trovare un terreno comune di intesa. In questo caso invece c'è solo una prova muscolare da parte della maggioranza. Si dice che la mediazione che è stata fatta è sul premierato, cioè che la maggioranza ha rinunciato al presidenzialismo che era nel programma elettorale ed ha optato per il premierato per venire incontro ai desiderata dell'opposizione. Francamente, non so quando l'opposizione abbia mai parlato di premierato nell'interlocuzione con la maggioranza, ma la mia impressione è che,

perché sapete che l'introduzione del presidenzialismo in questo Paese probabilmente sarebbe fortemente osteggiata. Ciò in quanto il presidenzialismo comporterebbe sostanzialmente l'eliminazione della figura del Presidente della Repubblica, alla quale invece gli italiani sono particolarmente affezionati perché hanno visto il ruolo che ha avuto anche in questi anni. Quindi avete detto: facciamo il premierato, così così quando andremo davanti agli italiani potremo dire che il Presidente della Repubblica non viene toccato, perché noi interveniamo solo sul Presidente del Consiglio (cosa non vera come dirò tra poco). Avete scelto questo *escamotage*

dove, dopo averla messa all'opera per qualche anno, sono precipitosamente tornati indietro

disattiva automaticamente) ...*a meno di forzare il sistema trasformandolo di fatto in un sistema presidenziale, che è quello che avete in testa voi. voi. Un *Premier* eletto direttamente dal popolo, se non ha la maggioranza in Parlamento, è un *Premier* azzoppato e il sistema non funziona. Questo è esattamente quello che è successo in Israele: il *Premier* veniva eletto direttamente, ma le maggioranze *pro tempore* potevano non essere in grado di supportare quel *Premier*. Allora voi cosa fate? Voi fate una forzatura, dicendo che approverete una legge elettorale che garantirà al *Premier* eletto nelle stesse elezioni direttamente dal popolo di avere la maggioranza parlamentare. Ma, attenzione, questo significa trasformare il sistema: non è più un sistema parlamentare, diventa un sistema presidenziale, perché c'è un Presidente che ha la maggioranza a sua disposizione e noi usciamo dal sistema, forzandolo in modo che diventi un sistema presidenziale.

che ha la possibilità di governare perché appunto è stato eletto direttamente dal popolo e quindi ha una fortissima legittimazione, che gli consente, anche se attraverso quel confuso meccanismo, alla fine di far cadere i parlamentari, nel caso in cui venga sfiduciato, questo è un sistema fortemente plebiscitario, nel quale il Parlamento è totalmente svuotato del suo ruolo e diventa una sorta di grande consiglio comunale. Chi ha esperienza di amministrazione locale

E noi possiamo permetterci che il Governo del Paese venga dato a una persona che ha questo potere anche nei confronti delle maggioranze parlamentari? Guardate che nei sistemi presidenziali i *check and balance*, cioè gli equilibri per evitare che ci sia una concentrazione di potere nei confronti della persona che viene eletta direttamente, sono fortissimi. Il Parlamento americano è il più forte Parlamento che esista al mondo, per compensare il potere che viene dato al Presidente degli Stati Uniti. C'è un Parlamento che è fortissimo, c'è un equilibrio straordinario in un sistema presidenziale puro. Voi qui introducete di fatto un sistema presidenziale senza alcun equilibrio, senza alcun riequilibrio; neanche ne avete voluto discutere. discutere. Ci sono altri modelli per garantire quella stabilità che avete tanto a cuore. Ce ne sono tanti, perché non ne avete voluto discutere? Perché non volete discutere di quelli sui quali noi abbiamo dato la nostra disponibilità? Guardate che la disponibilità che viene dall'opposizione significa che, il giorno che voi aprite davvero una discussione con l'opposizione, l'opposizione non può che essere lì a discutere con voi, perché l'abbiamo già dichiarato. Questo significa che c'è la possibilità, se solo lo si vuole politicamente, di portare a casa una riforma che dia stabilità al Paese, se solo lo volete, se solo volete abbandonare la prova muscolare, perché c'è disponibilità, da parte dell'opposizione, su alcune cose sulle quali si può ragionare insieme. Non capisco perché c'è questa prova muscolare e mi preoccupa il disegno che c'è dietro. Mi preoccupa perché insieme a quello - vedo anche altre cose, che francamente trovo che possano rischiare di mettere in discussione gli equilibri del Paese. Una democrazia si fonda sulla presenza di poteri e contropoteri, che devono essere bilanciati. Dicevo prima che il Presidente della Repubblica viene totalmente esautorato, perché ovviamente, di fronte a una legittimazione popolare del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica conta molto di meno e la sua opera di mediazione è molto ridotta e molto indebolita.

Se voi la demolite, voi mettete a repentaglio questa capacità di unificazione che c'è attorno a una figura così importante per questo Paese. È questa la ragione per cui io penso che questi disequilibri siano pericolosi e mi preoccupano perché si aggiungono ad altri progetti che io penso siano pericolosi. Oggi un membro del CSM, che è stato peraltro nominato da partiti che sostengono la separazione delle carriere in magistratura, ha detto in un'intervista che è molto preoccupato da quel disegno di separazione delle carriere perché lui ritiene che la separazione delle carriere porterà con sé la sottoposizione dei pubblici ministeri al controllo dell'Esecutivo. Lo ha detto un membro del CSM nominato da partiti che sostengono quella ipotesi. Io penso che abbia ragione e penso che questo sia un altro dei tasselli che rischiano di mettere a repentaglio uno dei poteri dello Stato che va salvaguardato nella sua autonomia e indipendenza come la magistratura. Così come mi preoccupano quelle norme, che ogni tanto fanno capolino nelle riforme che stiamo esaminando anche in Commissione giustizia, che

sono molto pericolose perché la libertà di stampa è un architrave della democrazia, come la definisce la Corte costituzionale.

di mettere a repentaglio l'autonomia e l'indipendenza dei pubblici ministeri, le norme che mettono a repentaglio la libertà di stampa, un po' mi preoccupo e vi invito a una riflessione sul punto.

tutti i presenti che avranno la pazienza e la voglia di ascoltarmi, ma soprattutto ringrazio la Ministra di essere tornata; grazie di essere tornata da noi ad ascoltare questi ultimi interventi. Vorrei inizialmente condividere con voi questa strana sensazione di *déjà vu* che ho in questo istante. Sapete quel fenomeno psichico che consiste nell'errata sensazione di aver già vissuto un avvenimento. Sì, proprio quello, proprio quella che è una situazione che io in realtà ho già vissuto. L'ho già vissuta nel gennaio del 2016, quando ebbi il privilegio di esprimere il mio parere su una riforma costituzionale che non condividevo e che, per dirla con le parole di allora del senatore Malan, qui presente: toglie la voce ai cittadini, permette di dare potere a pochissime persone libere di sprecare soldi dei cittadini per conquistare voti, ricchezza e appoggi personali. Bisogna dire no da adesso e ogni giorno fino a quando non ci sarà il *referendum* in cui gli italiani avranno l'ultima occasione per salvare la democrazia in Italia. Io stavo seduto lì, il senatore Malan era tre posizioni più in là; condividevamo parecchio tempo. Il senatore di Malan di allora era nel Gruppo Forza Italia-PDL, e diceva anche altro. Mi interessa oggi però far notare quanto, per queste parole, io fossi d'accordo con lui e sulle quali ancora oggi mi rivedo. Non so però se lui la pensi ancora così, visto che il disegno di legge che stiamo discutendo pone sostanzialmente nelle mani di una sola persona tutto il potere legislativo.*(Applausi)*. Per verificare di non essere in preda a quello che il senatore Lisei stamattina ha chiamato come odioso pregiudizio, ho provato a rileggere il disegno di legge, come se lo avessi scritto io, leggendo anche i molti documenti depositati dai costituzionalisti nelle audizioni in Commissione. Ho detto: sia mai che ho sbagliato a scrivere un documento brutto? Magari con quel parere dei costituzionalisti mi ravvedo e lo faccio meglio. Sono partito, quindi, valutando gli obiettivi dichiarati nella relazione al disegno di legge che sono trovare una soluzione a: instabilità del Governo, eterogeneità delle maggioranze, trasformismo parlamentare. condivisibili tutti questi obiettivi, si fosse aggiunto anche trovare una soluzione per l'astensionismo e riavvicinare i giovani alle istituzioni, sarebbe stato perfetto, cioè l'avrei votato e lo avrei scritto benissimo come lo avete scritto voi. Peccato che questo

l'abbassamento del *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica dal sesto scrutinio invece che al terzo. Un cambiamento epocale, si modifica l'articolo 83 e anche questo non mi pare precisamente attinente ai tre obiettivi. L'articolo 3 sopprime la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due Camere, quindi modifica l'articolo 88 della Costituzione. Sarà anche questo uno di quelli che risolvono i problemi? L'articolo 4 modifica la disciplina della controfirma degli atti del Presidente della Repubblica da parte dei Ministri, cioè si parla solo del Presidente della Repubblica fino adesso. Non saranno controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia, la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei *referendum*, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi. Questo sì che probabilmente sistemerà tutta l'instabilità del Governo. andiamo avanti. la previsione in Costituzione di un premio di maggioranza a livello nazionale, modificando così l'articolo 92 della Costituzione. Questo sistemerà tutto? Vedremo più avanti.

leggendo singolarmente gli articoli, mettendoli e confronto con gli obiettivi dichiarati, non mi pare che ci siano gli estremi per poterli raggiungere con questo disegno di legge. Ma siccome io non ho un odioso pregiudizio e siccome l'ho scritto io questo disegno di legge, vado avanti e spero di aver chiarito chiarito che invece gli obiettivi li raggiungo lo stesso. Temo, però, che voi stiate dicendo agli italiani che l'unico modo che avete voi di stabilizzare i Governi è quello di dare pieno potere ad una sola persona che sceglieranno loro. loro. Sarà però la sola maggioranza di chi andrà a votare a poter scegliere il Presidente del Consiglio, e tutti gli altri? E la stragrande maggioranza di chi non andrà a votare o voterà gli altri partiti? Pazienza. Peccato, inoltre, che da quasi due anni ci stiate dicendo che voi siete stati eletti dal popolo, siete un Governo finalmente politico e che governerete per cinque anni e che noi ci dobbiamo mettere l'anima in pace, ma se già è possibile governare ed essere legittimati dal voto popolare, perché volete cambiare il sistema? Andiamo avanti e permettetemi di rileggere, invece, questa perla che avete creato. L'articolo 7 recita che: «In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.». Nulla in contrario, sono d'accordo anch'io, lo voto subito. L'articolo prosegue stabilendo che: «In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.». Come si fa a dire, come ha fatto il senatore Lisei stamattina, che non si toccano e non si alterano i poteri del Presidente della Repubblica, quando lo si obbliga a sciogliere le Camere a comando, oppure lo si obbliga a dare il mandato ad un parlamentare eletto in collegamento col Presidente del Consiglio? Proviamo a fare un esempio pratico, visto che siamo tutti abbastanza pratici di quello che succede in Parlamento. Vince le elezioni una coalizione formata da due o tre forze politiche (scegliete voi, mettete anche i partiti che volete); il Presidente del Consiglio scelto dal popolo è un parlamentare di una delle due o tre

Capita però che, dopo qualche tempo, ci siano disaccordi apparentemente superabili, ma che portano comunque il Presidente del Consiglio alle dimissioni. Si aprono alcuni scenari: il primo è che il Presidente del Consiglio dimissionario obbliga il Presidente della Repubblica a sciogliere le Camere e questi le scioglie senza battere ciglio, alla faccia della separazione dei poteri. scenario il Presidente del Consiglio dimissionario chiede al Presidente della Repubblica di affidare un nuovo mandato a sé stesso; nel frattempo ha dimostrato alle altre forze politiche di coalizione di essere determinato a mandare tutti a casa e quindi che la minaccia è reale. Cosa faranno, secondo voi, le altre forze politiche e i loro parlamentari sotto questo ricatto? A voi la risposta. Nel terzo scenario, il Presidente del Consiglio dimissionario, invece, è una persona molto responsabile, decide di non ricattare - passatemi il termine colleghi - le altre forze politiche chiede al Presidente della Repubblica di affidare ad altro parlamentare eletto in una lista collegata l'incarico di formare il nuovo Governo. Il Presidente della Repubblica conferisce il mandato ad un parlamentare di una delle forze politiche che hanno espresso il precedente Presidente del Consiglio; questo questo parlamentare stringe accordi con altri, creando di fatto una nuova maggioranza, magari con un Gruppo di opposizione che abbia i numeri per sostituire una forza politica di maggioranza riottosa (scegliete voi anche in questo a chi assegnare la riottosità di volta in volta). Secondo voi quelli che ho elencato sono scenari impossibili? Direi di no. Avete evitato l'instabilità? Secondo me no. Avete evitato l'eterogeneità della maggioranza? Direi di no. Avete evitato il trasformismo? Neanche per sogno. Aspettiamo quindi al varco la legge elettorale che accompagnerà l'attuazione di questa modifica costituzionale. Vedremo come verrà scelto il Presidente del Consiglio: sarà scelto con due schede, due schede, una per il Presidente e una per la coalizione, oppure sarà scelto come un sindaco, con una scheda sola, collegato ad una coalizione, ovviamente senza ballottaggio, che voi tanto odiate? Presidente, per il suo tramite dico al senatore Malan che la legge elettorale che verrà fatta dopo avrà un'importanza fondamentale sulla tenuta di tutto il sistema, ma il sistema che avete creato con questo disegno di legge costituzionale non sta in piedi già così, perché non evita nessuno dei problemi che abbiamo, perché il problema è dato dalle forze politiche e basta. e basta. Pertanto, o le forze politiche si danno una democrazia interna, si scelgono i parlamentari con delle primarie, si scelgono dei parlamentari liberi e rafforzano la democrazia interna e quindi anche il Parlamento, oppure da qua non se ne esce. Potrete mettere tutte le norme costituzionali che volete, ma i parlamentari potranno, quando vorranno, andare dove vogliono, quando vogliono e fare il bene del Paese.

Questo non è un attacco politico, ma è un dato oggettivo, messo a nudo anche dalla pandemia. Il punto di non ritorno si è segnato nel 2001, quando la riforma del Titolo V ha creato tanti sistemi sanitari quante sono le Regioni italiane, acutizzando la sperequazione sanitaria. Basti pensare che solo nel 2017 quasi un milione meridionali sono emigrati al Nord in cerca di cure, con un trasferimento di risorse di 4,6 miliardi di euro. Il MoVimento 5 Stelle da anni sostiene la necessità di restituire allo Stato la cabina di regia della sanità nazionale. Ma sapete qual è stata la risposta? L'autonomia differenziata, che spingerà sempre più la sanità italiane verso un sistema privatistico. Ciò rinnega l'articolo 32 della Carta costituzionale, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Ancora una volta, nella sacralità di quest'Aula chiedo di rafforzare la sanità di prossimità. Inoltre, evidenzio che si è lasciato nel dimenticatoio il decreto ministeriale n. 77 del 22 giugno 2022, volto a supportare l'assistenza territoriale. Annuncio quest'oggi che ad ore depositerò un'interrogazione parlamentare in cui metterò a nudo anche un'altra grave distrazione del Governo, che è la mancata attuazione del DPCM del 12 gennaio 2017, che introduceva i nuovi LEA. Onorevoli colleghi, nel mondo si sta parlando tanto dei progressi della lotta contro il cancro. Da medico ricordo, e molti di voi lo avranno vissuto in prima persona, che la cura delle neoplasie è legata alla diagnosi precoce, la cui mancanza vuol dire l'inizio del percorso di una inesorabile cronicizzazione della patologia, di una qualità della vita scadente, di una marcata riduzione dell'attesa di vita. Ma qual è la situazione che si registra oggi in Italia? Una carenza di fondi per assumere medici e infermieri, un incremento dei viaggi della speranza dal Sud al Nord, una spirale di liste d'attesa infinite, che vanificano ogni tentativo di diagnosi precoce.

Presidente, così come ho scritto nell'interrogazione a mia prima firma, anche in quest'Aula chiedo al Governo di sapere le modalità attraverso cui il Ministero della salute intende garantire un eguale accesso alle cure lungo l'intero perimetro nazionale le tempistiche necessarie per l'introduzione dei nuovi LEA. Personalmente, ritengo urgente risolvere queste problematiche con una riforma strutturale che, *in primis*, dovrebbe portare ad una razionalizzazione della spesa e potenziare la riforma del sistema sanitario nazionale di cui un gioiello invidiato e copiato in tutto il mondo e che oggi assume le sembianze di un rudere sgretolato. Onorevoli colleghi, sia chiaro che il MoVimento 5 Stelle non chiede riconoscimenti di privilegi, ma solo il rispetto dei diritti di sessanta milioni di italiani. **Atti